Comunico che in data 25 giugno 2024 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate (1173)». Sospendo la seduta per qualche minuto. *(La seduta, sospesa

Signor Presidente, in questo intervento, che sarà uno dei più pregnanti della legislatura, le consegno il testo delle dichiarazioni che ho appena reso alla Camera dei deputati. Tornerò nel primo pomeriggio per il dibattito e le repliche.

Ne ha facoltà. finestra") **(ore 10,22)** (*Segue* SALVITTI). L'obiettivo che abbiamo di fronte e che non vogliamo assolutamente mancare è quello di accelerare e rafforzare l'attuazione degli interventi che porteranno alla riduzione dei divari territoriali e che saranno finanziati dalla politica di coesione 2021-2027. In questo percorso non possiamo non fare un passo indietro. La revisione del PNRR, tanto contestata e strumentalizzata dalle opposizioni, era nata dalla necessità di aggiornare e adeguare il Piano al mutato contesto internazionale. Il Governo, guidato da Giorgia Meloni, ha reso questa occasione un'opportunità per mettere a sistema tutti i programmi di investimenti finanziati con fondi europei. Il Governo ha lavorato tenendo ben presente l'unità strategica e avendo una visione comune, a differenza di prima. La riforma della politica di coesione è una delle sette nuove riforme inserite nella revisione del PNRR - rispetto al quale è bene ricordare che stiamo raggiungendo risultati straordinari, tant'è che siamo la prima Nazione che chiederà il pagamento della sesta rata - e rappresenta dunque l'ultimo tassello, l'ultimo pezzo di un mosaico ben più ampio. È parte integrante di un più ampio disegno strategico partito con la modifica della *governance* del PNRR e della politica di coesione, cui sono seguiti un decreto specifico rivolto alle politiche di coesione e per il Sud e un altro che perfeziona la revisione del PNRR. Nel dettaglio, il decreto legislativo riguarda quei programmi di investimento finanziati da 42 miliardi di euro di risorse europee e 32 miliardi di risorse nazionali per il suo ciclo di programmazione 2021-2027. Parliamo di ben 74 miliardi di euro di investimenti destinati a ridurre i divari territoriali. Se è vero come dimostrano tutti i maggiori indicatori economici - che il Sud della nostra Nazione cresce più di quanto fatto negli ultimi anni e in percentuale più del Nord, tanto da raggiungere un più 1,3 nell'ultimo periodo, come certificato, con questa riforma vogliamo assicurare il coordinamento tra gli interventi di coesione attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale. Epossiamo farlo solo promuovendo la complementarietà e la sinergia tra gli interventi della politica di coesione e gli interventi previsti dagli accordi per la coesione e dal PNRR. Finalmente tutti i principali strumenti di sviluppo e coesione vengono collegati all'interno del medesimo orizzonte strategico, per evitare sovrapposizioni inutili, inutili, grazie alla visione del Presidente del Consiglio e all'ottimo lavoro svolto dal Ministro. La riforma prevede l'individuazione di interventi prioritari in una serie di settori strategici condivisi con la Commissione europea. L'approccio di lavoro non è­ - come avvenuto finora quello dei finanziamenti a pioggia, trasformato molto spesso in mancette elettorali, bensì è un approccio orientato al risultato, con un Governo che ha una visione generale degli interventi da realizzare: rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi, che è anche la *ratio* del provvedimento che sfido chiunque a contestare in questo ambito. Parliamo di settori strategici, di risorse idriche, di infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, dopo anni di politiche ambientaliste illogiche che non hanno guardato alla tutela del nostro territorio, favorendo anzi lo spopolamento e l'abbandono di intere aree della nostra Nazione. Parliamo di rifiuti, di trasporti, di mobilità. Quello dei rifiuti è un settore che veramente grida vendetta, perché non riuscire a programmare sui propri territori un ciclo naturale dei rifiuti è una cosa pazzesca, se pensiamo che siamo nel 2024. Parliamo di energia, dopo aver pagato a carissimo prezzo la scelta di un approvvigionamento univoco che ci ha fatto scoprire totalmente dipendenti da chi poteva decidere da un giorno all'altro di girare un interruttore e farci stare senza alcun tipo di energia. Nel dramma del problema dell'approvvigionamento energetico, si nasconde però un'occasione unica, perché le crisi spesso portano con sé nuove opportunità: intanto, l'occasione di rimettersi in discussione e di non dare tante cose per scontate; l'Europa ha un problema di approvvigionamento energetico e il Mezzogiorno d'Italia ha un potenziale enorme come produttore di energia pulita. Significa per noi diversificare la produzione di energia non solo per noi stessi, ma per l'Europa intera. Con i giusti investimenti sulle grandi infrastrutture strategiche e sulla produzione di energia pulita, possiamo costruire un futuro e un pezzo di strategia per questa Nazione che guarda al domani, e in questo accordo di sviluppo e coesione c'è un pezzo di questa storia, di questa strategia. Ancora, parliamo di sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, l'unica strada percorribile per creare ricchezza, non certo assistenzialismo di Stato, che crea solo ed esclusivamente nuovo debito che non possiamo più sostenere, che qualsiasi Stato non può sostenere. Ogni riferimento al reddito di cittadinanza e al superbonus non è assolutamente casuale: basta leggere il *report* dell'Ufficio parlamentare di bilancio, perché dobbiamo ricordare che la ricchezza non la crea lo Stato, il lavoro non si crea per decreto, come la povertà non si abolisce per decreto. Il punto è che la ricchezza in Italia, come sempre, la fanno le aziende con i loro lavoratori e quello che devono fare le istituzioni è mettere quelle aziende e quei lavoratori nelle condizioni migliori di lavorare. Abbiamo perciò destinato risorse alle imprese, all'efficientamento energetico e alle infrastrutture strategiche fondamentali sul piano dell'energia e non solo. Abbiamo destinato altri fondi alla sanità pubblica e, dunque, le polemiche degli *agit-prop* di professione, di cui pure abbiamo dovuto leggere in questi giorni, sinceramente sono un po' fuori contesto e fuori dal tempo. Realizzare il coordinamento tra le amministrazioni centrali e regionali titolari è fondamentale. Le amministrazioni locali - come già dimostrato dal Governo che sosteniamo con convinzione e determinazione­ - non saranno mai lasciate sole in questa sfida, anzi. Non mancherà, infatti, il rafforzamento della capacità amministrativa, prevedendo inoltre un meccanismo incentivante per il conseguimento degli obiettivi. Tradotto per chi non legge i documenti e attacca per partito preso: le amministrazioni regionali che rispetteranno i tempi godranno di un sostegno aggiuntivo da parte del Governo, per liberare ancora nuove e ulteriori risorse, preziose come l'ossigeno per i bilanci degli enti locali. È un'attenzione particolare che abbiamo dimostrato anche con la revisione del cosiddetto superbonus, dando la responsabilità ai Comuni

tra le Regioni e il Governo possa aver fatto saltare sulla sedia chi ha sempre guardato all'interesse di parte piuttosto che a quello dell'intera Nazione, ma con il Governo Meloni la rotta si è invertita ed è chiaramente tracciata. Capiamo che il definanziamento delle opere non realizzate faccia storcere il naso a qualcuno. Ma il caso dei poteri sostitutivi è un meccanismo di responsabilizzazione per noi tutti ed è un sistema che garantisce la certezza di non disperdere risorse estremamente preziose. il decreto-legge in esame definiamo la modalità di adeguamento dei programmi nazionali e regionali dei fondi di coesione della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa In questo modo vogliamo sostenere i programmi di investimento produttivo e di ricerca e sviluppo, anche e soprattutto se realizzati da grandi imprese in ambiti di particolare interesse strategico per la Nazione. Senza sviscerare il decreto-legge, ricordo che ci sono fondi destinati a interventi di recupero dei siti industriali, per la realizzazione di investimenti nelle aree industriali, produttive e artigianali localizzate nei Comuni superiori a 5.000 abitanti nelle Regioni del Sud Italia per la produzione di energia da fonti rinnovabili. finanziamenti potremo aggiungere ulteriori fondi per implementare l'accessibilità e la qualità delle infrastrutture di queste aree industriali e artigianali, rafforzando il sostegno all'insediamento di nuove attività produttive e non lasciando abbandonate a sé stesse aree industriali ormai dismesse. In questi giorni successivi all'approvazione della legge sull'autonomia differenziata abbiamo letto tante ipotesi non veritiere e assolutamente infondate. L'accusa più assurda e inverosimile è sicuramente quella che punta il dito contro il Governo, che avrebbe l'intenzione di spaccare l'Italia in Mai affermazione è stata più falsa, come dimostra anche il provvedimento in esame, che prevede il riequilibrio della dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno e dei servizi connessi. È stata, infatti, prevista l'istituzione di un fondo perequativo infrastrutturale, che vincola la destinazione al Mezzogiorno di una quota pari almeno al 40 per cento delle risorse. Il provvedimento interviene altresì sui programmi nazionali della politica di coesione, con l'obiettivo di rafforzare la trasparenza e l'efficienza delle programmazioni, stando ben attenti a quelle che possono essere infiltrazioni, anche di carattere mafioso, nella realizzazione dei lavori. progetti chiari e definiti per avvicinare le politiche di coesione agli italiani. Non va poi dimenticato il capitolo fondamentale del lavoro, in un momento storico nel quale registriamo il più alto tasso di occupazione e la discesa costante dei disoccupati, grazie soprattutto agli interventi in materia fiscale messi in campo dal Governo. Non mancano provvedimenti per sostenere l'occupazione e rendere più efficace il mercato del lavoro. In particolare, il Programma nazionale giovani, donne e lavoro registra una dotazione finanziaria di oltre 5 miliardi di euro. risorse saranno investite in misure che agevolano l'inserimento lavorativo rivolte sia all'attività di lavoro autonomo, imprenditoriale e liberoprofessionale, sia a creare una nuova occupazione stabile, con una specifica attenzione al Mezzogiorno. Con il *bonus* giovani, gli sgravi contributivi per l'assunzione a tempo indeterminato prevedono l'esonero del 100 per cento dei contributi nelle zone ZES per oltre ventiquattro mesi. Potrei elencare il *bonus* donne, in favore delle lavoratrici svantaggiate, che prevede allo stesso modo l'esonero

soprattutto per il bene dell'Italia e non della maggioranza, che guarda a una prospettiva di rilancio industriale della Nazione e, nello specifico, del Mezzogiorno. È la dimostrazione che questo Governo agisce concretamente nell'interesse pubblico. La riforma - come già detto in precedenza - mostra un *focus* particolare per il Sud e prevede, tra le altre cose, l'individuazione di interventi prioritari in una serie di settori strategici condivisi con la Commissione europea, secondo un approccio orientato al risultato. L'Italia ha a disposizione 75 miliardi di euro. In passato non tutte le risorse sono state spese. Noi abbiamo l'ambizione di spenderle e di spenderle bene, invertendo le negative tendenze che abbiamo registrato negli anni scorsi. dire che il voto da parte del nostro Gruppo è sicuramente favorevole rispetto al provvedimento in esame. Signora Presidente, colleghi, il mio ragionamento sarà diviso in due parti. La prima parte è relativa a un giudizio tecnico su quanto stiamo votando: un *potpourri* - lo definirei così - di provvedimenti, finalizzati al tema della crescita in senso largo, che reputo senza anima e senza strategia. Tuttavia, questa volta proverò a dirvi, per ogni titolo degli interventi su cui si misura il provvedimento, le ragioni per le quali lo reputo insufficiente, potrei dire "aria fresca". Dall'altro lato, invece, farò alcune considerazioni politiche sulle modalità con le quali si è giunti al voto di fiducia e sulle ragioni più profonde del perché, alla fine, questo Governo ricorre a un voto di fiducia su un provvedimento così banale. Questo è un atto che interviene, per esempio, sul tema delle risorse idriche. È un tema fondamentale, decisivo anche per il nostro Paese in ambito europeo, su cui concentrare certamente azioni di sistema, legate a questioni che hanno a che fare con interventi infrastrutturali molto seri, per esempio relativi al contrasto della siccità siccità e alla realizzazione di dissalatori. Sono due componenti chiave della soluzione del problema idrico. interventi da parte del Governo sul tema dei dissalatori, "*zeru tituli*", non c'è un investimento, non c'è un'azione da parte del ministro Pichetto Fratin in questa direzione. Ci sono dichiarazioni, proclami di ogni genere, di ogni tipo, ma il Paese continua ad essere in grande difficoltà. Interventi del Governo rispetto alla dispersione idrica: è una delle questioni più importanti sotto il profilo ambientale. Chi vi parla - lo sapete benissimo - non è un'ambientalista dogmatica, anzi io contrasto gli ambientalisti dogmatici, perché penso facciano tanto danno al Paese e all'Europa. Ma, per contrastare il tema della dispersione idrica, ci vogliono degli investimenti che hanno a che fare con una revisione strategica di pensiero e con

si sarebbero risolti i problemi del costo dell'acqua, bisogna che qualcun altro faccia mente locale, si renda conto che quella era pura demagogia e rimetta in piedi investimenti seri nel settore idrico, che non vedo. Qui ci sono i due poli del problema: da un lato, chi sposa teorie demagogiche sulla questione dell'acqua pubblica e, dall'altro, un Governo che magari si dichiara contro l'ambientalismo dogmatico, ma non fa nulla in termini di riforma per cercare di cambiare e fare ciò quello che sarebbe essenziale per investire sul tema della dispersione, che è una cosa drammatica. È una cosa gravissima che in un Paese come il nostro ci sia ancora circa il 40 per cento delle reti che perde acqua. E poi parliamo di ambientalismo!

Al di là dell'azione di primo intervento in emergenza, che avviene quando ci sono i disastri, noi vi stiamo dicendo dall'inizio di questa legislatura che è necessario dotarsi di una struttura che abbia una capacità sistematica di investimento per quanto riguarda il tema del contrasto al dissesto idrogeologico. Ciò significa fare infrastrutture, scolmatori e argini;

la possibilità di avere maggiore sicurezza. Il Governo Conte aveva smantellato il piano messo in campo dal Governo Renzi, cioè quello di Italia Sicura. A fronte di questa sbagliata iniziativa da parte del Governo Conte, noi abbiamo ripetutamente chiesto di trovare un'alternativa: se non vi piace il nome Italia Sicura, cambiategli nome; oppure, se non vi piace l'idea che l'abbia fatto Renzi,

che il contrasto al dissesto idrogeologico possa avvenire solo intervenendo a valle? Oppure non capite che gran parte dei problemi nascono per lo spopolamento delle aree interne e per l'impossibilità di avere azioni che favoriscano la permanenza delle persone e delle famiglie in quelle aree del Paese? Per fare ciò non serve romanticismo, dicendo alle famiglie che sarebbe bello vivere come gli Amish nelle aree interne del Paese. No: bisogna essere in grado di mettere in campo azioni economiche,

di quello che serve a questo Paese per evitare che le famiglie percorrano 40 chilometri, mentre basterebbe un piccolo ponte o un viadotto per collegare quella zona. Non ne parlate mai, né voi, né quell'altra parte del mondo politico, che invece si rinchiude dentro la comoda via di chi è già garantito e di chi non ha bisogno, perché magari vive nelle città dove esiste l'Alta velocità. In questo Paese il mondo si divide in due: quelli che hanno l'Alta velocità e quelli che non ce l'hanno. Quelli che non ce l'hanno sono italiani con meno opportunità, compresi i giovani. Se tu sei un giovane meritevole, capace con ottimi profitti scolastici, ma vivi in un territorio isolato e non hai le possibilità economiche per andare in un territorio che ha facoltà, scuole e licei migliori,

che non sono egualitarismo per tutti, ma sono pari opportunità per tutti. Questo dovrebbe essere il cuore di un ragionamento di riforma. Presenza di questi interventi in tema di dissesto idrogeologico e protezione dell'ambiente? Zero. Passo Siamo in un Paese che ha una produzione ormai alta di raccolta differenziata e con un divario tra Nord e Sud, sostanzialmente

Anche qui: questo è un Paese che ha smesso di pensare completamente a questa strategia, lasciando e consegnando il tema della politica sui rifiuti solo ed esclusivamente alla facoltà o alle opportunità che si aprono con le aziende di Stato, senza mettere in campo una politica che sia in grado di aggregare. E ciò vale per il gas, i rifiuti e l'acqua. poi il tema dell'attrattività sulle imprese. Anche in questo caso il decreto-legge differenzia le opportunità tra Nord e Sud, riproducendo in modo persino banale quello che in passato era già stato fatto e quindi non rileva, perché ogni azione di incentivo, se non è applicata una riforma seria e strutturale del sistema, non va molto lontano. Allora per quale motivo penso che avreste avuto bisogno di coinvolgere le opposizioni in un percorso di proposta e di miglioramento del provvedimento? Evidentemente la testa del ragionamento qui non c'è. qui non c'è. Allora, in questi casi, forse è preferibile avere l'umiltà - chiamiamola così - che è anche un'opportunità, di cercare di coinvolgere l'opposizione. Invece voi che cosa fate? Mettete la fiducia su un provvedimento che

Cominciate anzi ad avere serie difficoltà, perché avete provato mille strategie, persino il fatto di provare a contare qualcosa in Europa, e non avete portato a casa niente, niente, perché nell'ambiguità non si porta a casa niente. Nell'incapacità di avere un disegno di riforma del Paese, un Paese che ha una denatalità incredibile e una crescita zero, ci vuole un pensiero lungo e, quando il pensiero lungo non c'è, i nodi, nonostante le vittorie, nonostante il vento in poppa, nonostante i media a favore, cominciano a venire al pettine. Posso dire la mia? Con l'atto di oggi, costruito senza la possibilità di un voto misurato qui dentro, ma con una fiducia e con la discussione di oggi, si svolta. Oggi - segnatevi questa data - è un giro di boa per questa amministrazione perché, con la discussione europea che si terrà oggi pomeriggio, cambia tutto qui dentro: voi non ve ne rendete ancora conto, siete distratti con i vostri telefonini, ma - ahimè - ho la sensazione che il percorso di questo Governo e di questa maggioranza di questa maggioranza da oggi cambi profondamente. Voteremo contro la fiducia perché non si sottopone un provvedimento di così scarsa qualità al voto di fiducia. Voteremo contro la questione di fiducia, perché voi siete in una fase di debolezza e, di fronte alla vostra debolezza, da noi una mano non l'avrete.

e per il fatto che è stata messa la fiducia un'altra volta su un tema che vorrei sviluppare - già ieri ne abbiamo discusso - un tema che avrebbe meritato e meriterebbe un grande confronto. È indubbio che

Non è colpa di questo Governo se la situazione sta in questi termini. Proprio per questo andrebbe valutata tutta la questione in qualche modo, cercando di dare un contributo. Invece, si è posta la questione di fiducia di fronte alla disponibilità da parte delle opposizioni a discutere di merito, perché

questo fatto è avvenuto anche per le scelte di politica industriale. Vorrei sottolineare che lo Stato inventò l'IRI per lo sviluppo del Paese. Ho già citato, in quest'Aula, che addirittura il movimento operaio si è mobilitato per gli investimenti nel Mezzogiorno. Vorrei ricordare la più grande manifestazione dei metalmeccanici nel 1977 su questo indirizzo, proprio perché le scelte vanno fatte dal punto di vista della dimensione e quindi c'entrano le risorse. In questo caso le risorse oggi ci sarebbero. La responsabilità di questo Governo è che noi siamo di fronte al fatto che ci sono

per ridurre le differenze. E voi cosa proponete e fate? Questo non lo fate, da un certo punto di vista. Dall'altro lato, avete inventato l'autonomia differenziata.

di un Paese sostanzialmente unito e non diviso, non di venti staterelli che pensano di fare da soli. Perché dico questo?

per cercare di dare almeno un segno di inversione di tendenza. Questo è il dato fondamentale. Invece noi questo non lo stiamo facendo.

dei siti ambientali, in particolare di quelli siderurgici, che è stata posta in essere quando era sottosegretario Antonio Pizzinato. Vorrei ricordarvelo, perché la stessa legge Bagnoli l'abbiamo utilizzata a Sesto San Giovanni; oggi, dove c'era la Falck, si sta costruendo il

Quindi, non è un'invenzione di oggi. Però, guarda caso, magari in un posto ha funzionato, nel senso che è stata utilizzata. Oggi si sta costruendo il sistema sanitario pubblico

Vi sto citando fatti che sono successi in questo Paese e hanno prodotto delle buone pratiche o delle cattive pratiche. La cattiva pratica va modificata e cancellata, mentre la buona pratica si dovrebbe provare a estenderla. Ma dove sta?

la questione di fiducia, ma fare una discussione di merito. Le nostre opinioni possono essere benissimo contestate, ma almeno

per arrivare a un più puntuale utilizzo delle risorse destinate alle aree meno sviluppate del nostro Paese. Il percorso verso la riforma della politica di coesione collegata alla revisione del PNRR è necessario per dare un ulteriore impulso soprattutto alla crescita del Meridione.

Ci sono punte di crescita del PIL molto importanti in alcune Regioni meridionali, in particolare in Sicilia, dove si è raggiunto un 2,2 per cento. C'è una ragione di fondo che motiva la necessità di una migliore razionalizzazione della spesa; ossia quella di non perdere nemmeno un centesimo dei fondi europei. Lo si può fare dando unitarietà strategica e visione comune delle principali politiche di sviluppo e coesione, ed è proprio quello che cerchiamo di fare con questo decreto-legge. Non dimentichiamoci che stiamo discutendo dei fondi che finanziano gli interventi della politica di coesione degli anni che vanno dal 2021 al 2027. Un puntuale utilizzo di questi fondi significa ridurre i divari territoriali che purtroppo ancora ci sono, nonostante - come abbiamo evidenziato - ci siano alcuni elementi che fanno ben sperare in una crescita migliore. Il lungo lavoro della Commissione bilancio del Senato ha aggiunto 11 articoli agli iniziali 38, insieme a decine di ulteriori disposizioni. Gli interventi normativi riguardano i settori delle infrastrutture per il rischio idrogeologico, della protezione dell'ambiente, delle risorse idriche, dei rifiuti, dei trasporti, della mobilità sostenibile, dell'energia, della transizione digitale, della transizione verde, del sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese. Si tratta di una serie di programmi di investimento per complessivi 74 miliardi di euro, finanziati con risorse europee per 42 miliardi, alle quali si uniscono le risorse nazionali pari a 32 miliardi. La *ratio* del complesso di norme è quindi quella di arrivare a un più puntuale coordinamento delle politiche nazionali e di quelle regionali, posto che la politica di coesione deve essere attuata in piena sinergia fra Stato e e Regioni, una complementarietà degli interventi che deve riguardare sia gli accordi di coesione tra Stato e Regioni che l'utilizzo dei fondi del PNRR. Trattandosi di un testo corposo, si è prestato a una vasta attività emendativa. Sono entrate nel testo tante altre disposizioni che riguardano - ripeto - soprattutto il Mezzogiorno, ma in generale gli enti del territorio e in questo il lavoro dei senatori di Forza Italia è stato particolarmente attento e puntuale sul testo ed è riuscito a far approvare tutta una serie di misure che rendano l'articolato più puntuale ed efficace. Le nostre proposte sono state accolte dalla Commissione bilancio, in particolare per quanto riguarda la presenza dei rappresentanti delle Province nella cabina di regia del PNRR, ma sono stati anche considerati prioritari gli investimenti del Piano al PNRR (PNC), oltre agli investimenti per interventi di trasformazione digitale. Abbiamo proposto che la realizzazione degli interventi prioritari avvenga nell'ambito della rilevazione dei fabbisogni delle amministrazioni centrali, regionali e locali per rafforzarne la capacità amministrativa. È stata approvata anche una nostra proposta per la semplificazione della gestione della cassa vincolata. Ha già parlato ieri il senatore Occhiuto della modifica che è stata proposta da Forza Italia sull'assegnazione alla Regione Calabria delle risorse FSC per prevenire e mitigare il rischio idrogeologico, come come si è parlato delle disposizioni sui lavoratori portuali, sempre della Calabria, e la non applicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco sempre nella Regione Calabria. Abbiamo anche proposto di individuare per gli interventi nella ZES unica la centralità delle proposte delle Province, Città metropolitane o di Comuni sede delle Città metropolitane, così come sono state accolte le nostre modifiche al campo di applicazione dei crediti d'imposta nelle zone logistiche speciali in alcuni territori prima esclusi. Sono state accolte, ancora, le misure a supporto della struttura subcommissariale della Regione Puglia e inoltre l'istituzione di due fondi presso il MUR a favore di associazioni, fondazioni ed enti del territorio. Ancora, sono stati accolti i nostri ordini del giorno, tra cui quello che impegna il Governo ad abolire - questione molto importante - il redditometro, individuando un nuovo strumento per contrastare i grandi evasori. La norma del redditometro, secondo le indicazioni recepite positivamente anche dal viceministro Leo, dovrebbe entrare in uno dei prossimi decreti fiscali all'esame del Parlamento. Finisce il redditometro, ma non si ferma ovviamente la lotta agli evasori, che lo scorso anno ha consentito di recuperare 25 miliardi di evasione alle casse dello Stato. Ci saranno strumenti molto più sofisticati, molto più elaborati, ma meno invasivi del redditometro, che era uno strumento ormai obsoleto, grezzo, che creava solo creava solo confusione, senza in realtà stanare chi davvero non paga le tasse. Siamo, dunque, in presenza di un decreto e di modifiche accolte che segnano un cambio di paradigma, che ora prevede un approccio pienamente improntato al risultato e il monitoraggio dei risultati ora viene fatto a livello centrale. Si punta altresì allo sviluppo delle tecnologie critiche, cioè di quei settori che hanno investimenti con un alto moltiplicatore, tra i quali i semiconduttori avanzati, l'intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche e le biotecnologie. Ovviamente, per affrontare queste sfide viene previsto un ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa di tutti i livelli di governo territoriale, soprattutto nel Mezzogiorno. Altro punto importante è quello di prevedere elementi premiali per chi centra gli obiettivi e poteri sostitutivi per chi, invece, non riesce a fare bene. Inoltre, viene rivista la disciplina e il finanziamento del Fondo perequativo infrastrutturale; è anche revisione della *governance* istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo e la ricognizione dello stato di attuazione degli stessi. Le zone di semplificazione e i benefici fiscali previsti per la ZES unica vengono estesi anche alle zone logistiche semplificate. Viene incrementato il Fondo di sostegno ai Comuni marginali da destinare ai consorzi industriali; ci sono, inoltre, misure per i Comuni svantaggiati, che avranno le risorse per sostenere economicamente le piccole e microimprese. I Comuni avranno anche risorse per realizzare alcune infrastrutture ritenute prioritarie. Nel decreto-legge, inoltre, c'è ampio spazio a disposizioni che intendono affrontare il principale problema del Mezzogiorno, cioè l'incremento dei posti di lavoro, con misure che in parte hanno anche un respiro nazionale. Il testo reca misure in materia di ricerca e università, ma anche disposizioni in tema di istruzione rivolte a colmare i divari territoriali e infrastrutturali. Vi sono poi le disposizioni per favorire gli investimenti per la rigenerazione urbana il contrasto del disagio socioeconomico e abitativo; altre disposizioni riguardano il recupero dei siti industriali, soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno. L'approvazione del piano di azione per il Programma nazionale cultura è indirizzata in particolare al Sud come elemento per valorizzare un territorio certamente vocato al turismo. A specifiche operazioni del Programma sicurezza per la legalità 2021-2027 viene attribuita la qualifica di operazioni di importanza strategica. Da ultimo, vi sono misure per favorire gli investimenti del PNRR. La Commissione bilancio ha anche introdotto delle disposizioni, che noi consideriamo molto positive, per affrontare la cronica carenza di segretari comunali e provinciali, che sono figure fondamentali per il buon funzionamento della macchina amministrativa a livello locale. In questo senso c'è ancora tanto da fare, fintanto che non saranno coperti i fabbisogni; noi suggeriamo quindi di valutare di ricorrere ai segretari comunali in pensione che si rendano disponibili a mettere a disposizione della pubblica amministrazione la propria esperienza negli anni successivi all'entrata

rilanciavano l'economia del Paese rispetto alle politiche di *austerity* che ci stanno di nuovo strangolando e che caratterizzano questo avvio asfittico di legislatura dal punto di vista di economia e crescita,

la coesione e anche nelle politiche per le ZES; dall'altra parte, vediamo l'autonomia differenziata sfrenata a vantaggio delle Regioni, che poi però mi domando come potranno dare attuazione a tali misure se tutti i fondi che hanno a disposizione vengono scippati e portati all'interno di un Ministero che sembra avere una certa bulimia amministrativo-gestionale delle risorse.

coesione, adesso vediamo la cabina di regia centrale su questi fondi, la riforma delle zone economiche speciali, che da otto diventano una unica: prima ognuna aveva il suo commissario e la propria autonomia, mentre adesso c'è un'unica struttura centralizzata. Ci sembra, insomma, che abbiate qualche difficoltà a decidere in che direzione volete andare: se l'obiettivo è quello di ridurre le disparità territoriali, avere migliore competitività, un'autonomia delle filiere strategiche, non potete pensare che, andando da una parte o dall'altra, riuscite a raggiungere obiettivi che in parte sono divergenti tra di loro, perché le autonomie implicano un'assunzione di responsabilità e una delega a chi gerarchicamente si trova al di sotto del Governo. Se però volete puntare sul coordinamento e sull'efficientamento delle risorse, dovete necessariamente accentrare. Decidete cosa volete fare da grandi, se grandi volete diventare. Per adesso, sentiamo solo tanti annunci e nulla di concreto. Annunci, dichiarazioni roboanti, come: "stop ai *bonus* a pioggia", "basta, bisogna fare politiche strutturali ed incentivi stabili", "riformiamo tutto, lasciamo fare chi vuole fare"

Non so se vi rendete conto che la vostra parola d'ordine è l'incoerenza, ma anche all'interno dello stesso decreto. Prima,

e poi date un contentino approvando un emendamento, bellissimo tra l'altro, che prevedeva maggiore partecipazione delle autonomie locali, processi di transizione generale, interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato.

disoccupati di lunga data, di formazione e istruzione della popolazione adulta, perché, giustamente, le persone non sono qualificate e quindi avete previsto alcuni strumenti, cancellando

trovare strumenti di conciliazione. Infatti, mi aspettavo anche l'approvazione di qualche strumento di *smart working* per i genitori, per agevolare le famiglie di cui tanto vi riempite la bocca. Ebbene, tutte queste meraviglie cui stavamo plaudendo in Commissione, che quasi ci spingevano a valutare un'astensione su questo decreto, le avete stralciate nel maxiemendamento che ci avete portato in Aula. Anche quel poco di buono che fate, dunque, entra dalla porta ed esce dalla finestra. Siete meravigliosi: nella vostra totale incoerenza, siete meravigliosi. Ovviamente, tutto questo si accompagnava a un'infinità di proposte respinte, come la messa in sicurezza della rete viaria, la transizione digitale dei territori, la riqualificazione e l'efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche. Neanche questo avete approvato. Va bene, teniamoci le scuole fatiscenti che abbiamo, sempre perché questo è il Governo delle famiglie, del futuro del Paese. Niente parti sociali nella cabina di regia: siete particolarmente allergici a questi discorsi. Non avete neanche ripristinato la dotazione originaria del fondo perequativo per il Mezzogiorno. Quindi, le politiche di coesione le facciamo, ma con le briciole, e la sostanza, quella che abbiamo tolto, miliardi e mezzo, mica spiccioli. Dimenticate che esistono realtà marginali anche nelle aree interne e montane del Centro-Nord Italia, per cui vi avevamo proposto un fondo specifico di soli 600 milioni: anche quello rispedito al mittente. Avevamo chiesto che, per gli interventi previsti al Sud, fosse destinato un 40 per cento specifico anche da parte delle aziende partecipate pubbliche. Improvvisamente, abbiamo scoperto che una cosa che è stata fatta con buoni risultati nel 2019, nel 2024 non si può più fare. Non si capisce bene perché. Forse questo sarà un altro dei tanti buoni suggerimenti che vi diamo con i nostri emendamenti, che respingete, salvo poi poi ritrovarceli inseriti nei vostri testi governativi, come già capitato diverse volte. L'interesse per i cittadini italiani ci spinge a dirvi "bravi", quando quei pochi consigli buoni che siete capaci di capire li accogliete e li rendete realtà. Vi avevamo chiesto platee più vaste per i vostri *bonus*. Magari, se non li chiamate *bonus*, ci rendete anche un po' più difficile polemizzare nei vostri confronti e mettervi di fronte alle vostre incoerenze. Abbiamo scoperto che per ridurre la disoccupazione non possiamo trasformare i contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, perché lo scopo del *bonus* è quello di aumentare i posti di lavoro,

li licenzia e assume "a", "b" e "c" a tempo indeterminato con il *bonus* che gli state fornendo voi. Il risultato è che l'occupazione non cambia e avrete lasciato a casa tre persone formate e qualificate per assumerne tre senza nessuna formazione; ma è l'unico modo per l'azienda per mantenere i *bonus*.

i contratti a tempo indeterminato inferiori a venti ore settimanali, altrimenti stiamo parcellizzando il lavoro, non stiamo aumentando l'occupazione. *(Applausi)*. Stiamo creando lavoro di pessima qualità e lavoratori poveri, a cui non date State solo aumentando la povertà nel nostro Paese, come dichiarano tutti gli indicatori economici. Voi continuate a nascondere la testa sotto il tappeto. Non avete neanche consentito l'accesso

alla partecipazione all'aggiornamento professionale, diventa "accompagnata". Quindi i poveri, gli ex percettori di reddito, sono obbligati a fare corsi di formazione e aggiornamento professionale, mentre le partite IVA, che tanto vi stanno a cuore, vengono solo accompagnate; poi chi se ne importa se

mi sembra evidente e lampante che questo Governo agisce con profonda dicotomia tra una parte della maggioranza che tira verso la maggiore autonomia delle Regioni e l'altra parte che, invece, mira ad accentrare tutto nelle mani di pochi Ministeri che detengono il potere. Il risultato finale del tirare da una parte e tirare dall'altra, se non l'avete mai visto, è l'immagine delle torture medievali sui prigionieri incatenati con le mani di qua e i piedi di là e un rullo che tira e spacca in due la persona. Ecco, il risultato finale delle vostre operazioni può essere solo questo: spaccare in due il Paese. Non ve ne rendete conto e, se ve ne rendete conto, non ve ne importa assolutamente niente, ma solo questo è quello che potrete ottenere, con questo modo assurdo di procedere sulle spalle dei cittadini italiani. Ma perché non fate l'unica cosa sensata che potete fare per questo Paese? Se le Regioni non vi piacciono, non le ritenete adeguate a svolgere compiti così importanti, sopprimetele, cancellatele, siate coerenti con le vostre idee per una volta. *(Applausi)*. Noi comunque, in coerenza con le nostre idee, voteremo convintamente contro questo provvedimento.

in materia di politiche di coesione. Ringrazio la 5a Commissione e i relatori per il lavoro proficuo e ordinato che è stato svolto. Il provvedimento è volto a definire un quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare L'Italia è un Paese che offre innumerevoli possibilità di sviluppo: grande opportunità viene data proprio dalle caratteristiche morfologiche e climatiche. Il nostro Paese non è però riuscito a far fruttare le risorse che negli anni gli sono state assegnate. Sono forse

e resilienza e dal Fondo di coesione e iniziare ad avere una visione d'insieme. Troppo spesso abbiamo visto infrastrutture che possono essere definite cattedrali nel deserto, che magari vengono realizzate con le risorse che ci sono state assegnate, ma che poi non hanno una destinazione, restando inutilizzate. Questo, in un periodo in cui le risorse e i sacrifici degli italiani sono tanti, non deve più accadere.

coordinamento di raccordo tra lo Stato e le Regioni, proprio per non sprecare questa grande opportunità.

Devo dire che i Governi che ci hanno preceduto hanno pensato di risolverla con il cosiddetto *bonus* rubinetti. Noi, in questo momento, pensiamo che la soluzione sia ben altra. alle infrastrutture per il rischio idrogeologico, mi trovo d'accordo con la collega Paita. È vero, non si può pensare di realizzare le infrastrutture a valle, ma bisogna partire dalla montagna. dalla montagna. Visto che lei ha sottolineato che i senatori di centrodestra sono distratti dal telefono, bisogna informarla che in Commissione affari costituzionali si sta lavorando sul decreto montagna del ministro Calderoli, che va proprio nella direzione di mantenere vivi i territori di montagna. *(Applausi)*. È forse un po' distratta e magari non è a conoscenza di quello che succede nelle altre Commissioni.

È importante cercare di creare nuova imprenditorialità e dare supporto ai giovani perché restino nella loro terra e creino lavoro. Stiamo parlando di 3 miliardi di decontribuzioni che vanno proprio verso i giovani e le donne svantaggiate. Occorre creare soprattutto per i giovani, dando loro la possibilità di stare nella propria terra, avere una busta paga e una casa. Questa credo che sia una cosa di non poco conto.

Credo che in questo decreto coesione, che viene convertito oggi in legge, abbiamo trattato temi veramente importanti per riuscire a cercare di colmare quel *gap* che si è formato negli anni tra Nord e Sud e forse si è cercato, anche nella narrazione di questi giorni, da parte delle opposizioni, di nascondere l'ottimo lavoro che sta facendo il Governo, cercando di demonizzare l'autonomia. Ebbene, signori miei, ve lo dice una donna che viene da una terra autonoma: io sono orgogliosamente ladina, orgogliosamente trentina e quando mi confronto con voi, quando vi porto la mia realtà e vi racconto il mio territorio, vi sento dire: tu vivi in un altro Paese, tu sei fortunata.

tutte le Regioni italiane di crescere in base alla responsabilità, perché amministrare significa essere responsabili, significa avere piena conoscenza del territorio che si amministra, significa gestire le risorse portando i servizi migliori ai cittadini. Se voi siete contro questo concetto, significa che non avete fiducia nei vostri amministratori, perché chi si candida per amministrare, che sia un Paese o sia una Regione, deve prima di tutto essere responsabile e portare le risposte ai propri cittadini Del resto, la legge sull'autonomia parte proprio dalla riforma del Titolo V, che, come vogliamo ricordare, è stata approvata nel 2001 con il Governo Amato. Questa è una legge quadro che quindi disegna le regole, la cornice di regole per dare attuazione al principio dell'autonomia differenziata che si andrà a definire negli anni. Voi agitate uno spauracchio e dite che ogni Regione sarà diversa dall'altra;

e se le risorse saranno maggiori, lo Stato, visto che lo prevede per legge, dovrà automaticamente trasferire le risorse necessarie per garantire i LEP uguali a tutte le Regioni.

Mi viene in mente l'ex ministro Boccia, che nel 2019 - io ero già in Senato - era Ministro agli affari regionali e lui stesso diceva

sua reazione, quando è stata esposta una bandiera regionale. Vorrei ricordare al Ministro che noi tutti qui rappresentiamo una Regione, rappresentiamo

perché siamo in un Parlamento, vogliamo restare quelli che la gente ha votato. signora Presidente, annunciando il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier e vorrei concludere con una frase che fu di Alcide De Gasperi: «politica vuol dire realizzare». Ecco, il Governo sta facendo questo e noi siamo sulla strada giusta. Signora Presidente, colleghi e colleghe, il Gruppo Partito Democratico voterà contro la questione di fiducia, che a nostro avviso il ministro Ciriani e il Governo hanno posto in maniera frettolosa e non credo nobile per il ruolo che quest'Aula deve assumere sempre di più come luogo di indirizzo nella fase difficile di conversione di un decreto. Una fiducia che i numeri in Parlamento oggi certamente vi consentiranno di confermare. Una fiducia, signora Presidente, che tuttavia, se guardiamo in faccia il Paese reale, il Paese reale, si sta più velocemente del previsto affievolendo nel rapporto tra la vostra maggioranza, il vostro Governo e il Paese reale. Ve lo diciamo ora per allora: non pensate di interpretare la vostra sconfitta elettorale alle elezioni amministrative nelle più importanti città attribuendo la responsabilità alle regole elettorali. Peggio ancora quando chiamiamo in campo la partecipazione dei cittadini. Signora Presidente, lei sa bene quanto noi che, per recuperare partecipazione, è necessario valorizzare la credibilità delle istituzioni e il ruolo dei partiti. Non ci si arriva attraverso le modifiche delle leggi elettorali che servono ad una maggioranza *(Applausi)*; ci si arriva presentando proposte concrete, concrete, ci si arriva cominciando ad interpretare il ruolo nobile di queste istituzioni, non esautorando il ruolo del Parlamento o negando la funzione fondamentale della rappresentanza. La legge n. 81 del 1993 è una buona legge: ha garantito trent'anni di stabilità al sistema delle autonomie locali ed è anche riuscita a caratterizzare e a valorizzare il ruolo del sindaco nelle sue funzioni fondamentali, che l'elezione diretta peraltro gli ha attribuito. È una legge che ha attraversato tutte le maggioranze parlamentari e attribuire alle regole la responsabilità di un primo vostro logoramento evidente nel rapporto tra voi e il Paese è l'ennesima scorciatoia che attacca i principi basilari della nostra democrazia. Noi non ve lo consentiremo. Lo dico con altrettanta chiarezza: state operando ferite evidenti, con l'autonomia differenziata e con il premierato, che, insieme alla riforma della giustizia, a nostro avviso minano le necessarie cooperazioni istituzionali tra Stato, Regioni ed enti locali. Nel procedere in questo scontro - ecco perché vi chiediamo di riflettere attentamente - noi compromettiamo anche il principio fondamentale di sussidiarietà, necessario necessario e indispensabile per dare piena attuazione non solo alle politiche di coesione, ma anche alla più complessa, unica e straordinaria opportunità nelle nostre mani, quella della piena attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Fermatevi, perché non è con i conflitti tra le istituzioni che si può governare un grande Paese. Dovete fare un salto di qualità. Non basta più - lo dico, Presidente, anche interpretando le parole del ministro Fitto di ieri sera - la retorica del sempre opporsi al passato. Il passato verrà giudicato dagli storici; a questa maggioranza il Paese chiede di garantire un futuro, chiede di garantire una prospettiva, una visione. La nostra preoccupazione principale dentro questo decreto è stata esattamente questa: provare a far emergere e correggere le tante contraddizioni che in questo decreto sono purtroppo ancora contenute. Non riusciamo a capire come stia insieme una voglia evidente di abbreviare i tempi, di correggere i percorsi, di non interpretarli anche nel rapporto tra Stato, Regioni ed enti locali, esclusivamente richiamandosi all'efficienza e alla velocità, quando dovremmo avere ben in testa il principio di legalità e di cooperazione istituzionale. *(Applausi)*. tra l'altro, come si può spingere verso processi di centralizzazione che, nel decreto originale approvato dal Consiglio dei ministri, avevano addirittura trascurato il ruolo degli enti locali, delle Regioni delle Province e poi, dall'altra parte, venderci l'autonomia differenziata come una grande opportunità per il Paese. *(Applausi)*. Voi state lacerando le istituzioni, senza avere un'idea di come le istituzioni invece, per poter raggiungere obiettivi importanti, devono cooperare Signora Presidente, il PNRR discende da quella che considero la più importante operazione in sede europea che dopo la pandemia abbiamo costruito. Noi ci sentiamo parte di quel nuovo volto dell'Europa che, dopo una pandemia, decise non solo di affrontare insieme l'acquisto dei vaccini, interpretando bene il ruolo della scienza, della conoscenza, della competenza, ma soprattutto di spingere importanti investimenti, una parte di essi anche a debito comune. È la politica del Next generation EU, che ha dato all'Europa un nuovo volto che a noi piacerebbe riprendere. Il futuro di fronte a noi richiede infatti un'altra volta un investimento europeo per aggredire i temi delle transizioni e delle trasformazioni,

ha vissuto esperienze amministrative sa bene che molti dei dati che voi nelle conferenze stampa con grande abilità siete in grado di promuovere derivano da risorse che i Governi precedenti hanno stanziato. Per realizzare un investimento occorrono i tempi necessari per un percorso e un processo. L'occupazione e la crescita economica in questo Paese tiene grazie agli investimenti che i Governi precedenti avevano determinato. Anche sulle politiche di attuazione europea non è vero che tutto quello che è stato fatto in passato era un errore. Lo dico perché gli accordi con le Regioni che insistono sull'FSC sono accordi decisivi e voi avete completamente saltato il cuore e l'essenza delle politiche di coesione, che, per quello che ci riguarda, richiedono formazione delle risorse umane. Se andate a vedere l'origine e la radice fondamentale dei fondi di sviluppo e coesione, questi hanno nelle politiche della formazione delle risorse umane la loro centralità; altro che cabine di regia nazionali, che di fatto saltano o bypassano il ruolo delle Regioni. Voi vi state avvicinando, con questi provvedimenti, ad una definizione che rende sempre più bilaterale la negoziazione dei processi di attuazione. Se, come dice il ministro Fitto, tutto va bene, non vedo le ragioni per le quali riteniate inutile il ruolo del Parlamento. Dovete portare in Parlamento un monitoraggio dell'attuazione *ex post* ed *ex ante* del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono troppe le aree di ambiguità. La crescita economica, la buona e piena occupazione, la riduzione dei divari territoriali non si raggiungono con le conferenze stampa, né con le relazioni che portate in Parlamento; si raggiungono se diamo il via ai cantieri, se abbiamo un progetto di sviluppo economico e sociale che metta al centro la buona e piena occupazione. La stessa formazione è l'essenza delle politiche della coesione. Diciamoci la verità, o siete Mandrake oppure non si può saltare il più importante investimento per ridurre le disuguaglianze in un sistema territoriale, ossia l'investimento sulle risorse umane. I divari territoriali nascono proprio dalle differenze di capacità di reagire ai cambiamenti. Anche il tasso di occupazione femminile, oltre a politiche importanti per i servizi alla persona, oltre a politiche necessarie per la genitorialità, richiedono ovviamente di sapere che cosa formare e su che cosa formarci. Voi non avete un'idea dello sviluppo economico se le transizioni ambientali, sociali e digitali vi spaventano; sono un problema, anzi per voi sono il problema. Per questa Europa rischia di diventare un problema se non ci mettiamo la testa e non capiamo che le transizioni ambientali, digitali e sociali debbono rappresentare una straordinaria opportunità dentro la quale dobbiamo portare il lavoro, e dentro la quale, per portarci l'Italia, dobbiamo fare un investimento più grande possibile sulle risorse umane. Non si scappa. Abbiamo bisogno di più scuola, di più qualità formativa; abbiamo bisogno di superare il concetto che l'immigrazione è una clava per gestire il consenso. L'immigrazione, di fronte all'inverno demografico, è una necessità da gestire nella legalità, perché a noi mancheranno le risorse umane per aggredire le grandi trasformazioni che abbiamo di fronte, mancheranno le risorse umane per qualificare la nostra manifattura. Voi purtroppo confondete tutto questo con la propaganda, con la conferenza stampa, l'abilità che riconosciamo sul piano politico a voi ed anche al ministro Fitto di una retorica che ci racconta un progetto, che però è senza le radici per essere attuato, perché state scardinando la coesione territoriale del nostro Paese e la capacità di lavorare insieme nella legalità, in una cooperazione istituzionale che negate alle radici per ragioni di propaganda e di consenso. Non cercate scorciatoie, abbiamo bisogno di un nuovo volto dell'Europa e di interpretare gli enormi cambiamenti che abbiamo di fronte come un'opportunità e non come un problema. Certo, dobbiamo spingere verso la transizione ambientale, sociale e digitale il lavoro, ma dobbiamo avere ben presente che occorre guardare alla piena e buona occupazione. Dovete cambiare l'agenda delle riforme: portate in Parlamento quelle che servono al Paese, non quelle che servono a unire la maggioranza e spaccano l'Italia. *(Applausi)*. Questo è il passaggio più importante: abbiamo bisogno di affrontare il problema dei salari, della sanità, del lavoro, della buona e piena occupazione; abbiamo bisogno di un'idea dello sviluppo industriale, altrimenti non sapremo mai chi e cosa formare. Pertanto voteremo contro questo provvedimento e la vostra fiducia.

al contrario di quanto ho sentito finora dai banchi dell'opposizione, per quanto mi riguarda, danno orgoglio e nobilitano il nostro ruolo, perché

una quota importante di quello che può essere poi l'*input* in termini di coesione e di soluzione di tanto divario territoriale fra Nord e Sud, ma anche all'interno

ieri il ministro Fitto, e non è il quantitativo economico, che comunque è ingente e importante e può essere rivoluzionario per tante situazioni che stiamo affrontando tutti quanti insieme, ma è la qualità della spesa e l'attenzione che viene posta per migliorare la qualità della spesa di questo ingente stanziamento economico. Ad oggi, abbiamo davanti agli occhi come non funziona il modello di spesa: lo abbiamo visto tanto

tra Regioni più ricche e Regioni più povere e all'interno delle stesse Regioni, evitando sovrapposizioni di investimenti e coordinando fonti di finanziamento differenti, laddove probabilmente questi finanziamenti

tutto questo non è stato poi trasformato in qualcosa che diventa accentramento e delegittimazione del territorio delle Regioni,

lungo nelle traiettorie e negli obiettivi e soprattutto sterile per quanto riguarda la cantierabilità degli eventi. Il decreto-legge punta inoltre l'attenzione e accende i riflettori su temi importanti. Non è un generico strumento per manifestare intenti positivi di trasformazione e investimenti per il Paese, ma individua temi specifici, come il rischio idrogeologico, le risorse idriche, le infrastrutture, il ciclo dei rifiuti, la mobilità sostenibile e la transizione digitale. Pensiamo proprio alla dispersione idrica, di cui sentivo parlare

oggi non hanno più la stessa *performance* di quando sono state costruite, mentre l'acqua è certamente un elemento importante, che va salvaguardato. Questi sono gli interventi che a noi interessano, che portano coesione e che determinano un'eliminazione o comunque un abbattimento del divario tra le Regioni. Le politiche di coesione, infatti, servono proprio a questo: all'inclusione e alla legalità. Non voglio fare polemica, ma

Il nostro concetto di legalità, ci dispiace, ma è molto diverso da quello di una parte dell'opposizione e della stampa, che riesce ancora a giustificare chi occupa illegalmente

tra chi vive in Regioni più ricche e chi in Regioni più povere. Non accettiamo che gli onesti e le famiglie che rispettano le regole debbano fare la fila per aspettare che appartamenti vengano liberati dalla Salis e compagni. Questa per noi non è legalità. Mi viene da sorridere, se penso a come una parte dell'opposizione va ancora parlando di fascismo e antifascismo, di storia e di preistoria, e ancora non riesce a fare i conti con conquiste di civiltà ormai secolari come la proprietà privata. *(Applausi)*. Non riesco a capire come facciate a giustificare ancora questa parte di

il clima di armonia istituzionale utilizzato per affrontare i temi fosse quasi una *diminutio* nei confronti della minoranza. Invece voi dovete essere orgogliosi se nella Commissione bilancio si parla nel merito dei contenuti, si affrontano gli argomenti, si fanno emendamenti migliorando il decreto-legge e non si fanno folklore o ostruzionismo. Faccio quindi i complimenti a quella parte della minoranza

fare istituzioni e occuparsi della cosa pubblica: non fare ostruzione o folklore, ma riuscire a lavorare in maniera armoniosa e istituzionale, certamente nel rispetto delle prerogative di maggioranza e di minoranza e non lasciando vane le prospettive e quegli spazi a carico della minoranza.

non certo quella delle case o dei divani, ma intesa come lavoro per tanti nostri giovani, che vedono oggi delle prospettive anche nel Sud Italia,

investimenti importanti per quanto riguarda la formazione, la scuola e l'università e tre miliardi per quanto riguarda la rigenerazione urbana delle città medie e delle piccole città. investimenti che non si vedevano da tempo per quanto riguarda i sistemi informativi della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Così si combattono la mafia ed il terrorismo: investendo in tale direzione. Questa per noi è legalità: investire nella direzione giusta, spendere bene i soldi, programmare e avere una cabina di regia centrale, laddove le Regioni non dimostrano di essere all'altezza,

come cabina di regia e anche come soggetto giudice, laddove le Regioni dimostrano di non essere all'altezza del proprio compito. In conclusione,

che è sempre più centrale nelle dinamiche nazionali e internazionali, ha una centralità nello scacchiere europeo e internazionale e ha la capacità, attraverso

considerata sempre meno nello scacchiere e che, attraverso una stampa loro amica, provano a far passare messaggi sbagliati sul il nostro instancabile ministro Fitto e la nostra bionica Presidente del Consiglio, saremo costretti a deluderli ancora. dichiaro il voto favorevole della mia compagine, del mio partito e della mia famiglia di Fratelli d'Italia, augurando che anche voi possiate fare uno scatto d'orgoglio ed essere partecipi di una pagina importante della nostra Nazione.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

nominale con appello. Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi

Visto che la nazionale di calcio giocherà fra poco, l'estratto non poteva che essere il Speriamo sia di buon auspicio. Invito la senatrice Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Galliani.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 60. Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15, con la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024. La seduta è sospesa.

innanzitutto l'onorevole Presidente del Consiglio per la sua relazione: una relazione improntata a coerenza, a senso di responsabilità, a visione dell'interesse nazionale. Ringrazio anche il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, per il lavoro davvero immenso che ha svolto in questi mesi, insieme al sottosegretario Matilde Siracusano. Il Governo Meloni è l'unico, tra i Governi dei tre principali Paesi dell'Unione europea, a essere stato premiato alle elezioni europee, con un risultato storico. *(Applausi)*. Eppure, c'è chi pensa di avere il destino dell'Unione per sempre nelle proprie mani. C'è chi crede che la volontà popolare possa talvolta passare in secondo piano. questo atteggiamento da Gattopardo è un ostinato tentativo di non voler confrontarsi con la realtà. Siamo all'inizio di un nuovo capitolo nella storia dell'Unione e la nostra Nazione, Paese fondatore del grande sogno che è l'Europa, riprende il ruolo che le spetta, con dignità e a testa alta. Il prossimo Consiglio europeo rappresenta non una tappa, ma una nuova partenza per il rilancio politico dell'Unione. Esattamente oggi, settantanove anni fa, veniva approvato lo Statuto delle Nazioni Unite, per un ordine mondiale libero, fondato sullo Stato di diritto. Proprio nel solco di questa appartenenza, un'Unione sempre più integrata e organica con l'Alleanza atlantica è il fulcro essenziale di un'architettura di difesa e sicurezza comune in grado di garantire stabilità e di prevenire e affrontare le crisi globali in modo responsabile. Responsabilità significa anzitutto guardare in faccia la realtà di due guerre di aggressione che devastano l'una una Nazione dell'Europa, l'Ucraina, l'altra il Medio Oriente. La prima, la criminale guerra di Putin, è direttamente sostenuta sul piano militare, politico e della disinformazione da Cina e Corea del Nord, governate entrambi da sistemi comunisti, e dall'Iran, regime islamico e fondamentalista. La seconda guerra, quella in Medio Oriente, è la guerra di aggressione di Hamas, sostenuta e teleguidata da Teheran, contro l'esistenza stessa dello Stato e del popolo di Israele. La risoluzione di maggioranza, che oggi presentiamo, incoraggia il Governo a prendere ulteriori misure nei confronti degli aggressori. Ecco perché, oltre ad assicurare all'Ucraina il massimo sostegno per tutto il tempo necessario, la risoluzione invita il Governo a far sì che i responsabili di tutte le atrocità commesse contro il popolo ucraino - penso alla disumana deportazione di bambini ucraini per azzerarne l'identità stessa della Nazione Ucraina - siano perseguite come prevedono il diritto e la giustizia internazionale. Al tempo stesso, si devono condannare con la massima fermezza massacri, violenze e sequestri di ostaggi perpetrati da Hamas. La proposta di risoluzione di maggioranza chiede di sostenere gli sforzi per giungere a una soluzione basata sul principio dei due Stati che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza all'interno di confini sicuri e riconosciuti, così come prevede la risoluzione dell'ONU n. 2735. Anche il G7 si è concluso con posizioni nette, chiedendo esplicitamente all'Iran l'immediata interruzione della sua attività destabilizzante nella regione; il Corpo dei *pasdaran* esercita un potere dominante in quella regione ed è un'organizzazione terrorista già sanzionata da diversi Paesi. Le conclusioni del vertice G7 sono un importante dato politico per il nostro Paese, che deve essere motivo di orgoglio in quest'Aula. Al G7 sono state riconosciute priorità importanti per l'Italia, che rientrano pienamente in questo Consiglio europeo: penso al Piano Mattei e alle politiche migratorie. È in questi due casi che l'approccio italiano è diventato l'approccio europeo. Guardiamo ad esempio alle realizzazioni immediate e concrete del Piano Mattei, con la *partnership* per le infrastrutture globali e gli investimenti; la sinergia fra Italia e Stati Uniti in Kenya per sfruttare l'energia geotermica; la realizzazione del Corridoio di Lobito con il Global Gateway dell'Unione. Sono tutte realizzazioni menzionate e spiegate da Presidente del Consiglio nella sua relazione. Il G7, presieduto dall'Italia, ha riconosciuto e adottato nella sostanza politica le stesse linee sostenute dal Governo Meloni nella ridefinizione anche del patto su migrazione e asilo, recepite in cinque regolamenti europei (realizzazione riconosciuta di successo dalla maggioranza degli Stati membri dell'Unione), il protocollo con l'Albania, così come gli accordi UE-Egitto, UE-Tunisia. Altro punto della proposta di risoluzione di maggioranza è quello che il presidente Meloni, nel recente incontro con il primo ministro Orbán, ha definito come riunificazione piuttosto che allargamento. Si tratta dei Balcani occidentali. Circa l'adesione dell'Albania, da sempre l'Italia ne è grande sostenitrice, così come per tutti i Balcani occidentali. È un punto esistenziale per l'intera Unione quello della riunificazione. È pure di grande soddisfazione il progresso dei negoziati di adesione con Ucraina e Moldova; deve essere mantenuta un'altissima attenzione su quanto accade in Georgia. Infine, nella proposta di risoluzione di maggioranza evidenziamo l'Agenda strategica dell'Unione per lavorare per un'Europa competitiva e autonoma nei settori strategici, perché le attività industriali e produttive siano al centro. Vogliamo politiche *green* sostenibili sotto il profilo economico, sociale e politico, di competitività e di occupazione. Deve essere non una rivoluzione, ma una transizione. Ricordo che vi sono grandissime criticità nei rapporti con la Cina. Lo sottolinea il G7 in ben 28 diversi punti del comunicato. Le pratiche commerciali di Pechino stanno generando gigantesche distorsioni di mercato e dannose sovracapacità che minano industrie, lavoro, catene strategiche di approvvigionamento per l'Europa. Il prossimo Consiglio europeo è la nuova partenza per un'integrazione marcatamente politica. Spetta all'Italia un ruolo di primissimo piano nel tracciarne il percorso, sulla base di una interpretazione assai più mirata e selettiva dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità. È un successo italiano - e l'ha ricordato bene nella relazione anche l'onorevole Presidente del Consiglio - l'aver ottenuto che, nel preambolo dell'Agenda strategica, vengano richiamati questi due princìpi cardine dell'Unione, per un'Europa concentrata su grandi priorità come politica estera, difesa europea, politiche demografiche, piani industriali equilibrati in grado di conciliare stabilità, crescita e autonomia; un'Europa che non sottragga, per partito preso, spazi necessari di azione per le Nazioni che ne fanno parte. L'Italia al Consiglio europeo… questo carattere fondativo per l'intera Unione.

perché prima dei Consigli europei il Parlamento le affida la sua rappresentanza. Però è un'occasione diversa rispetto a quelle passate e questa rappresentanza assume una assume una forza differente, perché, oltre alla nostra rappresentanza e al nostro voto, lei ha appena ricevuto l'investitura e la rappresentanza più importante, quella diretta del popolo italiano per il tramite del voto. Come ha ricordato il presidente Terzi di Sant'Agata, lei ha l'onore di essere l'unico *leader* a cui il popolo ha tributato una crescita di consensi. Questo non può essere ignorato in sede di Unione europea, in qualsiasi tipo di discussione. Ma dirò di più, e questo purtroppo invece le renderà il compito più difficile: tutte le componenti del suo Governo hanno avuto una crescita di consensi. Questo significa che i cittadini apprezzano il suo, il nostro Governo e lo apprezzano nelle diversità, mettiamola così, e quindi lei ha il compito un po' difficile, mi rendo conto, di mediare queste diversità di fronte ai suoi interlocutori. Le rappresento, quindi, il punto di vista di una parte del suo Governo e poi ci affidiamo a lei, ovviamente, per la rappresentanza di tutte le parti, inclusa la nostra. iniziamo con la bassa cucina, con la questione un po' stucchevole delle nomine e delle poltrone che sta tenendo banco.

e le sfide enormi si superano solo con il consenso popolare. Sinceramente, non capisco questo sistema con un gruppo di potere vecchio, passato, che vede la sua base di consenso erodersi nelle urne, quale vasto consenso popolare possa rappresentare. *(Applausi)*. L'impressione che si ha dall'esterno è che si tratti di una conventicola di personaggi che rappresentano poco più che loro stessi. L'unica

Paese, è uno Stato che ha la popolazione della Provincia di Brescia, questo sempre per cercare di mettere le cose in proporzione. Altrimenti, la von der Leyen è all'opposizione anche a casa sua, Costa è all'opposizione anche in Portogallo, riesce a essere all'opposizione anche la signora Metsola a Malta, un interessante Paese che ben conosciamo e che tutti amiamo, anche quando magari non si comporta benissimo con i migranti, che fa 500.000 abitanti, in cui la signora Metsola è all'opposizione. Questi sono quelli che sono stati scelti per fare il salto, per riuscire a fare la grande crescita e a raccogliere il vasto consenso popolare che deve portarci verso una fase nuova, il tutto sotto la regia di un presidente Macron - non riuscirò mai a replicare la sua espressione quando l'ha salutato *(Applausi)*, ma diciamo che ero con lei in quel momento, il mio cuore era lì

a questa gente e noi la sosterremo in ogni caso, quindi scelga lei cosa fare, ma dal nostro punto di vista può tranquillamente dire no, ha la nostra benedizione, la supporteremo in pieno. Se posso dare un consiglio da amico, non cerchiamo le vicepresidenze, il commissario di peso, perché stiamo pensando di attaccarci a un qualcosa che io, da economista, vedo come il Titanic e oggettivamente avere il ruolo di primo ufficiale nel Titanic non è che porti a grandi risultati. Le spiego perché in questo caso parlo di Titanic:

si trova di fronte a un problema molto difficilmente risolvibile, perché stiamo parlando di uno Stato che non ha passato tutte le sofferenze (inutili dal mio punto di

Questa sofferenza inutile, che ha portato a disoccupazione, chiusure, recessione e danni, però ha sistemato la bilancia commerciale; cioè, col fatto che non spendiamo e continuiamo a non spendere, esportiamo più di quello che importiamo e quindi entrano soldi in cassa. La Francia, che non ne ha voluto sapere di fare niente di tutto ciò, secondo me abbastanza a ragione, è fortemente in *deficit* di bilancia commerciale, quindi è in *deficit* sia dal punto di vista del bilancio semplice, cioè spende più di quello che incassa, e importa più di quello che esporta. Questo doppio *deficit* non può andare avanti costantemente, a un certo punto il nodo viene al pettine e si può risolvere soltanto in tre modi. ne individuerà un quarto, ma io conosco solo tre modi con cui si esce da una situazione del genere. Il primo è con la svalutazione: se la Francia avesse il franco, svaluterebbe e a quel punto i suoi problemi si risolverebbero, ma non può perché ha l'euro, così come non poteva la Grecia, così come non potevamo noi quando a un certo punto in passato ci siamo trovati in una situazione analoga. Il secondo modo è fare austerità,

quindi una bella tassa sulle case o su qualsiasi altra cosa, in modo tale da togliere molti soldi ai cittadini francesi. Credo che questo non lo tollereranno, per quanto conosco come reagiscono i francesi non appena si tocca il loro portafoglio. L'ultima ipotesi che mi viene in mente è una forte crescita per via di investimenti degli altri Paesi intorno; cioè se noi crescessimo fortemente e se la Germania crescesse fortemente facendo grandi investimenti,

di tutte le regole non si fa con quelle persone, ma attraverso gente come lei, con persone che hanno già capito cosa non funziona e che sono appoggiate dai propri popoli, perché solo con il consenso popolare si fanno i grandi cambiamenti e le rivoluzioni. Lei ce l'ha, sia la rivoluzione di questa Unione europea. Signor Presidente, signora Presidente del Consiglio, membri del Governo, colleghi, letto l'intervento che oggi il Presidente del Consiglio ha depositato in quest'Aula dopo averlo enunciato alla Camera e personalmente lo condivido integralmente, non per appartenenza, ma per profonda convinzione dei contenuti sviluppati al suo interno; contenuti che, secondo me, meritano alcune riflessioni. Noi abbiamo appena assistito a una campagna elettorale per le elezioni europee in cui tutti i Paesi e la quasi totalità delle forze politiche, a prescindere dalla loro collocazione e dal Gruppo di appartenenza, di fatto non difendevano lo *status quo* dell'attuale Unione europea; tuttavia, dai primi segnali dopo le elezioni, quei cambiamenti annunciati, sperati e a parole voluti da tutti, sembrano non concretizzarsi, nonostante il chiaro segnale

appartenenti alle forze di maggioranza, ha avuto di fatto una promozione dai propri cittadini e dai propri elettori. *(Applausi)*. Ma il dato del cambiamento, secondo me, va visto anche rispetto

Nel 2022, dopo i vari allargamenti, i 27 Stati dell'Unione europea hanno il 16,7 per cento del PIL mondiale. In questo stesso lasso di tempo, la Cina passa dall'1,8 per cento di PIL mondiale del 1990 cento del 2022. Dunque, se da un lato è probabilmente ineluttabile, anche da un punto di vista demografico, che ci sia uno spostamento di ricchezza dal Nord-Ovest dal Nord-Ovest del mondo al Sud-Est, dall'altro è evidente che questo tipo di cambiamento può e deve essere rallentato. Esso può e deve essere rallentato attraverso politiche di difesa delle nostre produzioni e delle nostre imprese, che probabilmente l'Unione europea ha tradito. Quando ci riferiamo all'Unione europea lo facciamo con una notoria definizione: il gigante burocratico, il nano politico e il verme militare, che andrebbe secondo noi esattamente ribaltata. Questa è la prospettiva che tutta l'Unione europea si dovrebbe dare e che a parole, questa è la cosa che un pochino più perplime, in realtà ha tentato di fare almeno in campagna elettorale. In caso contrario, infatti, si rompe quella cinghia di tra elettori e rappresentanti, che è il *vulnus* vero della democrazia e la cifra stessa della democrazia.

è stata sempre quella di un'Europa che ci imponeva cosa mangiare, quale macchina guidare, come ristrutturare le nostre case. Al contrario, invece, sono stati lasciati troppo da soli i popoli europei che avrebbero voluto e hanno la volontà di svilupparsi diversamente, nella tendenza ad una omologazione complessiva che sicuramente va combattuta. Questo perché, non solo il motto dell'Unione europea è «uniti nelle diversità» (e troppo spesso questo motto fondativo viene tradito),

è stata un nano politico nelle politiche di approvvigionamento energetico: e si sa quanto lo abbiamo pagato rispetto alle situazioni internazionali che sono occorse negli ultimi anni. Europa dovrebbe occuparsi anche di politiche migratorie, di contrasto all'immigrazione clandestina. Qualcosa era già cambiato prima delle elezioni, con un cambio vero di paradigma per affermare un principio geografico geografico e non politico: che i confini dell'Italia sono anche i confini dell'Europa, che gli accordi presi con Tunisia, Egitto e in forma diversa con l'Albania vanno perpetuati in ogni luogo del Mediterraneo. Su questo, si sono sentite critiche veramente bizzarre. Sull'Albania, oggi seguiamo il Governo socialdemocratico tedesco, che vede quell'accordo come un esempio da seguire.

Penso ad alcuni provvedimenti, anche della giustizia amministrativa recente, come il caso delle motovedette, che l'Italia, in seguito ad

con la Tunisia, per ora c'è un provvedimento cautelare, ma l'11 luglio ci sarà la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, che invece mina questo accordo per presunte violazioni da parte della Tunisia. Poi ci sono tante altre cose su cui, secondo me, abbiamo il dovere di interrogarci. Io mi interrogo anche su un altro tema che non è stato affrontato nell'intervento del Presidente del Consiglio, che però mi lascia parecchio perplesso, anche rispetto a quello di cui l'Europa si deve occupare: mi riferisco alla procedura di infrazione avviata contro l'Italia sull'assegno unico. L'assegno unico è quell'elemento di importante socialità che è stato potenziato, nonostante la scarsità di risorse economiche, da questo Governo: 16 miliardi di euro quest'anno, tre miliardi in più, un aumento medio di 720 euro a famiglia, con un meccanismo premiale per le famiglie più fragili. Oggi quel tipo di provvedimento viene impugnato dall'Unione dall'Unione europea, perché secondo la *ratio* di qualche normativa europea, quel tipo di aiuto, quel tipo di provvedimento dovrebbe essere esteso anche a chi, per poche settimane, lavora in Italia e a quei figli che in Italia non sono e sono rimasti nei Paesi d'origine. Credo che su questo serva una vera e seria riflessione anche da parte del Governo italiano, perché cose di questo tipo devono poter essere decise sul piano nazionale. Quindi, signor Presidente del Consiglio, le auguro domani o dopodomani di rappresentare al meglio non il Governo, non la maggioranza, non Fratelli d'Italia, ma di rappresentare al meglio l'Italia, convinto che anche chi tenterà di criticarla nell'intervento di oggi sarà al meglio rappresentato da lei che difenderà gli interessi di tutta la Nazione.

che nelle prossime ore lei avrà la responsabilità di fare scelte di grande importanza, capaci di determinare il futuro del nostro Paese e dell'intera Unione europea. A lei il compito di percorrere la difficile strada che divide l'interesse nazionale, di cui lei ha sempre dichiarato di essere prima portabandiera, dalle tendenze disgregazioniste, e spesso schiettamente putiniane delle forze delle destre estreme, perché in questa circostanza il suo ruolo di Presidente del Consiglio italiano confligge con quello di capo dei conservatori europei. La notizia che il presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, Orbàn, non aderirà all'ECR è positiva, ma è motivo di preoccupazione il persistente e dichiarato allineamento, o una malcelata tolleranza delle forze di maggioranza italiane verso il Governo ungherese. I temi della politica estera, diritti civili, salvaguardia delle libertà fondamentali, divisione dei poteri non possono essere accantonati come questioni accessorie. Un eventuale appoggio, sia pure esterno, a una Commissione von der Leyen non può dunque essere a scartamento ridotto, mera merce di scambio. Le farò un esempio: la MOL è la compagnia petrolifera nazionale ungherese con reti di distribuzione

europea, a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina, ha deciso di rinunciare al petrolio russo, l'Ungheria ha imposto l'esenzione totale relativa alle forniture di petrolio che fluiscono attraverso gli oleodotti. Doveva essere un'esenzione temporanea, mentre rimarrà in vigore a tempo indefinito. MCC Bruxelles è il ramo europeo del *Mathias Corvinus* Collegium, il più grande istituto scolastico privato dell'Ungheria, con sede a Budapest. Il Parlamento magiaro gli ha conferito una partecipazione del 10 per cento nella MOL e nell'azienda farmaceutica Richter, per un valore complessivo di 1,3 miliardi di dollari. Queste risorse hanno finanziato iniziative intese a condizionare il voto europeo, mettendo in discussione il consenso delle politiche

per estendere l'oleodotto russo Druzhba dall'Ungheria alla Serbia, formando un progetto trilaterale che potrebbe andare avanti nei prossimi due anni. La nostra proposta di risoluzione impegna il Governo ad assumere una chiara e determinata posizione nei confronti delle azioni destabilizzanti nelle aree di interesse dell'Italia e dei Paesi europei, in particolare nell'area dei Balcani, per evitare che si rafforzi ulteriormente l'influenza della Russia. Al *premier* Orbán avremmo auspicato fosse stata rappresentata la riprovazione dell'Italia nei confronti di strategie come quelle che sta attuando il Governo ungherese e chiediamo che, se vi sarà a Bruxelles un commissario espresso dal suo Governo, sostenga questa posizione e lei faccia altrettanto nel Consiglio europeo, perché di tutto abbiamo bisogno meno che di essere sodali politici di un Orbán o di un Fico. La benzina e il diesel russi della MOL non conoscono confini, ma i controlli imposti ai valichi principali con la Repubblica di Slovenia creano grande disagio per chi giornalmente passa il confine e non fermano certamente i flussi migratori, che seguono strade poco battute. La sospensione di Schengen doveva doveva essere una misura temporanea, ma ormai nemmeno si fa cenno a quell'intento originario, cui pure avevamo dato un provvisorio e prudenziale consenso. Del lavoro di centinaia di poliziotti e militari dislocati sui confini si esaltano le manciate di profughi intercettati, ma nelle città gli atti di violenza si moltiplicano e il personale è carente. Anzi, come ha denunciato ieri il sindacato di Polizia, sono destinati a diminuire per i pensionamenti, nonostante le promesse del ministro Piantedosi. Comprendo la difficoltà nell'accettare questo fatto da parte di alcuni, spero pochi esponenti della maggioranza, ma il confine dello spazio Schengen non corre più tra Italia e Slovenia, entrata nello spazio Schengen nel 2007, ma molto più a sud, ai confini con la Repubblica di Croazia e gli altri Paesi dei Balcani. Diffondere e speculare sulla percezione dell'invasione e soprattutto il vostro adottare misure spettacolari, ma ahimè inutili contro migranti che arrivano lo stesso, male si declina con il plauso che riservate, a ragione, al grande progetto di Nova Gorica e Gorizia comune capitale europea della cultura per il 2025. Forse, improvvisamente, nel 2025 ogni problema sarà dichiarato risolto? O pensate di destabilizzare l'area rendendo vana questa collaborazione proficua e amichevole tra le genti e tra i due Paesi, che abbiamo costruito con fatica e convinzione? Non è tutto. Dalla prospettiva dell'estremo Nord-Est d'Italia, torniamo a lanciare un più forte allarme sulle conseguenze di quanto sta avvenendo nel Mar Rosso, divenuto area di crisi a causa degli attacchi alle navi, impossibilitate al passaggio del Canale di Suez. Gli impatti sul settore del trasporto marittimo sono pesantissimi, con la riduzione del 50

per mantenere i volumi dei traffici, incluse le infrastrutturazioni di porti ed energetiche. Aspettiamo invano si prenda in mano seriamente la questione del porto franco internazionale di Trieste, come ho recentemente fatto presente a un rappresentante del suo Governo, a cui lei è stata impegnata da un ordine del giorno proposto dal suo partito. Il mio emendamento *ad hoc* incomprensibilmente non è stato accolto. Presidente, si tratta di un interesse nazionale e non certo locale, che potrebbe rappresentare un grande volano di capitali globali e traffici. Opportunità da non lasciare all'iniziativa di certe potenze asiatiche e agli influssi della Russia. Le ricordo, signora Presidente, che sono gli influssi di queste potenze a rappresentare una minaccia agli equilibri dei Paesi balcanici e che il tanto auspicato allargamento dell'UE ai Balcani occidentali al momento resta soltanto un ottimo proposito. Ma, si sa, i buoni propositi lastricano la strada per l'inferno.

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, membri del Governo, colleghi, siamo qui, come sempre, prima di un Consiglio europeo che ha un ordine del giorno molto intenso, con problematiche importanti, per il futuro della nostra Unione. Come sempre e come tanti, sembrerebbe un Consiglio come quelli che si svolgono periodicamente, con i tanti temi che coinvolgono le nostre istituzioni: si parlerà di Ucraina, di Medio Oriente, di immigrazione (sempre grazie all'Italia) e di tanto altro. In realtà non sarà un Consiglio come tanti altri, perché di fatto in questo Consiglio si tratterà di quello che sarà la nostra Unione europea del futuro, quale sarà la sua caratteristica dei prossimi anni, perché siamo reduci da una elezione europea che sembrerebbe dare delle indicazioni molto chiare. Lo ha detto anche lei, presidente Meloni, oggi alla Camera e lo vediamo con i dati alla mano: tutte le forze di Governo dei Paesi europei, tranne l'Italia, perdono, ma soprattutto sono quelle stesse forze che hanno guidato le politiche europee degli ultimi anni. Al contrario, tutte le forze politiche che nel corso di questi anni, anche da punti di vista differenti, hanno sostenuto la necessità del cambiamento dell'Unione europea vincono, sono premiate dagli elettori e hanno la capacità di dire che bisogna intraprendere strade nuove per quello che riguarda il futuro della nostra Unione. da questi risultati ci aspettiamo un vero e proprio cambiamento di indirizzo politico e direi di indirizzo culturale. Ne abbiamo parlato tanto in campagna elettorale (in realtà anche prima), però proviamo a fare qualche esempio di come si dovrebbe provare a cambiare. La visione *green* è una grande sfida e una grande visione; la lotta ai cambiamenti climatici e la lotta all'inquinamento sono sfide a cui nessuno può sottrarsi in assoluto. Ma quando quella sfida diventa una testarda ideologia che punisce senza motivo imprese e cittadini, ecco che gli elettori ci danno un'indicazione chiara, e cioè che le proprie case non possono essere sottoposte a nuove spese; che le proprie case non possono essere sottoposte a nuove tasse, soprattutto per le persone meno abbienti e per quelle che vivono nelle aree interne e nelle aree più depresse della nostra Nazione. Non si capisce perché la sinistra italiana invece continua dritta e convinta su questa strada. Poi ascolti la Salis, ascolti Fratoianni e lo capisci. *(Applausi)*. Per loro, infatti, le case degli altri possono essere occupate e sicuramente non pagate.

C'è un altro tema esemplificativo anche su questo aspetto e lo citava prima il collega Barcaiuolo, perché poi le persone non capiscono, però votano.

aiutate, con 9,5 milioni di minori assistiti da questa misura. *(Applausi)*. È una bella cosa, vero? Uno pensa: che bella questa misura; non ci aspettiamo certo un applauso da Bruxelles, però magari ci aspettiamo di poter continuare le nostre politiche su questo settore. Invece arriva una letterina dalla Commissione che comunica addirittura un'infrazione all'Italia, perché questa misura dovrebbe essere estesa, secondo

questo tipo? Qui c'è gran parte del Governo presente e anche la Presidente del Consiglio. Non spetta a me decidere su questo tema, però se davvero non si riuscisse a far capire alla Commissione europea quanto è importante questa misura e le sue ragioni, sinceramente preferirei pagare la multa comminata dal vigile europeo, piuttosto che cambiare questa normativa, perché essa contiene il manifesto di un Governo che ha a cuore le proprie famiglie e i propri figli, e questo è molto più importante di qualunque fumosa normativa burocratica. burocratica. Aggiungo la visione del Mediterraneo, la visione del Sud d'Europa. L'Unione europea che verrà dovrà guardare al Sud, perché ce lo insegna banalmente la storia dei nostri secoli passati: non c'è Europa senza Mediterraneo e non c'è Europa che possa esistere se non guarda al Sud. l'Italia è stata ed è in prima fila ad aiutare ad Est l'Ucraina nella sua guerra di difesa contro l'aggressione russa e a chi parla di pace ancora una volta ribadiamo che per fare la pace basta

noi guardiamo a Sud e anche l'Unione europea dovrà guardare a Sud e alle politiche dell'immigrazione, anche grazie agli sforzi fatti dal Governo italiano in questi mesi e in questi anni, come gli accordi con la Tunisia e con l'Egitto e il Piano Mattei, che deve diventare davvero un piano europeo a tutti gli effetti. Il Consiglio di domani e di dopodomani dovrebbe semplicemente prevedere e dare la garanzia ai cittadini che c'è la necessità e il bisogno di un'altra Europa, un'Europa più concreta, meno ideologica, un'Europa che torni alle origini anche dei padri fondatori, che entusiasmava e che dava gioia e non faceva stare lontani dalle urne i cittadini perché non si capiva più che cosa fosse questa Europa. è, speriamo che nei giorni che vengono l'Europa sappia ascoltare le idee e le linee dell'unico Governo in Europa che cresce per consenso e fiducia: quello italiano.

Ho letto, naturalmente, il discorso che ha tenuto alla Camera e ci sono due questioni che, secondo me, restano fortemente aperte e che segnano una distinzione e una grande differenza tra le sue posizioni e le nostre. Lei ha spiegato che nel 1990, quando la Comunità europea era a 12, il nostro prodotto interno lordo era il 27,5 per cento della ricchezza mondiale, mentre nel 2022, con un'Unione a 27, siamo scesi al 16,5 per cento e ci ha spiegato che tutto questo è dovuto al fatto che l'Europa non funziona, perché c'è troppa Europa. in effetti precisamente il contrario: se noi siamo diventati meno competitivi nel mondo è perché c'è meno Europa, perché c'è un'Europa piccola, perché, per esempio, non esiste un mercato unico dei capitali. Faccio un esempio. Parliamo tanto di intelligenza artificiale, ma le nostre imprese, quelle europee, su quel settore così strategico non hanno fatto un passo e la ragione è una sola: un'impresa che voglia imbarcarsi in quel *business* ha bisogno di enormi capitali e finanziarsi su 27 mercati separati è di fatto impossibile. Un'impresa americana o un'impresa cinese hanno sicuramente una maggiore facilità di accedere ai ai capitali per poter crescere e fare ricerca e sviluppo di una impresa italiana o di un'impresa europea e dunque noi dobbiamo andare diretti verso una maggiore integrazione, verso una forma federale che abbia appunto un mercato unico dei capitali e che abbia anche un'unione bancaria.

dell'Europa, ma in questo momento lei è la grande assente dell'Europa, perché tutto sta passando sulla nostra testa. *(Applausi)*. La ragione è che l'Italia è isolata perché gli altri Governi non si fidano e fanno bene a non fidarsi, perché cos'è il Governo di Giorgia Meloni? È il Governo filo-ucraino, è il Governo atlantista o è il Governo che litiga al G7 per eliminare l'aborto dal documento e non parlare di diritti civili e litiga con Francia e Stati Uniti per questo? *(Commenti. L'Europa non è soltanto quella che misura la curvatura delle zucchine, come pensa la Presidente del Consiglio, perché altrimenti non si spiegherebbe perché tanti giovani in Georgia resistano alle cariche della polizia alzando il vessillo a 12 stelle dell'Unione europea. *(Applausi)*. Allora bisognerà capire lei chi è, signora Presidente del quella che sostiene l'Europa, l'Occidente, o se è quella che è amica di coloro che negano quello che l'Europa veramente è, altro che zucchine: l'Europa è diritti civili, libertà, separazione dei poteri, Stato di diritto, tutto quello che i Governi e i partiti con cui lei si accompagna non vogliono in Europa. Se l'Italia resta isolata e le decisioni passano sulla nostra testa, questo avrà un grande prezzo, signora Presidente del Consiglio, perché noi abbiamo da discutere, per esempio, del patto di stabilità, dei 22 miliardi che dovrete trovare per cominciare a scrivere la legge di bilancio. Ebbene, avremo grandi difficoltà con la Commissione europea, perché purtroppo noi in Europa siamo soli.

i quali intervengono in modo talora apparentemente delicato, talaltra apparentemente ruvido, marcando comunque contributi importanti, mi asterrò dal toccare qualsiasi tema economico. Nei quattro minuti che ho, toccherò un solo tema che mi sembra più importante dell'economia, persino in politica, e cioè la coerenza, per declinarlo sotto quattro frammenti che ritrovo nelle sue dichiarazioni alla Camera e quindi anche al Senato. Il primo riguarda la sussidiarietà.

e la devoluzione in questi casi, secondo me, è imperativa, obbligatoria. Ci sono esempi già da dieci o vent'anni di questo, per esempio, nella stessa politica della concorrenza. Tuttavia, nella variabilità della storia, vengono in emersione altre materie che diventano più importanti di prima e necessitano maggiore coordinamento di prima: penso alla politica estera, come lei spesso giustamente e con vigore sottolinea. Io ho già avuto occasione di chiederle, in una precedente seduta di questo consesso, quale fosse la sua visione sulla posizione del Governo tedesco di diffondere, creando un *club* degli amici della maggioranza qualificata in politica estera, il superamento un giorno del veto in politica estera. Lei ha dato una risposta articolata che io, come dissi, non condivido, esaltando quasi il dovere di riservare a tutti gli Stati membri, compresi quelli che verranno, gli stessi poteri di veto che abbiamo avuto storicamente tutti. Si dà il caso che il suo Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri abbia, invece, aderito a quella dichiarazione e io credo che siano comprensibili le difficoltà che lei ha. Arriviamo così alla coerenza che, in questa fase della sua

parole sante che condivido. Tenga presente, signora Presidente del Consiglio, che quasi sempre sono gli Stati membri che aggiungono di loro (si chiama *gold plating)* ulteriori elementi di freno e di specificazione minuta alle direttive che la Commissione propone, sotto influenza, come sono gli Stati membri (è un fatto della vita), delle *lobby* dei vari settori industriali eccetera. Agisca quindi il mondo dell'industria europeo e agiscano i Governi europei contro sé stessi prima di di lagnarsi che la Commissione europea produce cose troppo burocratiche. Terzo punto, io auguro di cuore, a lei e al nostro Paese, di avere un grande successo nelle nomine che arrivano. le auguro anche di non dovere, per sottolineare quello che sarà di sicuro un successo, minimizzare ciò che è avvenuto prima di lei. In fondo, sia sotto Governi di sinistra sia sotto Governi di destra, l'Italia ha avuto spesso personalità di peso, come oggi si usa dire, nella Commissione. Ricordo il presidente della Commissione Romano Prodi, ricordo l'alta rappresentante per la politica estera Mogherini durante il Governo Renzi, ricordo il vice presidente Tajani, commissario durante il Governo Berlusconi. Ricordo, se posso, me stesso, commissario al mercato unico sotto il Governo Berlusconi e alla concorrenza sotto il Governo D'Alema.

La gravissima crisi della Francia può farci piacere, in una certa prospettiva, ma è un gravissimo problema per l'Europa e per la sua integrazione. Questo lo sappiamo. proprio ora che lei è calda di riflessioni sul premierato, non tenesse in conto che la ragione di base di questa dilaniante crisi francese è che quello è l'unico Stato europeo dove il capo del potere esecutivo è eletto direttamente dal popolo. *(Applausi)*. Per governare, ha dovuto dilaniare il suo popolo. si dice, ma io oso sperare che non sia vero, che magari ricorreranno ad un governicchio tecnico: quelle cose che ogni tanto succedono. Io oso sperare di no.

Signor Presidente, offrire un sincero sostegno alla presidente Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo oggi è più che un semplice passaggio formale. Sarebbe un errore trascurare la grande importanza di questo incontro. Le scelte che verranno prese domani e nelle prossime settimane non solo definiranno la linea politica della Commissione europea per i prossimi cinque anni, ma saranno cruciali per garantire all'Italia il ruolo che merita all'interno dell'Unione. Non a caso la presidente Meloni ha parlato di Italia e non di Governo italiano, nonostante quest'ultimo abbia ricevuto un mandato forte dalle elezioni. La partita che si gioca a Bruxelles riguarda il nostro Paese, non una singola fazione politica, non il centrodestra, non la sinistra. Sfortunatamente, la sinistra sembra quasi compiacersi e persino trovare un certo masochismo all'idea che il Governo possa essere escluso dai tavoli decisionali sulla *governance* europea. In momenti come questi dovremmo tutti essere dalla stessa parte, indossare insieme la maglia della nazionale, tifare per il bene dell'Italia, sostenere il Governo, qualunque sia il suo colore politico, perché i risultati saranno nell'interesse di tutti: famiglie, cittadini, imprese e lavoratori. L'opposizione non riesce a comprenderlo, preferendo piuttosto giocare e sabotare: come se fare del male danneggiasse il Governo e non l'intero Paese. Questo significa essere contro gli interessi italiani, tradire gli interessi della Nazione e anteporre il proprio tornaconto politico al bene dell'Italia. Il voto delle elezioni europee ha parlato chiaro in tutta Europa. La stragrande maggioranza dei cittadini europei ha chiesto un cambiamento. I socialisti e i verdi perdono le elezioni. Francia e Germania ne escono ridimensionate pesantemente ma, malgrado questo, pretendono di continuare a dare le carte, di fare e di disfare. Noi, come forza principale del PPE, abbiamo sostenuto lealmente la passata Commissione e abbiamo contribuito a farla nascere, ma alcune scelte sono state totalmente miopi nei confronti dei cittadini, con le politiche dissennate dell'ultra ecologista Timmermans. Questo è il capitolo che dobbiamo chiudere. Questo è il motivo perché è necessario quel cambio di passo. La Commissione deve avere la solidità e la determinazione per cancellare i danni provocati dalla follia delle case *green*, perché parliamo di persone, di famiglie

modo, è urgente e necessario fermare quella direttiva che blocca le auto a benzina e diesel, perché rappresenta un colpo mortale per le molte aziende automobilistiche che saranno costrette a convertire la loro produzione a costi elevatissimi, con il concreto pericolo che molte di esse esse falliscano e, di conseguenza, mandino a casa milioni di lavoratori. Sono o non sono ragioni sufficienti per avere una Commissione forte? Sono o non sono ragioni sufficienti perché l'Italia abbia un ruolo di primo piano nella Commissione e prima ancora al tavolo delle trattative, con la garanzia del rispetto che merita il nostro Paese, uno dei pochi uscito dalle elezioni più solido e credibile di prima? Secondo noi sì. sì. È per questo che le chiediamo, signora Presidente, di continuare a lottare con l'energia che le riconosciamo ogni giorno, di andare domani a Bruxelles, perché intorno a quei tavoli stanno facendo i conti senza l'oste, senza l'Italia, e ricordare loro che senza l'Italia non si va da nessuna parte. Quello che sta accadendo a Bruxelles in questi giorni mette in luce i limiti di una costruzione europea, spesso caratterizzata da una mancanza di democrazia nel processo decisionale. Che senso ha infatti, dopo le elezioni per il Parlamento europeo, elezioni che arrivano dopo un periodo di guerra e di pandemia, riproporre lo schema che ha portato a quella che è forse la più concreta umiliazione del progetto europeo? Le elezioni europee non formano un Governo, come avviene a livello nazionale, poiché i Governi democraticamente eletti trovano il loro spazio e il ruolo nel Consiglio europeo. La Commissione europea ha una funzione diversa: essa esprime e afferma quella logica comunitaria che sostiene e dà significato al processo di integrazione dei popoli europei. Per questo motivo l'esclusione politica di una parte significativa dell'elettorato europeo rappresenta un vero smacco alla costruzione comunitaria. L'Europa deve tener conto della volontà popolare, altrimenti apparirà come una fortezza di privilegi e di interessi elitari, incapace di difendere le aspirazioni dei popoli. Allo stesso tempo va detto che l'Italia, grazie soprattutto alla volontà politica di Silvio Berlusconi, è stata in grado di favorire un'integrazione tra popolari e conservatori nell'interesse della Nazione e sarebbe opportuno che in sede europea il rapporto tra popolari e conservatori maturasse al punto da poter influenzare l'agenda della nuova Europa che i cittadini hanno espresso con il loro voto. Quindi che fare? Sappiamo bene che la Commissione europea ha bisogno di numeri in Parlamento e siamo anche realisti. Come detto, auspichiamo l'unione di centrodestra di Governo, ma, se così non fosse possibile, mi sento di dare un consiglio non richiesto, avendo avuto il privilegio di sedere su quei banchi: attenzione a coloro che invitano ad andare avanti senza tener conto dell'espressione dei cittadini, perché in Parlamento, quando ci sarà bisogno dei voti, non ci saranno i burocrati europei, ma parlamentari eletti dal popolo che al popolo rispondono e spesso si muovono con logiche difficili da incardinare nei classici schemi di partito. Già nel 2019, in una diversa epoca mancarono molti voti, pur disponendo di una sponsorizzazione politica più solida di quella di oggi. Non aprire a forze che rappresentano milioni di cittadini per una chiusura mentale e ideologica e per ascoltare forze di sinistra è un rischio. Bene ha fatto il ministro Tajani a sottolineare come l'eventuale apertura ai Verdi metterebbe a repentaglio il nostro voto e non solo. In conclusione, ci auguriamo ancora una volta che l'Italia possa ottenere il ruolo che gli spetta di diritto: lo dobbiamo alla storia dell'Italia, Paese fondatore dell'Unione europea, che può garantire la piena realizzazione delle intuizioni di Adenauer, di Schuman e di De Gasperi, nel progetto politico chiamato Europa unita. Buon lavoro, Presidente.

facciamo il tifo per lei e soprattutto per l'Italia. Speriamo però che la sua presenza in Europa non sia come le ultime presenze, perché fino ad oggi ha fatto semplicemente la comparsa, senza aver portato nessun euro in più all'Italia e agli italiani e senza alcun risultato. Nella sua relazione lei auspica una serie di situazioni a favore dell'Italia e a favore dell'Europa: auspica la necessità di cambiamenti nelle politiche europee; auspica la modifica dello *status quo* delle regole europee; auspica la pace (anche se poi concorre nell'inviare sempre più armi e sempre più sofisticate); auspica una maggiore crescita, ma dimentica, presidente Meloni, che la crescita in Italia è ferma allo zero virgola, con una produzione industriale ferma da oltre quindici e dimentica anche, presidente Meloni, di aver accettato le politiche europee ispirate all'*austerity*, fatte di tagli e di tasse; auspica una deregolamentazione a livello europeo, però attenzione, presidente Meloni: le regole europee servono per indirizzare l'innovazione, la competitività e la produttività. Spesso accade come nell'ultima sentenza della Corte di giustizia, in cui è la giustizia che deve intervenire per modificare le distorsioni dei Governi, e come nel caso Ilva, in cui ancora vi accanite senza tener conto delle tante sentenze. Proprio ieri la sentenza della Corte di giustizia su Ilva ha tolto tutte le ambiguità tra le produzioni industriali inquinanti e il diritto alla salute. Lei ha auspicato anche maggiori risorse per gli investimenti, dimenticando però, forse, che lei stessa quegli investimenti in Italia li ha completamente bloccati,

presidente Meloni, è aumentata del 5 per cento. Avete solo favorito gli evasori con 19 condoni. Altro che «lasciamo in pace chi vuole fare»; voi avete lasciato in pace chi evade le tasse.

E qui noi vi sottolineiamo che la storia si ripete. Chissà perché, ogniqualvolta che le destre vanno al Governo (2005, 2009, 2022), l'Italia entra in una procedura di infrazione. Era già accaduto nel 2009 con il Governo Berlusconi, che voi dimenticate. Sì, presidente Meloni, lei sta ridendo, ma è così; adesso glielo ricordo. Il Governo Berlusconi entrò in una procedura di infrazione, nel 2009, per un *deficit* eccessivo

sarà ricordata per il *record* del debito pubblico e avrà una medaglia per questo, cara presidente Meloni.

Noi ancora non sappiamo qual è la posizione del Governo italiano. Abbiamo perso già la sovranità monetaria e abbiamo perso la sovranità bancaria. Il tema della sovranità bancaria è ancora incompleto perché mancano le tutele dei risparmiatori sui depositi, in caso di crisi bancaria. Oggi si parla del mercato unico dei capitali per andare a mettere le mani negli oltre 30.000 miliardi di risparmio privato, prevalentemente quello italiano. Non sappiamo dove questa *governance* che si vorrebbe istituire andrà a indirizzare questi capitali, quindi vi chiediamo di prestare attenzione su questo. Attenzione anche al rischio delle diseguaglianze, perché nel momento in cui i capitali seguono la maggiore redditività, andremo ad accentuare il rischio delle diseguaglianze, quindi attenzione a queste due problematiche. Con riferimento alla competitività economica, invece di puntare su una maggiore integrazione dei capitali, vi chiediamo di puntare molto sul debito pubblico europeo comune, quello che noi abbiamo portato in Europa e grazie al quale abbiamo finanziato il PNRR. *(Applausi)*. Inoltre, presidente Meloni, noi chiediamo una maggiore integrazione economica e fiscale, facendo una una lotta al *dumping* fiscale che danneggia le nostre aziende (quindi per un fisco più equo), ad un *dumping* salariale per la lotta alle diseguaglianze. Soprattutto chiediamo una unificazione fiscale, una tassa unica europea su grandi capitali e un nuovo *welfare.* Presidente Meloni, nella sua relazione lei non cita mai le grandi emergenze del Paese, come quella delle diseguaglianze, della povertà, dei salari fermi, di riscrivere il *welfare* in Italia e della sanità pubblica. In ultimo, vorrei dedicare dello spazio al tema della guerra in Ucraina. Oltre 100 miliardi spesi come sostegno finanziario, 35 miliardi in spese militari. Meloni, il veto sulle armi inviate e sulle spese sostenute e dica agli italiani che già oggi avete anche sottoscritto la partecipazione al Fondo europeo per la pace; altro che per la pace: state finanziando esclusivamente le armi e le spese per le attrezzature militari con quel fondo. L'Italia è impegnata a raggiungere 2,1 miliardi di spesa. Scommettete sulla pace e non sulla vittoria sul campo di guerra, che non avverrà

Non è servito a nulla. Le banche russe concorrono con le banche europee a *record* mai raggiunti: 37 miliardi nel 2023. Un'economia, quella russa, in crescita perché si è trasformata in un'economia di guerra. Poi l'assurdità: le banche europee continuano ad operare in Russia. Un'inchiesta del «Financial Times» ha svelato che le banche europee, anche quelle italiane, hanno realizzato extraprofitti ed hanno pagato tasse in Russia per circa 800 milioni di euro. Gli extraprofitti di cui noi chiediamo una tassazione a livello europeo ancora non sono tassati. tassati. Vi rammento che questo conflitto ha realizzato un asse forte Russia-Cina; la bilancia commerciale della Russia è ormai orientata più verso la Cina: oltre 200 miliardi di

Sulla guerra in Medio Oriente prendiamo una posizione chiara a livello europeo per dire basta al genocidio che la popolazione palestinese sta subendo dopo l'orribile attacco di Hamas. lei domani andrà in Europa e noi facciamo il tifo per lei. Speriamo che torni con le soluzioni a tutte le emergenze del Paese e soprattutto con le risorse necessarie. In caso contrario, presidente Meloni, se non troverà

il tempo delle mele è terminato: non vogliamo trovarci con quello delle spine. *(Applausi)*.

nel prossimo Consiglio europeo ci diranno quale direzione l'Europa vorrà seguire e il ruolo che vorrà riconoscere all'Italia, anche alla luce dei recenti risultati elettorali. Le notizie che arrivano non sembrano indicare un cambio di rotta, come abbiamo auspicato, e sembra invece che vogliano servirci la solita minestra riscaldata, tra l'altro neanche arricchita di nuovi ingredienti. Il dato dell'astensione, che supera quello dei votanti, impone un cambio di passo; non tenere in considerazione il risultato elettorale sommato al dato dell'astensione, proponendo vecchi schemi, vecchi accordicchi e vecchi nomi, vuol dire non aver capito nulla e che tuttora prevalgono egoismi a discapito del bene comune e, in questo caso, dell'interesse dei cittadini europei. In uno scenario geopolitico in continua evoluzione, abbiamo la necessità di un'Europa stabile e coesa, mentre sembra che si stia scegliendo di andare in tutt'altra direzione, ovvero in quella dei compromessi al ribasso. Gli avvenimenti attorno a noi non sono tranquillizzanti: la guerra in Ucraina, quella in Palestina, la situazione del Mar Rosso con gli attacchi degli Houthi alle navi in transito, attacchi limitati grazie alla missione Aspides che vede l'Italia al comando delle Forze in mare e mi lasci ringraziare per suo tramite, signor Presidente, gli uomini e le donne imbarcati sulla nave Duilio, che sono impiegati nella missione nel Mar Rosso a garanzia della libertà di navigazione. A parte gli scenari più noti, abbiamo una serie di riposizionamenti e nuovi contatti che dovrebbero farci riflettere e che dovrebbero far riflettere l'Europa e chi oggi imposta le basi per il suo futuro. L'attacco di Hamas a Israele è avvenuto mentre si stavano perfezionando gli Accordi di Abramo e quindi l'auspicata normalizzazione delle relazioni tra Arabia Saudita e Israele e l'attacco è avvenuto, guarda caso, il mese successivo rispetto alla firma dell'Accordo della via del Cotone, il corridoio India-Medio Oriente-Europa, che poteva essere concorrenziale alla Via della seta. Oggi abbiamo nuovamente la tensione tra Israele ed Hezbollah, che potrebbe aprire un nuovo fronte dopo Gaza. In Niger abbiamo in fase di ritiro un migliaio di militari statunitensi, la Francia ha già lasciato in buona parte il Sahel. In sostituzione, le giunte militari che hanno preso il potere in Mali, Niger e Burkina Faso stanno aprendo le porte a russi, cinesi e turchi. Il Niger sembra interessato ad avere una vera e propria base militare delle forze armate russe, il Burkina Faso sta facendo carico di veicoli blindati, armi, mezzi e camion provenienti dalla Cina. Ricordiamo che il Burkina Faso nel 2023 è stato il Paese più colpito al mondo dai terroristi. A tutto questo aggiungiamo che qualche giorno fa due navi da guerra russe sono arrivate nel porto di Tobruk, in Libia, ambito dalla Marina russa, che lo vorrebbe come seconda base navale nel Mediterraneo, dopo quello in Siria. quindi possibili scenari futuri legati all'approvvigionamento di materie prime, emigrazioni di massa e terrorismo, che possono diventare un potenziale pericolo, in modo particolare per l'Italia e per l'Europa. Da non sottovalutare sono anche il cambio di vertice NATO e la scadenza elettorale americana di novembre. Siamo, in sostanza, in un periodo molto delicato e di massima vulnerabilità, in cui l'Europa si deve dare un'identità e una postura nuove, per rispondere principalmente al mandato ricevuto dagli elettori, che come risposta non vogliono un'Europa in cui pochi intimi decidono per tutti gli altri e più che mai c'è bisogno di un'Europa forte. Occorre un'Europa in cui si inizi realmente a parlare di politica estera comune prima che di difesa comune, passando da decisioni collettive e non da balzi in avanti elettorali, come abbiamo visto fare di recente a Macron, perché ogni dichiarazione scomposta di chi rappresenta uno Stato membro mette in pericolo tutti gli Stati membri. L'Europa non può trovarsi nuovamente esposta per non aver attuato le misure in cui tutti i Paesi europei sono parte attiva e non semplici comparse. Se l'approccio è quello che abbiamo visto in questi giorni, non è escludendo l'Italia dalle scelte sul futuro dell'Europa che l'Europa verrà rafforzata. L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione europea, siamo la seconda manifattura del continente, il terzo per popolazione, e abbiamo un Governo nuovamente legittimato dal risultato elettorale, contrariamente agli altri Paesi europei;

Rivendicare ciò che siamo e ciò che ci spetta è il mandato che ci hanno nuovamente consegnato gli elettori. Nel rivendicare questo, signora presidente del Consiglio Meloni, troverà la Lega sempre al suo fianco.

non dopo aver fatto rilevare a tutta l'Assemblea che siamo in presenza di terribili reati, ma un conto è il reato tale è - di immigrazione clandestina, che si basa sulla disperazione, e un conto è il reato di sfruttamento e caporalato, che si basa su ingordigia e avidità. Non sono la stessa cosa e noi come italiani, dobbiamo farci carico, dell'aberrazione di ciò che succede quotidianamente. Il Consiglio europeo sarà decisivo. Consiglio, le sue parole possono essere riassunte così: più Europa. Se ci muoviamo in un mondo di carnivori, non c'è più spazio per gli erbivori e noi siamo tali. C'è la necessità di più Europa;

siamo irrilevanti, se procediamo in ordine sparso. Non solo noi, anche la Francia e la Germania, che è il Paese più importante d'Europa. La globalizzazione ci chiama a delle sfide. Guardate cosa sta capitando nel Mediterraneo: rischiamo di essere spettatori nel mare nostro, perché la potenza neo-ottomana e la Russia rischiano di dare le carte, anche per quanto riguarda aree di influenza e di esplorazione assolutamente fuori dalle aree di loro pertinenza, che però sono rivendicate. Dunque abbiamo bisogno di un'Europa, ma così com'è non ci soddisfa. Io non ho visto qualcuno in campagna elettorale che abbia detto che l'Europa ci soddisfa: tutti hanno detto che non ci soddisfa; tutti hanno detto che c'è troppa burocrazia in Europa; tutti hanno detto altre cose, che sono state riprese in questa sede. Penso alle obbligazioni europee per gli investimenti: è un'ottima idea. Chiediamo alla Banca europea degli investimenti un impegno in materia di difesa; chiediamo una condivisione rispetto alle questioni di immigrazione per Paesi come il nostro, che sono di primo approdo; chiediamo, ad esempio, che su tante materie ci sia una responsabilità europea, proprio per questo si parla di difesa comune.

europea, rispetto a questi indispensabili teoremi che lei ha riproposto il Parlamento, sono proprio quelle forze sovraniste che si rifanno a un nazionalismo che non vuole comunitarizzare alcuna competenza con l'Europa. *(Applausi)*.

Draghi - che noi, nella filiera dei partiti sovranisti, troviamo anche tutti gli amici di Putin. Se pensiamo a chi, a livello europeo, sta sta operando per evitare, magari mettendo dei veti, che l'Europa si muova in una direzione di solidarietà reale all'Ucraina, questi non sono né i socialisti né i popolari: sono i sovranisti europei.

a livello europeo, che si ripropone con la von der Leyen Presidente. È la fotografia della realtà, non è polemica. È dire che la situazione europea è complessa e non si può tagliare con l'accetta, perché le contraddizioni sono ovunque. Meloni a testa in giù? No, assolutamente. Chi la vuole a testa in giù? Noi la vogliamo a testa alta. Noi vogliamo che l'Italia pesi al prossimo vertice

senza confondere gli interessi che rappresenta statutariamente, come Presidente del Consiglio, con gli interessi del Gruppo politico dei sovranisti, che peraltro è diviso in tre o quattro gruppi a livello europeo. L'Italia ha diritto a rivendicare le posizioni che le spettano e non può fare la passacarte a livello europeo. Io, ad esempio, auspico che ci sia un commissario di peso e questo lo riterrò

il presidente Gentiloni, che ha fatto un buon lavoro a livello europeo nell'interesse dell'Europa, certamente non confliggendo con il nostro interesse

l'Italia, è importante averle e questo è assolutamente necessario. Ultime due osservazioni. Sull'Ucraina, signor Presidente, nessuna pace può coincidere con la sottomissione dell'Ucraina. Questa è una grandissima contraddizione e chi la avanza si assume responsabilità altissime. Noi dobbiamo continuare sulla linea del Governo Draghi e del Governo Meloni, minimo comun denominatore di valori condivisi. Non possiamo stare dalla parte di chi dice: né, né. E neanche possiamo salvarci la coscienza chiedendo pace e basta, perché la pace non si costruisce sulla

Io dico da sempre "due popoli, due Stati". La DC, nella Prima Repubblica, diceva "due popoli, due Stati". Il PCI diceva "due popoli, due Stati". Tutti dicevamo "due popoli, due Stati", poi però, se vogliamo essere coerenti, quando ci sono migliaia di insediamenti illegali, non possiamo far finta di girarci dall'altra parte e non dire una parola al Governo Netanyahu che continua nella politica degli insediamenti. aderendo e dimostrando piena solidarietà a Israele, non possiamo non pensare che ci sono più di 34.000 morti dalla parte dei palestinesi. Capisco le cautele del ministro Tajani, le capisco, ma penso che dovremmo anche incominciare ad avere un po' più coraggio per quanto riguarda il riconoscimento dello Stato palestinese, perché questo non contraddice affatto i nostri sentimenti di solidarietà verso Israele. Israele è una cosa, il Governo Netanyahu è un'altra. *(Applausi)*.Possiamo benissimo dire che Israele è nel codice genetico delle nostre amicizie, ma il Governo Netanyahu da noi è considerato nefasto per gli interessi di quello Stato.

Presidente, onorevoli colleghi, il Consiglio europeo sarà fondamentale per definire il corso che l'Unione europea seguirà nel prossimo futuro. Si parla tanto di nomi e di nomine, come ha fatto poc'anzi il senatore Casini, su chi andrà a occupare le caselle e i vertici delle istituzioni europee, ma francamente all'Italia interessa poco un dibattito che non sia incentrato su ciò che l'Unione europea vorrà essere nei prossimi anni e su ciò che vorrà costruire. A noi - l'abbiamo sempre detto - non piace un'Europa che si occupa di troppo, ma non di ciò che è davvero importante, che si sostituisce agli Stati e si intromette nei loro affari interni. Noi crediamo in un'Europa che affermi gli interessi comuni dei popoli europei, capace di avere un peso a livello globale ed in grado di prendere decisioni forti e coraggiose di fronte a crisi internazionali che minacciano la sicurezza e la stabilità del nostro continente. Ecco perché, ad esempio, il sostegno convinto all'Ucraina contro l'invasione russa deve restare un punto fermo nell'agenda europea e il Governo italiano guidato da Giorgia Meloni continuerà a fare orgogliosamente la propria parte per per evitare che qualcuno nel mondo pensi di poter impunemente invadere e soggiogare il proprio vicino calpestando il diritto internazionale e facendo valere la logica delle armi. Per noi, cari colleghi, la bussola in politica estera è sempre e solo l'interesse dell'Italia *(Applausi)* e difendere l'Ucraina significa affermare il diritto internazionale contro la prepotenza e difendere i confini europei e quelli dell'Alleanza atlantica.

autorevoli rappresentanti da poco eletti tra le fila del Partito Democratico quella NATO vorrebbero scioglierla. *(Applausi)*. Noi staremo sempre dalla parte di chi difende la libertà e la democrazia dai regimi autoritari. Al tempo stesso, l'Europa dovrà dare centralità al Mediterraneo, al rapporto col vicino Oriente e soprattutto con l'Africa, un continente che sta vivendo una fase di grande espansione, non soltanto demografica, e che dev'essere messo nelle condizioni di crescere, di svilupparsi e di dare un futuro ai propri figli. In questo il Piano Mattei lanciato dal Governo rappresenta davvero un cambio di paradigma: non si guarda più all'Africa come a una preda da spartirsi, ma nemmeno come a un continente che si può reggere soltanto sugli aiuti umanitari e che non potrà mai camminare con le proprie gambe. Il nostro è un approccio paritario, non predatorio e nemmeno paternalistico. Non vogliamo derubare l'Africa delle sue risorse e non vogliamo insegnare ai popoli africani come devono governarsi, ma vogliamo siglare accordi mutualmente vantaggiosi con loro e cooperare su tutte le questioni più rilevanti per l'Italia e per l'Europa, come la lotta al traffico di esseri umani, l'energia, la sicurezza alimentare, le infrastrutture e lo sviluppo economico. L'Italia di Giorgia Meloni ha fatto da apripista nella costruzione di un nuovo rapporto con l'Africa e ha fatto comprendere chiaramente all'Europa che il problema dei flussi migratori riguarda tutti i Paesi europei e non si può risolvere soltanto con la redistribuzione dei migranti. Bisogna lavorare con i Paesi d'origine e di transito dei migranti, sostenerli nel garantire ai loro cittadini il sacrosanto diritto a non emigrare *(Applausi)*, creare *hot spot* fuori dai confini europei ed evitare che siano gli scafisti a selezionare chi può entrare e chi non può entrare e chi non può entrare in Europa in base a quanto è disposto a pagare. Guardate, cari amici e colleghi della sinistra e dell'opposizione, che i dati del Ministero dell'interno ci dicono che gli sbarchi nel 2024 sono crollati a un terzo rispetto al 2023 *(Applausi)* e si sono significativamente ridotti anche rispetto al 2022, quando questo Governo non era in carica. Negli ultimi due mesi si è passati dai 23.000 dello scorso anno ai 9.000 sbarchi di quest'anno: quasi la metà dei 17.000 sbarchi del 2022, quando al Governo c'eravate voi. Presidente, certificano il successo delle politiche migratorie del Governo Meloni. E noi ci impegneremo affinché la nuova Commissione e il nuovo Parlamento che si stanno per insediare in Europa mettano il Mediterraneo, l'Africa e la difesa delle frontiere esterne in cima alla propria agenda. Le elezioni europee hanno dato un segnale molto chiaro, in Italia come nel resto d'Europa. I cittadini europei non vogliono più l'Europa della burocrazia, dell'iper-regolamentazione, del fanatismo *green* e della deindustrializzazione. deindustrializzazione. Vogliono l'Europa della crescita, del lavoro, dell'innovazione e dello sviluppo e un'Europa sempre più autosufficiente e indipendente, che sappia coniugare la sostenibilità ambientale con quella sociale ed economica. L'Europa del futuro deve cambiare passo. Basta direttive che distruggono la nostra industria automobilistica e il nostro patrimonio immobiliare in nome di un approccio ideologico che strumentalizza l'ambiente per colpire i veri obiettivi delle sinistre: la proprietà privata e le imprese. *(Applausi)*. La sinistra propone patrimoniali, espropri e occupazioni; ecco perché non stupisce che il vostro campo largo, che si fa rappresentare in Europa da chi, come Ilaria Salis, da esperta in materia, strepita in difesa del diritto a occupare le case altrui,

Per noi il lavoro, l'impresa e la proprietà privata sono sacri. Senatore Magni, non mi costringa a un provvedimento che non voglio prendere. È dall'inizio della seduta che la richiamo. Prego, senatore Speranzon, concluda, le do trenta secondi in più. noi siamo e saremo sempre diversi dalle forze politiche di colore rosso e verde che in Europa non si sono mai battute in difesa degli interessi concreti dei cittadini europei, men che meno di quelli italiani. Siamo anche diversi da chi tenta di avvelenare il clima e il dibattito politico in Italia, come in Europa, parlando di fascismo di ritorno, derive autoritarie o addirittura (coprendosi di ridicolo) di famiglie in crisi, persino di insonnia e depressione per il rischio di una vittoria della destra alle elezioni in Francia. Cari colleghi, siamo felici di distinguerci anche da chi, in un dibattito parlamentare sull'autonomia differenziata, minaccia nemmeno troppo velatamente gli esponenti di questa maggioranza, invocando piazzale Loreto, dicendo che con il *karma* non si scherza e che, prima o poi, noi, i nostri figli e i nostri nipoti la pagheremo! *(Applausi)*. Ma che significa, colleghi, che vorreste assassinarci tutti e appenderci a testa in giù? È questo? Chi semina odio non ci vedrà mai scendere al suo livello. I cittadini italiani l'hanno capito benissimo e l'hanno dimostrato con il loro voto, che ci ha premiato. Un voto che faremo pesare in Europa e di cui l'Europa dovrà tener conto.

Voglio ricordare che l'ordine degli interventi è dato dall'ampiezza dei Gruppi parlamentari: decidono i cittadini, con il loro voto, chi parla prima e chi parla per ultimo; tutto lì, non è che lo decido io. Comunico che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dal senatore Terzi di Sant'Agata, Zanettin, Murelli, De Poli e da altri senatori, n. 2, dal senatore Borghi

Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito breve, ma interessante, che offre alcuni spunti. Non tornerò sulle materie che sono già state

e poi riprendere la materia che è stata oggetto della gran parte degli interventi, relativa al posizionamento dell'Italia, ai suoi rapporti e alla discussione di merito e di metodo sulle prossime nomine di vertice dell'Unione europea. Intanto voglio ringraziare il collega Barcaiuolo, che ricordava nel suo intervento il tema dell'assegno unico. Ho parlato di questa materia anche questa mattina nell'Aula della Camera, perché è uno di quei temi che

ne ha aumentato le risorse per 3 miliardi. Tutti lo consideriamo un elemento fondamentale del nostro sostegno alle politiche di natalità, materia che, come sapete e come ho detto questa mattina nella mia relazione, credo debba essere portata a livello europeo perché c'entra con questo dibattito. Come sapete, colleghi, la Commissione europea ha recentemente deciso di aprire contro l'Italia una procedura d'infrazione contro l'assegno unico, ritenendo che, così come formulato - ricordo che lo riconosciamo a circa 6 milioni di famiglie italiane - sia discriminatorio e che l'Italia dovrebbe dovrebbe immaginare la stessa previsione anche per tutti i lavoratori stranieri e tutti i lavoratori extracomunitari, perfino per quelli che hanno figli in patria. Voi capite benissimo che, se seguissimo un'impostazione che considero molto irragionevole e abbastanza ideologica che ci viene indicata dalla Commissione, la misura sarebbe per noi insostenibile e l'unico risultato che avremmo sarebbe quello di togliere uno strumento fondamentale per circa sei milioni di famiglie italiane. Anche perché, come capite bene, conoscendo il funzionamento dell'assegno unico, diventerebbe molto difficile per il Governo italiano verificare il reddito ISEE di un lavoratore che viene magari dal Pakistan e ha i figli lì. Intendo quindi battaglia - e lo dico a nome del Governo italiano - contro questa iniziativa totalmente irragionevole della Commissione europea. Mi auguro che su questo si possa trovare il consenso dell'intero Parlamento darci una mano su una battaglia fondamentale. Queste sono alcune di quelle storie che raccontano e spiegano bene perché serva un approccio più pragmatico e meno ideologico a a livello europeo, da parte della Commissione europea e del Parlamento europeo. In Europa abbiamo un enorme bisogno di invertire la tendenza demografica, che è la madre di tutti i nostri problemi, banalmente perché, se dovesse andare avanti com'è, con nessuna delle Nazioni europee che raggiunge il cosiddetto tasso di sostituzione, cioè il numero di figli per donna necessario alla continuità delle nostre società, potremmo potremmo continuare a parlare di come investire sul *welfare*, di come modificare il nostro sistema pensionistico e di come dare una mano ai nostri lavoratori, ma fondamentalmente non saremmo in grado di sostenere il sistema di *welfare* e la civiltà che abbiamo costruito in questi decenni. Ci si aspetterebbe una discussione in Europa su una materia come questa e invece tutto quello che abbiamo visto per ora è che ci sono iniziative della Commissione che di fatto si dichiarano contrarie a provvedimenti che vanno nel senso di sostenere la demografia. Voglio dire alla senatrice Rojc, che parlava di forze disgreganti, che non so cosa si intenda esattamente con questa espressione, ma penso di poter dire cosa penso io che sia cosa penso io che sia disgregante, ovvero la linea politica di chi ha o sembra avere come priorità all'interno della costruzione europea l'obiettivo di mettere all'angolo intere Nazioni perché non si condividono i Governi che i cittadini di quelle Nazioni hanno scelto in libere elezioni. *(Applausi)*. Penso che questo sia disgregante e penso che sia particolarmente sbagliato in un tempo politico come quello nel quale viviamo, perché ne abbiamo parecchi di avversari, che si stanno organizzando e non credo che la cosa più intelligente da fare sia cercarne

dire da molti colleghi dell'opposizione - non me ne vogliano - su come si leggono le politiche europee. Vado alla questione delle nomine, delle competenze e dell'agenda strategica. Ribadisco quello che ho detto stamattina, vale la pena di tornarci su. Allo scorso Consiglio europeo, mi sono permessa di segnalare, rispetto a come si apriva e come si svolgeva quella riunione, una questione di merito e una questione di metodo, che intendo tornare a sottoporre all'attenzione del Consiglio europeo e che volentieri sottopongo di nuovo anche a voi. La questione di merito è la seguente: abbiamo fatto una campagna elettorale nella quale tutte le forze politiche in Italia e probabilmente quasi tutte le forze politiche in Europa

perché tutti ci rendiamo conto che l'Europa sta perdendo di competitività. I dati che il senatore Barcaiuolo ricordava nel suo intervento sono quelli che citavo questa mattina: il

La Cina era all'1,8 per cento del PIL mondiale nel 1990 e oggi è al 18 per cento del PIL mondiale. Ho detto questa mattina nella mia relazione - può essere una lettura che non si condivide - che, dal mio punto di vista, uno degli errori che l'Europa ha fatto è fatto è comportarsi in un modo un po' troppo autoreferenziale, guardando soprattutto al suo interno senza considerare quale fosse lo scacchiere che si muoveva intorno, come se in qualche maniera gli altri dovessero adeguarsi alle scelte che noi facevamo. Il mondo non è andato così, il mondo è andato in un'altra direzione. Sono state fatte scelte strategiche importanti, quella relativa alle catene di approvvigionamento su tutte o l'approccio che abbiamo avuto con la globalizzazione, che è un'altra critica che mi sono permessa di fare spesso. L'ho detto probabilmente già anche in quest'Aula: ricordo un mondo nel quale si diceva che il libero commercio senza regole

ha funzionato così: la ricchezza, piuttosto che distribuirsi, si è verticalizzata e si è concentrata e sistemi che erano meno democratici dei nostri, grazie a quel libero commercio senza regole, hanno guadagnato campo nel mondo e noi abbiamo perso terreno perché, perché, consegnando il controllo delle nostre catene di approvvigionamento, ci siamo trovati esposti a qualsiasi *shock*, e l'abbiamo visto quando è arrivata la pandemia e quando è arrivata la guerra. Abbiamo cominciato a correggere alcune scelte che erano state fatte, ma chiaramente ci vuole tempo e occorre stabilire le priorità adeguate. Sono riflessioni che si possono condividere o no, ma sicuramente tutti condividiamo il fatto che le cose così non stanno andando bene: bene: non vanno bene la ricchezza e la competitività delle nostre aziende; non va bene, come citava, se non vado errata, il senatore Monti, l'iperregolamentazione di cui questa Europa, nella foga di occuparsi di tutto, si è resa protagonista, facendo trovare tutte le sue imprese, ma particolarmente quelle piccole e medie, in una condizione di grande difficoltà per poter competere su mercati che intanto diventavano estremamente aggressivi (anche questo lo abbiamo visto).

che la pace che abbiamo avuto, e di cui sicuramente la costruzione europea è stata la principale protagonista, fosse qualcosa che potevamo dare per scontato. Un giorno, però, ci siamo svegliati e abbiamo scoperto che scontato non era; un giorno ci siamo svegliati abbiamo anche scoperto che, se chiedi a qualcuno di occuparsi della tua sicurezza, devi anche sapere che questo sarà un limite per la tua capacità di prendere le decisioni e che quindi la libertà è qualcosa che va difeso e ha un costo. Questo lo abbiamo scoperto noi italiani, ma l'ha scoperto l'Europa, che oggi deve correre ai ripari non solo sull'assenza di una colonna europea dell'Alleanza atlantica che, come sapete, auspico da tempo, ma anche proprio sulla sua capacità di avere un'industria della difesa e dei campioni europei della difesa che oggi

più volte denunciato in Consiglio europeo, cioè stabilire che abbiamo strategie e priorità, ma sia chiaro che non intende fornire agli Stati membri gli strumenti necessari a perseguirli. Pertanto, vogliamo sì una politica di difesa, la transizione energetica, la transizione digitale e la transizione verde, ma sia chiaro che ognuno si organizzi come può, perché non ci sono soluzioni diverse da dare. Io penso che su alcune grandi strategie necessarie necessarie all'Europa e alla nostra complessiva competitività si debba anche ragionare su quali sono gli strumenti che si mettono a disposizione per centrare quelle strategie. Sono analisi che abbiamo fatto tutti: le abbiamo fatte noi e sono state fatte all'interno dei partiti, nei Parlamenti e dai cittadini, che hanno fatto le loro scelte con il voto dell'8 e 9 giugno. Dopodiché, si arriva al primo Consiglio europeo successivo a quel voto

e, quando si arriva al Consiglio europeo, qualcuno prende la parola e propone chi debba ricoprire gli incarichi apicali, dopo che i negoziatori di alcuni partiti si sono visti e hanno stabilito quali nomi ricopriranno

questo merito postelettorale. Dopodiché, sul metodo voglio tornare su quello che dicevo questa mattina. Oggi vediamo tre partiti che si considerano una maggioranza e distribuiscono alcuni incarichi apicali. *(Commenti).* Lo vedremo in Parlamento, senatore Delrio, lo vedremo in Parlamento con il tempo. Fatemi finire il ragionamento, perché non mi risulta di avervi interrotto. Fatemi finire il ragionamento, perché vi spiego dove sto arrivando. Si considerano una maggioranza. Io credo che quella maggioranza sia molto fragile, ma non è questo il tema che mi interessa. Il problema è che, in teoria, le istituzioni europee non funzionano così. Quando gli incarichi apicali delle istituzioni europee sono stati immaginati, non sono stati immaginati in una logica di maggioranza e opposizione. Sono stati immaginati come incarichi neutrali, che dovevano garantire tutti gli

per gli incarichi apicali, indipendentemente dal fatto che vi siano una maggioranza e un'opposizione nel Parlamento, dice di seguire il peso politico che i cittadini hanno scelto di dare ai Gruppi presenti in Parlamento. Stamattina la collega Madia diceva, giustamente: presidente Meloni, lei si lamenta, ma la democrazia funziona così. Il Il Partito popolare europeo è il primo Gruppo del Parlamento europeo e quindi indica il Presidente della Commissione. Il Partito socialista il secondo Gruppo del Parlamento europeo e quindi indica il Presidente del Consiglio. I liberali sono il terzo Gruppo al Parlamento e quindi indicano l'Alto rappresentante.

al netto di quelli che possono essere i miei desiderata, una cosa del genere non è mai accaduta. Non è mai accaduto che, partendo da quelli che dovevano essere incarichi neutrali neutrali nella loro appartenenza politica, pur rispondendo a un'indicazione che arrivava dai cittadini, ma che non erano immaginati in una logica di maggioranza e opposizione,

su questo punto noi e voi proprio non la vediamo alla stessa maniera. Diceva il collega Scalfarotto: presidente Meloni, se lei non è d'accordo, quando arriva il Patto di stabilità dovrete fare la legge avrete dei problemi. Quindi, mi si sta dicendo che in Europa funziona così. Mi si sta dicendo che l'Europa aiuta o non aiuta gli Stati membri, che utilizza una linea o un'altra linea, se ci si piega o non ci si piega a quello che una presunta maggioranza ha deciso? Signori, è *outing*. Qui si sta facendo *outing*. In alcuni casi, io ho sostenuto che mi sembrava che alcune cose non accadessero nel modo giusto, ma penso che sia molto grave sostenere una cosa del genere.

Quindi, quello che spetta all'Italia, non è quello che le spetta in ragione del fatto che è un Paese fondatore, che è la terza economia europea, che è la seconda manifattura d'Europa, che è, tra le grandi nazioni europee, quella che ha anche il Governo più solido. No, dipende dal fatto che l'Italia dica sì o no a quello che alcuni hanno deciso. Non è la mia idea d'Europa e non è la mia idea di quale debba essere il ruolo dell'Italia. Non è la mia idea di quale debba essere il ruolo dell'Italia e, se qualcuno prima ha ragionato così, consentitemi di dire che questo mi chiarisce moltissime cose.

la consapevolezza di quale debba essere il ruolo dell'Italia non manca mai; manca solamente, a volte, da parte dei rappresentanti del popolo italiano e a me dispiace perché ci sono partite sulle quali, indipendentemente dal fatto che noi non siamo d'accordo sostanzialmente su niente, si dovrebbe lavorare insieme. Ho considerato anche abbastanza grave che proprio in queste ore e in questi giorni, di fronte a scelte che non solamente io considero francamente un po' bizzarre, anche nella metodologia (penso che in cuor vostro

non bisogna trattare con la Meloni *(Applausi)*. La Meloni fino a prova contraria è il Presidente del Consiglio dei ministri italiano, scelto dal popolo italiano e chi dice che non bisogna parlare con la Meloni sta chiedendo di escludere la Nazione che rappresenta *(Applausi)*. Anche questo è grave, consentitemelo, e lo dico da persona che all'opposizione non si è mai permessa di dire una cosa del genere, avendo fatto pure, come si sa bene, un'opposizione molto dura, perché ci sono delle cose che per me vengono prima del resto. L'interesse nazionale italiano per me viene prima degli interessi di partito. Il presidente Casini diceva di non sovrapporre i ruoli. Non intendo sovrapporre i ruoli; io sto sostenendo una tesi per quello che secondo me è il bene dell'Europa, perché se noi accettiamo delle logiche nelle quali ci sono delle debolezze in patria, i cui conti si saldano usando le istituzioni europee, ci facciamo molto male, ci facciamo molto male, particolarmente in questo contesto. Penso che dobbiamo uscire un po' dai nostri confini, perché le nostre - mi passi il termine - non facevano danni finché eravamo in pace, quando eravamo in un altro contesto. Oggi concentrarci sulle nostre microbeghe, dividerci fra di noi, può essere esiziale per il destino del continente europeo. Questo è il ragionamento che cerco di fare. Poi continueremo a non essere d'accordo su mille cose, ma mi sarebbe piaciuto - lo dico francamente - una volta tanto che si fosse potuto ragionare seriamente di questo, invece di continuare con l'etichetta «Sei amico di Orbán». Io queste semplificazioni nella politica estera francamente non le condivido e mi fanno anche abbastanza Diceva il collega Scalfarotto che noi blocchiamo l'unione bancaria. Collega Scalfarotto, la invito a approfondire: temo che lei non si sia accorto che a bloccare l'unione bancaria è la Germania prima di tutti, considerata forza europeistissima. Quindi, vi prego: queste semplificazioni lasciano il tempo che trovano e secondo me,

Orbán e il MES, prima con la Polonia, poi la Polonia ha eletto un Governo che adesso vi fa comodo ed è sparita dai radar *(Applausi)*. Queste sono le tre cose, ma sto cercando di fare un ragionamento più complesso; la campagna elettorale è finita, forse in questa occasione ci saremmo potuti permettere… sto finendo, perché è difficile intervenire, tra l'altro, quando si ha difficoltà con la voce. Quindi, la campagna elettorale è finita, apriamo una nuova legislatura europea, molto complessa, in un contesto estremamente complesso. Si può decidere di continuare

dell'uno, né dell'altro. Penso che debba difendere il suo interesse nazionale e, questo sì, vuol dire camminare a testa alta. Non l'ho visto accadere molto spesso, sicuramente lo vedo accadere adesso e penso che anche per questo, perché c'è un Governo capace di camminare a testa alta e di dire quello che pensa, di farlo lealmente, di farlo senza sotterfugi e senza andare in giro con il cappello in mano, l'Italia, anche in questa partita, porterà a casa quello che le spetta, indipendentemente dal fatto che io, come sempre, dirò quello che penso.

di risoluzione n. 2 del Gruppo Italia Viva esprimo parere contrario sulle premesse e contrario sull'impegno n. 8, favorevole sugli impegni n. 2 e n. 4, favorevole sull'impegno n. 1 con la seguente riformulazione: espungere le parole da "anche promuovendo" fino a "per l'Ucraina". parere favorevole sull'impegno n. 3 con la seguente riformulazione: espungere le parole "di un esercito comune e". dell'Unione europea e una politica migratoria solidale e umana, adoperandosi per garantire la sicurezza interna dell'Europa attraverso una gestione efficace e coordinata dei flussi migratori". Esprimo parere favorevole sull'impegno n. 6 con la seguente riformulazione: sostituire le parole "a sollecitare" con le parole "a facilitare", aggiungere dopo le parole "dell'Unione europea" le seguenti parole "ai Balcani occidentali" e espungere le parole "della Georgia e". Esprimo parere favorevole sull'impegno n. 7 con la seguente riformulazione: espungere le parole "in particolare le cosiddette «*dual

favorevole sull'impegno n. 1 con la seguente riformulazione: "a promuovere e rafforzare l'impegno nel sostegno politico, finanziario, economico, umanitario e militare all'Ucraina, attuando quanto previsto dal documento finale del G7 italiano del 13-15 giugno 2024;". parere favorevole sull'impegno n. 5 con la seguente riformulazione: sostituire le parole da "risoluzione fino al 2024" con le seguenti "risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2735". parere favorevole sull'impegno n. 7 con la seguente riformulazione: espungere le parole da "prevedendo" fino a "nel lungo periodo". Esprimo parere favorevole sull'impegno n. 9 con la seguente riformulazione: "a definire una strategia commerciale europea che identifichi e promuova *partnership* con Paesi e regioni affidabili, per ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione, nel rispetto delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio e degli accordi commerciali esistenti". Sulla proposta di risoluzione n. 5 del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra esprimo parere contrario sulle premesse

favorevole sugli impegni nn. 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 11. Esprimo parere favorevole sull'impegno n. 5 con la seguente riformulazione: "a sostenere ogni iniziativa delle Nazioni Unite volta a ottenere un immediato cessate il fuoco e la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani, tutelare l'incolumità della popolazione civile di Gaza, garantire la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi, sicuri e senza restrizioni all'interno della Striscia, rispettare la legalità internazionale e il ruolo dei suoi organi giurisdizionali, rilanciare il processo di pace". parere favorevole sull'impegno n. 8 con la seguente riformulazione: sostituire le parole "a sostenere" con le seguenti "a confermare". Esprimo parere favorevole sull'impegno n. 10 con la seguente riformulazione: dopo la parola "estremismi" aggiungere le seguenti "di ogni colore politico". parere favorevole sull'impegno n. 12 con la seguente riformulazione: espungere le parole da "unitamente" fino a "comune". Esprimo parere favorevole sull'impegno n. 13 con la seguente riformulazione: "ad avviare un dibattito nelle sedi istituzionali e con le parti economiche e sociali, orientato a definire le azioni e gli interventi in attuazione degli obblighi e delle scadenze da rispettare in relazione al nuovo Patto di stabilità". Infine, esprimo parere favorevole sull'impegno 15 con la seguente riformulazione. Si chiede di sostituire le parole "e in particolare negli" con le seguenti: "anche attraverso il conferimento di". finestra"). Colleghi, se c'è bisogno di qualche chiarimento potete richiederlo agli Uffici, perché capisco che la lettura possa avere dato adito a qualche

Signor Presidente, colleghi, è stata sottolineata in maniera ripetuta l'importanza dell'appuntamento in agenda. Le elezioni ormai si sono concluse, gli elettori europei si sono espressi, ora bisogna sciogliere i nodi politici e bisogna farlo possibilmente mettendo da parte propaganda e facili *slogan*. Mi verrebbe da dire che bisogna farlo ora o mai più, perché la sfida alla quale è chiamata l'Europa è una sfida esistenziale. Si è discusso di Ucraina, di Medio Oriente, di intelligenza artificiale, di cambiamenti climatici, di una visione industriale comune: sono sfide da far tremare i polsi e per le quali servirebbero vere *leadership* europee. Spiace invece registrare che ad oggi il dibattito attorno ai *top job* dell'Unione europea non sia stato all'altezza e soprattutto consapevole delle sfide geopolitiche alle quali l'Europa è chiamata. Voglio ricordare in quest'Aula e ribadire la nostra vicinanza e il nostro orgoglio per il contingente italiano che opera in Libano e in altri Paesi stranieri. Voglio ribadire che Azione è al fianco, con orgoglio, della Marina italiana, che guida una missione internazionale nel Mar Rosso; anche a quei soldati dobbiamo serietà, coerenza e verità. Se guardiamo lo scacchiere europeo, vediamo che l'asse franco-tedesco dalle elezioni europee è uscito indebolito. Potrebbe essere il momento dell'Italia. Il suo Governo, che pure è uscito premiato dalle urne, potrebbe svolgere una funzione importante, ma non mi pare stia andando così. Oggi l'Italia appare isolata, eppure di questo dato non solo noi non ci compiacciamo, ma riteniamo che l'Italia, indipendentemente dal colore politico di chi la governa, sia un Paese fondatore, uno dei primi Paesi europei dal punto di vista economico e quindi meriti Aggiungo anche che chi pensa di poter fare a meno dell'Italia e chi pensa di isolarla fa un danno alla stessa Europa. Anche l'Italia e anche questo Governo devono credere però di più nell'Europa, perché l'ondata di voti sovranisti non c'è stata e oggi bisogna prendere atto che non è possibile formare un Governo europeo senza popolari e socialdemocratici. Anche mettere insieme i diversi sovranismi è un qualcosa di molto complicato. Allora quale deve essere l'atteggiamento corretto nei confronti dell'Italia in questo delicato frangente? L'Unione europea non è il luogo dove proseguire una campagna elettorale permanente, ma una responsabilità, per la maggioranza, di anteporre l'istituzione agli interessi di partito e, per l'opposizione, quello di giocare la propria sfera di influenza non per danneggiare il Governo, ma per fare anche dall'opposizione gli interessi dell'Italia. Vengo non solo alle poltrone, come è stato detto, ma anche al tema dei contenuti e dei programmi. Cito velocemente le sfide, avendo pochissimo tempo. L'Ucraina: la prima minaccia è l'attacco all'Ucraina, perché quello è un attacco all'Europa, alle sue libertà, ai suoi valori. Su questo serve un punto di chiarezza tanto nella maggioranza quanto nelle file dell'opposizione, perché il sostegno all'Ucraina deve proseguire. Il sostegno ad un Paese in guerra, anche per la nostra libertà, si fa anche con le armi. Serve poi una forte soggettività europea e serve un'Europa forte anche per difendere la democrazia israeliana dai suoi nemici, per respingere l'antisemitismo dilagante anche in Europa, per proteggere il popolo palestinese non da Israele, ma dai terroristi di Hamas, e riaffermare una politica che si fondi sulla logica dei due popoli e due Stati, senza dimenticare il *pogrom* del 7 ottobre. Queste sono alcune delle sfide, unitamente anche alla sfida economica che Mario Draghi ha più volte sottolineato. Quello che serve sicuramente non è un'Europa dei nazionalismi e delle piccole patrie, ma un'Europa forte, con con la schiena dritta, capace di affrontare queste sfide con un autentico spirito europeo e quello che dobbiamo realizzare - dalla maggioranza chi è in maggioranza e dall'opposizione chi, come la sottoscritta, è all'opposizione

quello che sta per riunirsi è un Consiglio europeo cruciale, lo ha chiarito il presidente Meloni nella sua relazione e lo hanno determinato gli elettori con il voto della scorsa tornata di giugno, un voto che dimostra la nostra forza, il nostro radicamento in Italia e l'efficacia

Siamo tornati autorevoli e per questo possiamo rivendicare un portafoglio di rilievo nell'Unione, dobbiamo rivendicare un ruolo da protagonista nelle prossime trattative per i vertici europei, senza alcun tentennamento. Solo due giorni fa i dati arrivati dalla Commissione hanno certificato che siamo il primo Paese ad avere rispettato gli impegni presi col PNRR e ad aver potuto chiedere la quinta *tranche* del finanziamento con largo anticipo sugli altri. Una conferma importante è arrivata grazie grazie al lavoro del presidente Meloni, coordinato dal ministro Fitto, insieme alla proficua collaborazione degli enti locali. Siamo testa di serie in un cambiamento importante in atto nella nostra grande comunità europea, giunto a seguito di un forte impulso di questo Governo, che ha imposto la revisione e l'approvazione del nuovo PNRR, comprensivo anche del REPowerEU. Sul tavolo, ancora una volta, il tema della guerra in Ucraina, la sicurezza e la difesa comune, la pace, la crisi a Gaza, i nomi che guideranno le istituzioni europee, la crescita economica, la gestione dei flussi migratori con il prosieguo della politica dei patti con i Paesi africani. Le questioni da affrontare sono molteplici e per ognuno il contributo del nostro Paese è risultato fin qui centrale. L'Italia si è ritagliata un ruolo chiave e non si possono ignorare i segnali che sono fin qui arrivati. Dobbiamo preparare il terreno per garantire l'unità dell'Unione europea e la sua stabilità attraverso una *leadership* che che ascolti tutte le forze che sono uscite vincenti e rafforzate dalle urne, un'indicazione che è lo specchio di politiche ben precise sull'immigrazione, come sulla crescita e su come si dovranno declinare le questioni della transizione energetica e digitale. Partendo dal primo punto, se l'Europa vuole continuare ad essere ago della bilancia per la sua storia e la sua posizione nel mondo, è inevitabile che il sostegno all'Ucraina debba continuare con forza come questo Governo ha sempre garantito insieme a tutte le forze di centrodestra. Continuiamo a perseguire la pace, ma una pace giusta, per la quale è imprescindibile che l'Ucraina continui nella sua autodifesa, grazie al sostegno dell'Europa e della NATO e naturalmente un piano di pace senza l'indirizzo di un'Unione europea forte non è minimamente pensabile. L'esito delle elezioni europee contribuisce a delineare i rapporti di forza tra i vari Gruppi politici, ma nella scelta dobbiamo tenere in conto e in considerazione anche gli impegni presi e la salda collocazione atlantica del nostro Continente. L'accordo politico su cui i *leader* hanno lavorato è stato pensato da tutti i Paesi fondatori, e non solo, per continuare a dare stabilità, coesione e forza alle future scelte delle istituzioni europee e per garantire quella libertà e quei principi democratici che sono alla base della nascita della stessa Unione. Per quanto riguarda il nuovo assetto dei vertici delle istituzioni europee, è chiaro che l'asse sulle priorità programmatiche del semestre, dall'immigrazione alla sfida demografica e alla determinazione della sovranità dell'Unione europea, dovranno orientare le scelte che saranno prese dai *leader* a Bruxelles. Solo ragionando su basi programmatiche si potrà dare all'Europa una giusta guida. Sull'immigrazione si apre un altro capitolo fondamentale. L'Italia ha indicato la strada per politiche di gestione dei flussi realmente comunitarie, orientate a un coinvolgimento stabile dei Paesi africani e mediterranei tutti; un elemento che consentirà di capire anche come i confini dell'Unione potranno ampliarsi a seguito della condivisione di politiche di gestione dei flussi che non pesino solo ed esclusivamente sulle spalle dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, tra cui l'Italia. Il superamento di questi schemi è arrivato grazie alle politiche portate avanti dalle forze di centrodestra, determinando cambi negli equilibri politici degli altri Paesi che sono emblematici. Penso, ad esempio, alla Francia, che presto andrà al voto, ma anche alla Germania e alla Spagna, dove le forze socialdemocratiche hanno subito un ridimensionamento chiaro, inevitabilmente collegato alle politiche economiche che non mettono al centro protezione e competitività. L'Italia ha dimostrato che serve maggior flessibilità delle politiche finanziarie e che i conti devono essere in ordine solo per consentire ancor più investimenti e sviluppo. L'*austerity* fine a sé stessa ha fallito. Le imprese ci chiedono un cambio di passo per affrontare alla pari le sfide che arrivano dai nuovi Paesi del blocco asiatico. Dobbiamo proteggere i nostri *asset* e promuovere gli investimenti, facendo pesare sempre meno una burocrazia elefantiaca e non in linea coi tempi che viviamo. Anche in questo il nostro Governo ha dato una sveglia a tutti gli altri Paesi. Identica questione si pone sul fronte energetico. La partita per l'Europa è fondamentale, se non vogliamo continuare ad essere un gigante coi piedi di cristallo. Il nostro Paese potrebbe assumere una nuova centralità in qualità di garante della sicurezza energetica europea. Est-Ovest, basato sull'interdipendenza energetica tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Russia, si è infatti disgregato, lasciando uno spazio immenso all'eventuale sviluppo di un nuovo asse Sud-Nord. In questo scenario, l'Italia può diventare una cintura energetica con un nuovo ruolo strategico; ruolo rivendicato attraverso il Piano Mattei, un progetto ambizioso della nuova gestione dei flussi migratori attraverso il sostegno diretto alle popolazioni africane. Dobbiamo guardare all'importanza del gas naturale, che in questa crisi energetica ha dimostrato ancora una volta quanto potenziale ci sia nel continente africano e nel Mediterraneo allargato, come alternative strategiche al blocco che sta a Est. In ultimo, la questione della transizione energetica e delle politiche *green*, che in questo momento stiamo mettendo a terra attraverso la realizzazione del PNRR. Nessuno nega i cambiamenti climatici e l'urgenza di politiche di difesa del suolo e di contrasto ai fenomeni estremi sempre più frequenti. Purtroppo abbiamo visto con le ultime alluvioni, ad esempio in Veneto e in Lombardia, quanto sia necessario invertire la rotta, ma possiamo farlo coniugandolo allo sviluppo economico, che non deve essere penalizzato. Dobbiamo accompagnare il cambiamento culturalmente, senza prevaricazioni e con attenzione alla sostenibilità di tutte le scelte che faremo. il peso storico delle scelte che andremo a compiere e che porteremo in Europa perché, come hanno detto in tanti, queste sono state le elezioni più importanti della storia dell'Unione, siamo a un bivio fondamentale. Per tenere saldo il nostro progetto europeo dobbiamo cambiare ora, oppure non avremo molto altro tempo, come si vince anche dalla disaffezione che i cittadini hanno dimostrato per questo voto, praticamente in tutti i Paesi membri. Per farlo, l'Italia, come Paese fondatore dell'Unione, dovrà avere un ruolo di massimo rilievo nel nuovo assetto istituzionale europeo, perché riteniamo che così avremo capacità e forza per promuovere quel cambiamento che i cittadini col voto europeo hanno sollecitato. Il popolo, come ha detto lei, presidente Meloni, ha dato un'indicazione chiara. Giochiamo una partita che vale il bene, non di questo o di quel partito, ma dell'Italia e degli italiani. Questo è lo spirito con cui dobbiamo muoverci alla vigilia di questo importante appuntamento nell'agenda europea

Presidente, signora presidente Meloni, lei ha sottolineato più volte che il popolo europeo ha dato un'indicazione chiara. Questa indicazione, però, dice che le destre sono il primo partito solo in cinque Paesi. In tutti gli altri hanno vinto i popolari, i socialisti e i liberali. Infatti, questi partiti sono in grado di individuare i *top job* proprio perché hanno la maggioranza dei voti. Allora, temo che non saranno i popolari a dover decidere tra i verdi e i conservatori, ma sarà lei a dover decidere da che parte stare giocare fino in fondo il ruolo di guida morale della destra estrema, insieme ad Orbàn e Le Pen, oppure sostenere la maggioranza ed avere un peso sulle questioni che qui ha illustrato. Purtroppo, su questa cruciale questione, lei non ha ancora dato una risposta. In compenso, ci ha illustrato con chiarezza la sua visione dell'Europa. Un'Europa delle nazioni, che fa poche cose e le fa bene, senza intromettersi nelle decisioni che gli Stati possono prendere autonomamente. Ci si chiede quali sarebbero queste poche cose che dovrebbe gestire l'Europa. Questa risposta ce la dà lei. Oltre alla difesa comune e alle politiche migratorie, gli investimenti. Tradotto: l'Europa dovrebbe fornire i soldi, come è successo col PNRR, ma non immischiarsi su come vengono spesi; non avere una linea politica sul futuro del continente; non deve intromettersi su come abitiamo, cosa mangiamo e come circoliamo, come lei ha sottolineato spesso. Ma un'Europa così non funzionerà, perché quelle che voi chiamate intrusioni, sono, in realtà, principi solidaristici senza i quali semplicemente l'Unione non esisterebbe. Lei ha sottolineato che l'Europa è troppo occupata con sé stessa senza guardare al di fuori dei suoi confini. Io temo che questo valga soprattutto per approcci come il suo. Perché altri Paesi dovrebbero aderire alla logica dell'Italia *first* o dell'Ungheria *first*? Sarebbe la fine dell'Europa che è basata su uno spirito dove tutti gli Stati devono anche dare e preoccuparsi degli altri. Soprattutto, presidente Meloni, perché tutti quelli che non la pensano come lei devono essere definiti ideologici? Ma ci vuol far credere davvero che la destra non abbia un'ideologia? Che le vostre posizioni sul MES, sull'aborto, sui diritti LGBTQ e sulla maternità surrogata non siano legate a una precisa ideologia? Questa accusa di essere ideologici vale in particolare per quelli che hanno una posizione più rigorosa sulla transizione ecologica. Sono d'accordo che dobbiamo tutelare le donne e gli uomini che nella natura vivono e lavorano. Soprattutto le piccole aziende di montagna devono essere meglio sostenute. Una decisa azione di contrasto all'*italian sounding* e la risoluzione del problema dei grandi carnivori, che non sono più in pericolo di estinzione. Trovo, invece, irresponsabile raccontare ai cittadini che possiamo salvare il Pianeta mantenendo tutte le nostre abitudini, così come sono sempre state e senza alcun sacrificio. Chiedo se sia più ideologico chiedere di ridurre il consumo di carne o vietare la produzione di carne coltivata, che tra l'altro non esiste neanche. Per quanto riguarda le politiche demografiche, non è vero che tutti i Paesi europei sono sullo stesso livello. Se andiamo a vedere il tasso di fertilità, ci sono Paesi dove le cose vanno decisamente meglio rispetto all'Italia e sono proprio quei Paesi dove è più alta l'occupazione femminile. È alla loro esperienza che bisogna guardare, alle misure che hanno introdotto, più di vent'anni fa, anche in termini di equa distribuzione tra i genitori dei compiti di cura familiare. In quei Paesi non solo i mesi di congedo parentale sono ben retribuiti, ma ci sono anche dei meccanismi premiali per quei genitori che si dividono equamente i mesi di congedo e, se non si riesce ad aumentare la natalità, l'unico modo per non collassare demograficamente è puntare sull'immigrazione. In Italia, invece, manca completamente una politica dell'integrazione e anche la sua narrazione che, grazie al suo Governo, l'Europa ha cominciato ad affrontare la questione, non è corretta. È già da tempo che in Europa se ne discute, solo che tutti i Paesi si confrontano con un lato diverso della problematica. Vede, qualche settimana fa uno dei suoi compagni di partito mi ha rimproverato di non sapere bene l'italiano. Ebbene, il mio italiano non sarà perfetto, ma il mio tedesco lo è e pertanto riesco a seguire i dibattiti anche in Germania e Austria. Mentre in Italia ci si lamenta di essere il Paese di primo approdo, quasi tutti i migranti cercano di raggiungere la Germania, l'Austria e la Svezia, perché lì ricevono una specie di reddito di cittadinanza, a differenza dell'assegno unico che l'Italia, ripresa dalla Corte europea, cerca di dare solo agli italiani, ma, come abbiamo sentito oggi, anche la Corte europea, che applica solo la legislazione All'interno dell'Unione deve esserci una comprensione dei problemi degli altri e deve esserci una maggiore integrazione per uniformare i sistemi fiscali e sociali. Noi del Gruppo per le Autonomie siamo federalisti, siamo per un'Europa delle Regioni e per questo abbiamo sostenuto anche la vostra legge sull'autonomia differenziata. Pensiamo che i troppi nazionalismi ci portino indietro ai tempi bui, quando, come lei stessa dice, i Paesi europei erano in guerra tra di loro. Questo non vuol dire non cambiare niente in Europa. Anzi, l'Europa deve adeguarsi alle nuove sfide, deve costruire una difesa comune e introdurre il principio di maggioranza. Certamente possono essere criticate certe derive, ma sempre in un'ottica costruttiva e non distruttiva. Pertanto, speriamo che lei, presidente Meloni, domani faccia la scelta giusta, collocando l'Italia dalla parte dell'Europa che conta, non dalla parte dei sovranisti, che di sicuro non rappresentano il futuro. degli interventi della presidente del Consiglio Meloni si può dire ovviamente bene o male, ma nessuno può metterne in discussione due caratteristiche: la chiarezza e anche l'onestà intellettuale. Perlomeno è sempre stato così, a giudizio di uno che ha contestato quasi sempre i suoi interventi. Oggi mi pare che queste due caratteristiche siano venute meno, tanto la chiarezza quanto l'onestà intellettuale, perché, se capisco bene, il *fil rouge* dell'intervento della Presidente e delle sue repliche è «vogliono fare un torto all'Italia, ci tengono fuori dalla stanza dei bottoni, pur avendo noi ottenuto un grande risultato alle europee». È vero, questo ragionamento? Io credo di no. Non vogliono fare un torto all'Italia; in un gioco politico, dentro le regole europee, vogliono premiare una linea politica che non è quella del Partito europeo che Giorgia Meloni presiede. Questo passaggio è molto importante, perché noi dobbiamo essere onesti intellettualmente, innanzitutto noi, perché la Meloni in Italia le elezioni le ha vinte, noi no. Il nostro sogno idealista degli Stati Uniti d'Europa è andato a sbattere. La mia onestà intellettuale sta nel dire in questa sede che tutto quello che noi avevamo detto in campagna elettorale non è stato accolto dai cittadini, quello che ha detto la presidente Meloni sì. La presidente Meloni ha preso il 29 per cento e diceva: votate me, votate la Meloni, votate Giorgia e io avrò i voti per contare in Europa e per cambiare l'Europa. Questa era la campagna elettorale: noi a parlare di Stati Uniti d'Europa e di Ventotene, la Meloni a dire «votate Giorgia». Cosa è accaduto? È accaduta una cosa naturale. Il vice presidente Tajani e il ministro Fitto potranno confermare alla Presidente quello che sto dicendo. Già in altri momenti della vita istituzionale europea si è avuto un voto non unanime sui *top job*; nel 2014 chi vi parla ne fu testimone. Quando si trattò di votare Jean-Claude Juncker, espressione del Partito Popolare Europeo (non del PD, non della sinistra), David Cameron a lui) e Viktor Orbán (allora iscritto al PPE) votarono contro Jean-Claude Juncker e il giorno dopo lavorarono insieme. Può accadere la stessa cosa. Si legge che l'Italia, la Slovacchia e l'Ungheria siano contro. Non lo sappiamo, ma questo non è un atto contro l'Italia; è un fatto politico, cioè i numeri in Europa contano. Io vorrei un sistema in cui si fa l'elezione diretta del Presidente della Commissione europea. L'ho proposto in tutta la campagna elettorale ed ero l'unico che parlava di questo evidentemente non ha riscosso un grandissimo successo, vedendo i risultati. Quello però che voglio dire a lei, signora Presidente, per il tramite del Presidente del Senato, è che da lei ci aspettavamo un discorso di chiarezza e di onestà intellettuale. Ci aspettavamo che lei venisse qui e dicesse: siccome ho detto che l'Europa va cambiata e ho chiesto i voti per contare, dico no a Ursula von der Leyen, perché ritengo che i cinque anni appena trascorsi siamo stati un fallimento. Questo discorso lo avrei apprezzato, perché avrebbe avuto una logica. Ursula von der Leyen, con il *green deal*, la debolezza (dico io) sullo Stato di diritto, e le incertezze sulla politica estera, va mandata a casa. Questo discorso dalla Meloni ce lo saremmo atteso. ci saremmo attesi un discorso uguale: ho detto di no a tante cose, ma ho ottenuto qualcosa per cui dico sì ai prossimi cinque anni di Ursula von der Leyen e credo che questo sia un legittimo atto politico. Lei, presidente Meloni, è venuta qui e ci ha riempito di un grande forse. Ci ha raccontato una storia a metà tra la grande statista e la piccola fiammiferaia: la grande statista che ha la forza per poter cambiare il mondo, la piccola fiammiferaia che si lamenta perché non la chiamano ai caminetti. E lo dice alla sinistra. non faccia difendere la sinistra a me, Presidente, la prego. Ma, se lei vuol sapere chi non l'ha chiamata ai caminetti, si volti piano piano verso destra (piano piano, è Tusk che ha detto «non voglio parlare con la Meloni» ed è iscritto al Partito Popolare Europeo. *(Applausi)*. È Mitsotakis che l'ha chiamata per dire che avrebbero votato una persona una persona e che lei non era stata coinvolta nell'accordo. Non faccia fare questa parte a me, signora Presidente, la prego. Per l'antico rapporto personale, abbia l'onestà intellettuale di dire che non è che non hanno rispetto per l'Italia: non vogliono lei e le sue idee politiche. O forse la vogliono, ma allora lei si deve chiarire. Sgombriamo il campo da un punto e poi veniamo alla fine. Lei dice tutte le volte che quelli di prima non ottenevano risultati; ora c'è lei e si ottengono i risultati. vent'anni) hanno preso una Presidenza di Commissione, un Alto Rappresentante, due Presidenti del Parlamento europeo e un Presidente di Banca centrale europea. Ed hanno idee diverse, perché una volta c'era il Governo d'Alema, una volta Renzi, una volta Conte, una volta Gentiloni, una volta Berlusconi. All'Italia i *top job*, con maggioranze diverse, li hanno sempre dati. Se stavolta non glieli vogliono dare, non è un problema della bandiera e del tricolore; il problema è che lei non ha avuto la forza di fare le maggioranze necessarie al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e alla Commissione europea. Questo è il punto cruciale del nostro ragionamento, se vogliamo prendere sul serio ciò che dice Meloni, e io sono per prenderlo sul serio, anche nella parte che non condivido. Il passaggio sul libero mercato senza regole come causa del declino europeo non lo condivido. Ritengo che ci sia un declino europeo e apprezzo i dati che la Presidente ha offerto, anche in ordine al PIL, penso che ci sia un declino anche demografico, oltre che economico, e condivido il fatto che l'Europa sia un meccanismo che non funziona per la crescita; però non credo che il problema sia stato il libero mercato senza regole, perché anzi, al contrario, dico che di regole ce ne sono state fin troppe. L'America inventa, la Cina copia, l'Europa regola; è un qualcosa che non può funzionare. Ma quello che per me è chiave in questa discussione è capire se abbiamo un'idea che il nostro Governo porta, che è legittima. Il Governo, condiviso da una percentuale importante degli elettori, ha tutto il diritto di scegliere quello che crede: sia di votare la von der Leyen che di votare no. Il problema è che il Governo al suo interno è diviso nelle forze politiche - anche questo argomento dobbiamo avere il coraggio di dirlo - perché la Lega è per il no alla von der Leyen; perché il PPE ha portato la von der Leyen come *Spitzenkandidat*; perché Fratelli d'Italia si trova nella scomoda posizione, che peraltro è molto più comoda che stare all'opposizione, di essere costretto a fare una scelta. Non venite però ad attaccare noi, non venite a giocare la carta dell'*escalation* verbale. Abbiate il coraggio di dire: abbiamo un problema, dobbiamo risolverlo; questo si chiama politica. Quando qualcuno in Aula le dice che lei deve finire a testa lei ha e avrà sempre la nostra solidarietà. *(Applausi)*. Chi dice frasi del genere non soltanto è profondamente in errore, ma utilizza un linguaggio verbale di odio. di odio. Presidente La Russa, lo dico a lei perché lo riferisca ai colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia: in questi anni di espressioni di odio verbale ne abbiamo sentite da tante parti e noi di solito ne siamo stati oggetto da parte di tutti, siamo stati collante costituzionale, cioè le prendevamo da destra e da sinistra, le prendevamo dagli uni e dagli altri. Lo dico alla Presidente del

che, proprio a proposito del linguaggio d'odio, quel cognato è stato assolto perché il fatto non sussiste *(Applausi)*; eppure non una dichiarazione è arrivata da Fratelli d'Italia o dal «Fatto Quotidiano», che erano i due soggetti che la Meloni citò in quel video. Il punto finale qual è? La presidente Meloni ha ragione a dire che noi viviamo una stagione complicatissima. Sono davvero profondamente d'accordo con lei, perché penso che mai come in questo momento abbiamo una situazione di crisi. Cito Ronald Reagan, sì, lo faccio io: sappiamo bene, fin troppo bene - diceva il presidente Reagan nel 1980 - che la guerra non arriva quando le forze della libertà sono forti; la guerra arriva quando le forze della libertà sono deboli. La guerra che sta dividendo il nostro mondo è una guerra che deriva dal fatto che le forze della libertà sono deboli e che l'Europa è debole. Dobbiamo lavorare insieme dando sostegno al Governo e a tutte le forze della libertà perché questo non accada. Ha ragione la Presidente del Consiglio a dire che c'è un grande tema complessivo. Pensate soltanto al 7 ottobre: l'attacco di Hamas doveva dividere i Paesi arabi, ma ha finito con il dividere la cultura occidentale e le università occidentali; ha finito con il dividere nel profondo la nostra stessa comunità civile. Quello che però manca

L'intelligenza artificiale porterà all'esplosione dei *data center*; il petrolio, che tutti dicevano avere le ore contate, ha i secoli contati, non le ore contate. Abbiamo una vicenda totalmente nuova da scrivere insieme, però per farlo, signora Presidente, ci risparmi i toni da vittima e ci dia indicazione su dove vuole andare. Noi potremmo dirle di sì o di no, ma non accetteremo mai di essere considerati come dei disturbatori, perché quello che vogliamo chiederle è chiarezza e onestà intellettuale, che nel suo intervento stavolta non ho trovato.

che l'Europa debba cambiare radicalmente e che questo messaggio sia arrivato in maniera molto chiara dall'elettorato qualche settimana fa. Tra gli elementi critici citati però da lei, presidente Meloni, mi dispiace dirle che è del tutto assente quello principale, la ragione principale di questo cambiamento richiesto, cioè le immense e crescenti diseguaglianze economiche che oggi flagellano l'intera Unione europea. Questo e non altri è il motivo vero della sfiducia, della disaffezione, dell'astensionismo.

Come sappiamo, il problema centrale che il prossimo Consiglio affronterà sarà il tentativo di trovare un accordo sui vertici delle istituzioni europee, stiamo parlando di questo. A me pare evidente, Presidente, al contrario di quello che avete raccontato nelle scorse settimane su una presunta centralità italiana, l'isolamento, invece, del suo Governo. Glielo dico senza nemmeno particolare soddisfazione,

e dall'avvio di una procedura di infrazione che rischia di essere pagata a prezzo molto caro da tutti i cittadini, soprattutto da quelli più deboli. All'Italia servirebbero autorevolezza e alleanze per chiedere una revisione delle regole di *governance* dell'Unione, per provare, per esempio, ad avviare politiche anticicliche, cosa difficile perché si dà il caso non sia dovuto semplicemente a questioni di politica interna francese o tedesca, che pure ci sono, com'è stato detto da molti colleghi nei loro interventi, ma anche dalla poca credibilità della sua maggioranza di governo, signor Presidente. Se ogni giorno tra di voi viene fuori qualcuno che inneggia alla X Mas e poi un'altra volta viene fuori qualcuno che è nostalgico del Ventennio e poi un'altra volta viene fuori qualcuno che addirittura declama gli *slogan* della vecchia Germania nazista, senza che dai vertici dei vostri partiti e men che mai dal Governo arrivi non dico una drastica sconfessione,

si è soffermata molto poco sulla guerra in Ucraina, lo ha fatto soltanto per confermare le scelte politiche compiute fin qui dall'Europa ignorando, io credo, il fallimento, purtroppo, di quella strategia. Davvero non so come si faccia a non vedere che soltanto la ripresa, anzi l'inizio di una reale iniziativa diplomatica possa mettere in difficoltà Putin; l'Europa - l'ho detto tante volte in tutti questi mesi - dovrebbe smettere, dovrebbe smettere, anzi, di abdicare al proprio ruolo e dovrebbe iniziare a muoversi con la propria autonomia, esattamente come dovrebbe provare ad avanzare una proposta per fermare la mattanza nella Striscia di Gaza, alla quale noi tutti assistiamo con un'indifferenza che in futuro sarà considerata alla stregua di un crimine. Non ho problemi a dire che sul conflitto russo-ucraino il Governo italiano abbia fatto bene ad opporsi all'uso delle armi fornite a Kiev per colpire il territorio russo. È certamente un passo in avanti, ma non è abbastanza, presidente Meloni: bisognerebbe avere il coraggio di ammettere che la strada che è stata seguita finora, quella della sola fornitura di armi a Kiev, non solo non è servita a cambiare il corso della guerra e a fermarla, ma purtroppo non ha impedito le tragedie che ci sono state in tutti questi mesi e che all'inverso ha facilitato l'*escalation*

su tutt'altro argomento. Nelle dichiarazioni di autorevolissimi esponenti del Governo italiano appare evidente l'intenzione di mettere una pietra tombale sul *green deal*, che pure appariva, soltanto qualche anno fa, la grande sfida che l'Unione europea metteva in testa alla lista delle sue priorità. Voi liquidate quel progetto parlando di ecologismo fondamentalista, come se i cambiamenti climatici, Presidente, fossero una teoria politica e non invece una clamorosa e drammatica realtà. Questa è davvero una scelta gravissima, non solo nei confronti delle generazioni più giovani e di quelle che verranno, ma perché rischia di rendere l'Unione un soggetto insignificante su un fronte essenziale anche dal punto di vista economico, come quello della transizione energetica.

Da giorni sentiamo ripetere che questo hanno chiesto i cittadini europei con il voto per le forze di destra: il pugno duro contro l'immigrazione. Lasciatemi dire innanzitutto che le cose non stanno esattamente così come le raccontate.

non è certamente avanzata in Italia (si sbaglia su questo il senatore Renzi), dove la destra perde oltre un milione di voti, anche perché evidentemente sempre più nel nostro Paese diventano chiari agli elettori i vostri intendimenti, come quello vergognoso della secessione dei ricchi attraverso quello scellerato progetto che si chiama autonomia differenziata. *(Applausi)*. È talmente chiaro, peraltro, che avete perso le elezioni,

per tornare all'Europa, penso che bisogni dire con chiarezza che le politiche che avete in mente sull'immigrazione sono del tutto inefficaci sul versante del contrasto all'immigrazione clandestina, ma sono purtroppo efficacissime per agevolare la riduzione in schiavitù di migliaia di persone, come oggi ci accorgiamo drammaticamente dopo la morte - anzi, l'omicidio - di Satnam Singh. Singh. Ho finito davvero, signora Presidente, ma penso che su questo punto, anche alla luce di quello che è successo nei giorni passati, se sono vere le parole che la presidente del Consiglio Meloni ha voluto dire stamattina, stamattina, rammaricandosi ovviamente e naturalmente di questa drammatica vicenda, se fossimo conseguenti, dovremmo fare una cosa sola: abolire il prima possibile la legge Bossi-Fini,

L'Europa, del resto, non dev'essere solo produttrice di regole per legare e per bloccare, ma deve indicare obiettivi di crescita; non dev'essere soltanto, com'è stato detto stamattina alla Camera, un gigante burocratico; dev'essere piuttosto un faro puntato verso il futuro.

da chi ci invade, perché ci sono anche guerre ai confini d'Europa e diremo che abbiamo i conti in regola e comanderanno altri. Sarebbe un paradosso. Teniamo i conti in regola, però restiamo vivi con il nostro sistema produttivo e con le nostre popolazioni. Parliamo della concorrenza sleale anni fa ha fatto la scelta della via della seta, svendendo gli interessi del nostro Paese; noi ce lo ricordiamo questo fatto, non ce lo siamo dimenticato. Oggi si impongono dazi, lo decide l'Europa; non è una politica illiberale, anzi è tesa a garantire una concorrenza normale. L'auto elettrica non potrà essere importata solo dalla Cina; vogliamo avere un'industria che possa essere competitiva. Servono quindi tempi diversi per avere un'industria quantomeno europea, magari italiana, che ci possa dare prodotti che non dobbiamo per forza di cose acquistare solo dagli altri. Forza Italia ha l'orgoglio di far parte del Partito popolare europeo, prima forza politica del continente, che ha vinto le elezioni e che reclama il giusto spazio al vertice delle istituzioni europee. Voglio citare il vice presidente del Partito popolare europeo, che è qui presente, perché è anche vice presidente del Consiglio, bisognerà tenere conto della nuova situazione europea e dei risultati ottenuti dai singoli Gruppi. Il PPE ha vinto, i socialisti non hanno vinto, i liberali hanno avuto delle difficoltà. Il PPE dev'essere tenuto in grande considerazione per i vertici apicali. Giorgia Meloni è il capo dei conservatori, famiglia politica storica, che ha già avuto incarichi e ruoli in Europa e che quindi ne potrà rivestire ancora. Il fatto che al Governo italiano, poi, ci sia una forza centrale come la nostra, riferito a Forza Italia nel Gruppo PPE, rende più forte il Governo italiano e quindi anche la nostra *Premier*. Come Italia, ha detto Tajani, chiederemo un Commissario di peso e un Vice Presidente. L'Italia merita un ruolo centrale. Bisogna allargare la maggioranza. Le elezioni hanno parlato chiaro. Sull'ambiente serve una terza via che non sia negazionista, ma nemmeno estremista, come quella di Greta Thunberg e Frans Timmermans. Quindi, non ci si può alleare con i Verdi. Questa è la posizione che è stata espressa dal Vice Presidente del PPE, segretario anche del nostro partito: è dunque una posizione che non posso non condividere, ma la condivido realmente, non solo per disciplina. Noi non vogliamo l'agenda Timmermans o l'agenda Greta. Vogliamo un'agenda dell'Europa come quella che indica soprattutto il Partito Popolare Europeo. In primo luogo, dire con chiarezza che l'Europa deve avere un ruolo importante: i singoli Stati da soli e le singole Regioni non vanno da nessuna parte. Il presidente Meloni ha presieduto con grande capacità il G7. L'India nel 2023 ha superato come popolazione la Cina:

Dobbiamo essere uniti per poter contare e guardare al futuro. Dobbiamo avere un'industria attiva e produttiva. Serve acciaio. Dobbiamo fare delle navi per mandarle nel Mar Rosso, a difendere la libertà dei commerci. L'acciaio ci serve per difenderci dai fondamentalisti Houthi che costringono le navi a costringono le navi a fare il periplo dell'Africa con costi, alla fine, anche per i nostri consumatori. Serve un'industria anche per avere una difesa. Non possiamo fare programmi. Tutti vogliamo un mondo meno inquinato, ma anche un mondo in cui siamo vivi. difesa europea, dobbiamo svincolare le spese per la difesa dai parametri e dai limiti di bilancio. Dobbiamo raggiungere il 2 per cento che la NATO ci chiede rispetto al PIL, ma dobbiamo farlo con una flessibilità diversa. Voglio anche oggi ricordare che il generale Graziano ci indicava come obiettivo, presiedendo il Comitato europeo di difesa, una difesa europea che ancora non c'è, ma che ci dovrà essere. Dobbiamo difendere la nostra agricoltura e dobbiamo avere una politica seria per l'immigrazione. Noi vogliamo dare in Africa, col Piano Mattei, un futuro a milioni di africani: non un seggio a uno solo, che poi viene espulso dal partito che gli ha dato il seggio. Questa, infatti, è stata la politica dell'immigrazione di qualcuno. Noi li vogliamo aiutare tutti ad avere uno sviluppo e un lavoro. Il Piano Mattei ha avuto attenzione nel G7, che non era frequentato da sprovveduti; e in quest'Aula del Senato abbiamo fatto un vertice importantissimo con tanti Paesi africani. Sulla vicenda di Latina, signor Presidente del Senato, mi chiedo come mai la magistratura, sempre così attiva, sia stata così lassista nei confronti di un protagonista italiano di una storia di orrore: si muovano; arrestano tanta gente, non arrestano quelli giusti, qualche volta, ci viene da dire. viene da dire. Serve buonsenso anche nella transizione verso un traguardo ambientalista migliore. Noi vogliamo difendere la flora e la fauna, ma pensiamo anche alle politiche per la natalità e la famiglia. C'è una questione antropologica primaria, cioè la presenza dell'essere umano, che va salvaguardata. Dobbiamo ricordare che, quando si parla di diritti, il primo il primo è quello alla vita, perché, se non si è vivi, non si ha nessun altro diritto. Difendiamo quindi anche il diritto alla vita in Europa, oltre che fare questo o quel proclama. Dobbiamo riscrivere le regole sull'agricoltura, le direttive sulla casa e su altri temi. Questo lo abbiamo detto con chiarezza, come lo hanno detto anche i Ministri di questo Governo e del mio Gruppo parlamentare e lo ha detto il Partito Popolare Europeo. Vogliamo un futuro di sviluppo e crescita. Sulla rappresentanza italiana, visto che c'è una polemica, vi è una differenza tra ruolo dei Governi e ruolo dei partiti, non ci sfugge, e noi abbiamo detto che il partito conservatore in particolare ha una storia nobile e importante e deve far parte, secondo noi legittimamente, di una maggioranza,

che ogni tanto qualcuno si misuri con le urne. Il presidente Monti lo ha fatto, non ebbe particolare fortuna quando si cimentò con le urne, ma è sceso in campo e questo è un atteggiamento che va rispettato. Oppure leggo di Enrico Letta, ma non è che se uno perde le elezioni, poi deve avere una poltrona a Parigi o a Bruxelles.

Italia non abbiamo bisogno di dire che la Lega e Fratelli d'Italia sono forze di Governo: lo sono nella realtà democratica e popolare italiana ed europea. Noi, insieme con loro, governiamo Regioni e territori e riteniamo che i paletti vadano messi in altra direzione. Voglio ricordare anche

c'è un *record* di occupazione al 62,3 per cento, la disoccupazione scende al 6,9. Questi sono fatti; non basta, certo, lo sappiamo, ma sono fatti. Quando c'era la politica dell'assistenzialismo e del reddito di cittadinanza, questi risultati erano molto peggiori, perché è l'impresa e l'economia produttiva, quella che l'Europa deve difendere, incoraggiare e non soffocare, che può dare queste risposte. Noi vogliamo difendere le imprese e il lavoro, dalle spiagge, Presidente, delle nostre belle coste alle periferie industriali. Vogliamo un'Europa dei popoli o un'Europa senza popoli e senza elettori, con l'astensionismo? Poi ci si lamenta dell'estremismo, che nasce da un'Europa che non riscalda i cuori e non entra nel cuore

quale avrà il rappresentante nella Commissione europea che il Governo italiano designerà, senza veti e senza barriere. Mi auguro anche che sia un politico, perché i politici hanno esperienza e capacità di misurarsi anche con burocrati, a volte un po' rigidi e ottusi. A volte ce ne sono anche di italiani, presidente Meloni, un po' ottusi, non è solo un *record* di alcuni Paesi esteri. Sono convinto che avremo un portafoglio importante, che conteremo e peseremo nella prossima Commissione

Siamo PPE, ma siamo Forza Italia; difendiamo l'Italia. Guardate che a noi non deve dare patenti nessuno: siamo non soltanto fondatori dell'Unione europea, siamo fondatori della civiltà europea, per cui quello che ci spetta ci dev'essere riconosciuto senza chiedere permessi a nessuno. Andiamo avanti con orgoglio e con coraggio.

«Anatomia di un fallimento». Quest'Europa così vicina e così lontana, Presidente, le era sembrato di poterla afferrare in un attimo ed è sfuggita, è tornata ad essere lontana, come purtroppo lontana la sentono ancora

ancora da troppi italiani costituisce per lei un vantaggio, anche perché non tutti si renderanno conto dello scacco abissale che lei ha subito in queste ore a Bruxelles e che la costringe oggi ad avere una scelta davanti: scegliere di esibirsi in uno di quelli che sono diventati ormai suoi numeri famosissimi, ossia il triplo salto carpiato, una piroetta aerea, oppure arrendersi all'irrilevanza. Esattamente un mese fa, il 26 maggio 2024, lei dichiarava spavalda: il mio obiettivo è costruire una maggioranza alternativa, una maggioranza di centrodestra, e mandare e mandare la sinistra all'opposizione in UE. Oggi si è presentata in Aula ad occhi bassi, senza quella boria che generalmente la contraddistingue; però però il coraggio di dire la verità le è mancato anche poc'anzi. Lei quella maggioranza non l'ha raggiunta ed è stata esclusa dall'accordo con i socialisti e con i liberali, perché lei quella maggioranza non ce l'ha. In quell'accordo, Presidente (le è stato ricordato poc'anzi), ci sono anche i popolari. Lei accusa altri di fantomatici complotti e di comportamenti scorretti, ma ce l'ha alla sua destra, ce l'ha con i suoi alleati: sono loro che hanno fatto quello che lei ha definito degli inciuci e che l'hanno esclusa. *(Applausi)*. Dica la verità agli italiani, abbia abbia il coraggio di dire la verità agli italiani, perché domani quell'accordo che arriva sul tavolo con i nomi di von der Leyen, Costa e Kallas lo hanno chiuso i suoi alleati. È la sua spregiudicatezza che ha portato l'Italia a doversi accontentare di un osso. Capisco che, dopo la fatica fatta di portare von der Leyen in lungo e in largo per tutta l'Italia in processione come una Madonna, lei oggi ci sia rimasta male ma non ha che se stessa con cui prendersela, perché il suo amico Viktor (Orbàn, per chi è un po' meno intimo) ha già dichiarato in maniera altisonante che lui voterà contro. Noi da lei parole di chiarezza invece non le abbiamo ancora ascoltate e quindi si prepara - come dicevo - a due cose: a fare sottobanco accordi con la vituperata sinistra e con gli odiati macroniani (sempre che i macroniani la accettino) oppure a condannare l'Italia all'ininfluenza. Il dilemma che lei oggi ha davanti è questo: tradire o sparire. Questi sono i grandi successi a cui ha portato l'Italia in Europa. Tradire o sparire è lo stesso dilemma che lei affronta qui oggi in Italia, perché, se oggi qualcuno digita sul *web* «Meloni e Regioni» trova due video. In uno c'è Giorgia Meloni che afferma, boriosa e altisonante, che le Regioni vanno abolite, che sono carrozzoni inutili e dispendiosi e quindi vanno abolite. Nell'altro video sembra ci sia sempre Giorgia Meloni, a meno che non sia una sosia, che, in un'atmosfera idilliaca, con uno sbiadito tricolore alle spalle, decanta le lodi dell'autonomia differenziata. Allora ci dica chi è Giorgia Meloni: quella che voleva abolire le Regioni o quella che oggi è costretta a decantare le lodi dell'autonomia differenziata, sogno proibito della vecchia Lega Nord? In quel video

che ha paura che tutto le si frantumi tra le mani, perché il gioco spregiudicato e pericoloso, Presidente, che lei ha intrapreso, stringendo questo patto di potere scellerato con i leghisti, rischia di farle saltare tutto il banco. E lei questo lo sa benissimo. In quel video si rivolgeva ai suoi si rivolgeva ai suoi deputati del Sud, che tutti i giorni sono bersagliati per via dell'autonomia differenziata. *(Applausi)*. Si rivolgeva al suo elettorato del Sud, si rivolgeva ai vari Occhiuto d'Italia, ai suoi alleati, che le stanno dicendo: Presidente, si fermi, perché questo progetto è deleterio. Lei è deleterio. Lei ha cercato di arrampicarsi e di accusare chiunque, ha parlato di complotti, ha dovuto fare l'eziologia e la genesi dell'autonomia differenziata, spiegando che la colpa è di tutti, tranne che la sua. Presidente, la responsabilità politica dell'attuazione dell'autonomia differenziata oggi è in capo a lei. Non sfugga alle sue responsabilità: è tutta in capo a lei. Inutilmente sventolava quel tricolore sbiadito alle spalle; tricolore che infatti, non a caso, è stata proprio la causa scatenante dell'aggressione squadrista alla Camera, attraverso i suoi sodali *(Applausi)*; aggressione squadrista per la quale - lo ripeto per l'ennesima volta - non abbiamo ancora sentito parole di condanna. Anche questo denota la sua debolezza. Anzi, lei ha capovolto le responsabilità: ha parlato dei provocatori anziché parlare dei brutali picchiatori e non ha speso nemmeno una parola per quel Ministro, che guarda caso corrisponde con il promotore dell'autonomia differenziata, che di fronte al tricolore è sbiancato e ha fatto tre passi indietro; nemmeno si trattasse del ministro Sangiuliano di fronte ai libri di storia! A proposito di merito e di persone adeguate: lo facciamo dimettere, Presidente, il ministro Sangiuliano? Visto che va in Europa, chieda ai suoi omologhi che cosa fanno quando un Ministro si dimostra palesemente e reiteratamente inadeguato.

se fa dimettere il ministro Sangiuliano, ci garantisca però che al suo posto non ci metterà un cugino, un fratellastro o un cognato, perché della famiglia *Melones* anche basta. La debolezza e l'infingardaggine della sua gestione politica sono evidenti anche dalla reazione scomposta che ha avuto di fronte alla *débâcle* degli ultimi ballottaggi. Anziché ammettere elegantemente la sconfitta, come fanno le persone mature e sicure di sé come fanno le persone mature e sicure di sé *(Applausi. Commenti)*, lei ha mandato avanti due suoi colonnelli, il Presidente del Senato e il Presidente della Commissione affari costituzionali, a dire che le che le regole sono sbagliate e i ballottaggi vanno aboliti. *(Applausi)*. Voi questo fate: quando le cose non girano come volete voi, cambiate le regole. Sono questi il vostro senso della democrazia e il vostro grande senso di rispetto della volontà popolare. Stesso disegno a cui risponde il progetto del premierato: un voto solo, una volta sola, per una persona sola, perché l'elettorato deve disturbare il meno possibile; perché la democrazia è un fastidio.

Meloni ha due facce. C'è una Meloni che vuole abolire le Regioni e c'è una Meloni che vuole fare l'autonomia differenziata. come ha fatto ancora oggi, di due popoli e due Stati in Medio Oriente per Palestina e Israele e poi si astiene su tutte le risoluzioni che chiedono due popoli e due Stati in Israele. C'è una Meloni che dice di volere la pace, ma si accinge oggi ad autorizzare il nono invio di armi. C'è una Meloni che dice di voler cambiare l'Europa, ma quando ne ha avuto la possibilità con il Next generation EU si è astenuta cinque volte, solo perché non era farina del suo sacco; alla faccia del patriottismo. Oggi di nuovo ci ha ripetuto che vanno messi prima gli interessi dell'Italia e poi quelli del partito. C'è una Meloni che aveva dichiarato guerra agli extraprofitti delle banche, ma, appena i banchieri hanno tossicchiato, s'è rimangiata la tassa sugli extraprofitti delle banche. Vagheggia di ripartenza economica, ma sigla il Patto di stabilità che strangolerà l'Italia e che la condannerà a 12 miliardi di tagli annui su istruzione, sociale e sanità. C'è la Meloni del G7 che sigla il patto di 50 miliardi di euro ancora in armamenti.

Il suo gioco è chiaro, ma non è chiaro soltanto a noi; è stato chiaro anche a una donna molto influente nella sua maggioranza, Marina Berlusconi. Ha sentito il siluro che le ha tirato questa mattina Marina Berlusconi, signora Presidente? Ha sentito le…

con la linea del Governo, la sua. Dice che in tema di aborto, di fine vita e di diritti LGBT si sente più in sintonia con la sinistra di buonsenso, perché ognuno dev'essere libero di scegliere. Dice che il successo alle europee di movimenti con idee antidemocratiche non può non allarmare. Se non è una mozione di sfiducia,

e quello che sta succedendo in Europa in questo momento, purtroppo, sta mettendo in evidenza il fatto che questa Unione europea non ha compreso o quantomeno ha iniziato e vuole proseguire sul declino intrapreso già negli ultimi tempi. In un momento così difficile

e quindi naturalmente più fragile, denotando un'Europa senza anima, con divisioni interne, che addirittura portano a far sì che alcune formazioni politiche dicano che con i conservatori e con Identità e Democrazia non si debba parlare perché sono di destra e che con alcuni Paesi Paesi fondatori come l'Italia non si debba parlare perché c'è un Presidente del Consiglio di centrodestra che non risponde a determinate esigenze. La domanda vera è se siamo sicuri non finirà per indebolire l'Europa a livello internazionale e quindi per fare il gioco della Russia. Non tanto i movimenti sovranisti rischiano di fare il gioco della Russia, ma questa Europa divisa, che non capisce e non comprende che in un momento simile

Signori, è inevitabile, è un copione che abbiamo già visto: perdono le elezioni, cercano di dividere i vincitori, demonizzano una parte, così da continuare a fare il bello e il cattivo tempo, senza capire quello che sta succedendo non solo in Europa, ma nel mondo, in un momento di grandissima difficoltà internazionale come quella che si sta vivendo ora. Si mostrano poco rispetto per un Paese fondatore e poco rispetto per i cittadini che hanno chiesto un cambiamento. Forse ha ragione la Lega nel sostenere che bisogna lavorare a tutti i costi per costruire un'alternativa, se questa Europa vuole avere ancora un futuro e vuole diventare anche protagonista

all'ultima spiaggia, se pensiamo che è più interessata alle nostre concessioni demaniali piuttosto che a proteggere il fronte Sud dell'Alleanza *(Applausi)*, quel Mediterraneo allargato oggi in mano a Paesi ostili, che utilizzano l'immigrazione clandestina come arma ibrida contro l'Italia e contro tutta l'Europa. Quanta miopia c'è in questo momento in questa Unione europea? Ci auguriamo davvero che si possa costruire un'alternativa e che si possa riportare la ragione in un continente che la sta perdendo giorno dopo giorno. Sul tema degli strumenti comuni del finanziamento, a prescindere dalle finalità, ci teniamo a dire che bisogna tenere alta l'attenzione; lo diciamo al Governo, perché non diventino scelte obbligate, finendo poi per comprimere ancora di più la sovranità nazionale, la cui eventuale cessione - ricordiamolo - resta sempre nelle mani di una decisione di carattere politico e non tecnico; per questo motivo, il Parlamento dev'essere centrale

non eletti e, tra l'altro, anche dotati di un'immunità che viene chiamata funzionale (funzionale per modo di dire, se andiamo a vedere l'immunità riservata a questi signori). strumenti comuni legati all'industria europea della difesa, ma noi riteniamo che il miglior strumento di difesa comune sia la diplomazia, che va riscoperta e deve tornare a far parte del nostro modo di ragionare. Anche su questo, l'idea di affidare la diplomazia europea ad un falco anziché a una colomba in un momento come questo la dice lunga:

la sconfitta di Macron e Schölz dopo quello che hanno detto per tutto il tempo della campagna elettorale, quindi non aver capito quello che i cittadini e i popoli europei hanno cercato di mettere in campo. Vorrei parlare dell'Ucraina, così ci chiariamo una volta per tutte, visto che ho sentito qualcuno dire che in maggioranza servono chiarimenti (non solo in maggioranza, ma anche all'opposizione). Cominciamo a fare chiarezza noi. giustissimo muoversi all'interno delle alleanze tradizionali (ci mancherebbe altro) e all'interno dell'atlantismo e assicurare il sostegno europeo all'Ucraina in tutte le sue forme, com'è scritto nella proposta di risoluzione che ci accingiamo a votare, scongiurando ulteriori avanzate russe. Certo, ma va fatto con buonsenso, evitando anche incidenti che possano portare ad un'*escalation* che sarebbe drammatica non solo per tutta l'Europa, ma per tutto il mondo.

per evitare che ci sia un coinvolgimento diretto da parte della NATO nel conflitto. Spiegatemi una cosa, così ci chiariamo: se qualcuno non è d'accordo, alzi la mano e lo faccia in questo momento. Affermare che, parallelamente al sostegno alla difesa ucraina, si debba aprire un canale diplomatico ufficiale che possa cominciare a far sì che l'Ucraina e la Russia tornino a parlarsi *(Applausi)*. Ditemi se qui dentro c'è qualcuno che è contrario a una proposta simile: alzi la mano, sono qui per vedere. Visto che ci dobbiamo chiarire, facciamolo in modo definitivo. È un tale dramma ritenere che, parallelamente alla resistenza ucraina, si possa aprire questo canale diplomatico? Del resto, a qualcuno forse è sfuggito che lo stesso ministro ucraino Kuleba ha ammesso che arriverà il momento - uso le sue parole - in cui sarà necessario parlare con la Russia. Certo, senza confondere aggressore con aggredito, ma a tal proposito il nostro auspicio è che alla prossima conferenza di pace alla prossima conferenza di pace venga invitata anche la Russia, non perché siamo amici di Putin, ma perché siamo amici del popolo ucraino, che da due anni è stremato e perde cittadini e civili tutti i giorni, così come il popolo russo; e siamo ugualmente amici dei popoli europei, che stanno pagando a caro prezzo e che potrebbero pagare di più la continuazione di questa guerra. di questa guerra. È questa la verità: bisogna avere anche il coraggio di sostenere queste cose e di andare contro il politicamente corretto sostenuto da tutti, che in quest'Aula dicono certe cose e poi nei corridoi sostengono esattamente il contrario. È per questo che l'Italia, parlando con le grandi potenze - questa è la vera sfida che ci può aspettare - ed anche con il Consiglio di sicurezza dell'ONU, può giocare un ruolo di ricostruzione, di garanzia, di sicurezza e di neutralità dell'Ucraina.

che dia fastidio sentire la verità! Tra tanti *leader* internazionali zoppicanti, il presidente del Consiglio Meloni può trovare la forza e il coraggio di intraprendere questa linea. Kissinger, grande diplomatico, diceva che l'Ucraina doveva diventare un ponte tra l'Occidente e l'Oriente e non l'avamposto dell'uno contro l'altro. L'Italia ha questa capacità storica di mediazione e, anche grazie alla sponda della Santa Sede, che sta giocando un ruolo importante sulla diplomazia,

sul tema delle riformulazioni, preferiamo rimanere al testo originale, perché pensiamo sia il momento di essere molto netti, soprattutto quando si affronta un Consiglio europeo delicato come questo. Ed è bene che emerga con chiarezza la posizione del Partito Democratico, anche per aiutare e sostenere lo sforzo del Governo che, quando va all'estero, è anche il nostro Governo, che quindi speriamo sempre abbia successo quando è nei *forum* internazionali. Se ha successo il Governo, ha successo l'Italia e noi ce ne compiacciamo. Parto da qui per dire che che accettiamo la sfida della Presidente del Consiglio, quando dice che il mondo è cambiato e chiede se l'Europa deve rimanere uguale. No: noi pensiamo che l'Europa debba cambiare, ci mancherebbe altro. Una crisi economico-finanziaria che ha cambiato i confini dell'Europa dell'Europa e della competizione internazionale; tutta la questione legata al Covid-19 e a come l'Europa ha reagito, unendosi e investendo maggiormente nella dimensione europea; poi, una guerra nel cuore dell'Europa: tutto ciò che è avvenuto chiede più Europa. Noi vorremmo sapere dal Presidente del Consiglio se è d'accordo con quanto scrive Letta nel suo rapporto sul completamento del mercato interno. Noi vogliamo sapere se è d'accordo con Mario Draghi e con il suo rapporto sulla competitività,

partiti sovranisti, alcuni dei quali parte della famiglia europea presieduta dalla Presidente del Consiglio e dal vice ministro Salvini. Lo ricordo perché, quando bisognava investire su più Europa, purtroppo siamo stati da parti diverse. Il Partito Democratico era dalla parte di chi investiva *(Applausi)* e dall'altra parte c'era chi ha fatto la campagna elettorale gridando meno Europa. Vale su questi temi, che sono fondamentali per il futuro del nostro Paese: mercato finanziario dei capitali, unione fiscale e capacità di investire sul debito comune, grande conquista del Governo precedente, che voi dovreste rivendicare. Ci dovete dire se siete d'accordo o no sul lavoro che abbiamo fatto nel passato Governo per portare a casa il PNRR e per investire in quella dimensione

ma la politica chiede non di fare solo la critica, ma di indicare gli strumenti. Noi vogliamo capire se è d'accordo su quello che dice l'Europa, ossia di investire maggiormente sul *green deal* europeo e su come farlo. Certamente va governato, perché sappiamo bene che le case le case vanno efficientate. Sappiamo bene che, se si vuole andare verso l'auto elettrica, bisogna mettere in campo soldi e politica industriale e costruire una filiera. Bisogna mettere dazi temporanei sulla Cina. Sappiamo benissimo che dobbiamo fare un nuovo Sure, debito comune per assistere e costruire una cassa integrazione che ci permetta di governare, da questo punto di vista, la transizione ecologica e digitale. Allo stesso modo, sull'unione sanitaria abbiamo imparato la lezione della pandemia. Apro e chiudo una parentesi: sarebbe stato bello, a proposito di costruire terreni comuni, che proprio in queste ore la legge a prima firma della segretaria Schlein sulla difesa della sanità pubblica avesse avuto esito diverso e voi *(Applausi)*. Non è con i meccanismi e con gli espedienti tecnici di dire che non ci sono coperture che si affronta il tema. Se è un terreno su cui ci riconosciamo tutti, quello della difesa e della tutela della sanità pubblica, cerchiamo di trovare soluzioni comuni. Ugualmente, siamo disponibili a fare una battaglia comune sul tema dell'assegno unico. A noi piace ricordarla come la legge Delrio, che ha investito molto del lavoro della passata legislatura. Come Partito Democratico, rivendichiamo di aver lavorato con quel Governo sull'assegno unico. Invitiamo la Presidente del Consiglio a rivedere i conti e le coperture, perché sono molto meno, purtroppo, di 3 miliardi; ce ne vorrebbero molti di più per assistere e costruire un nuovo *welfare* che permetta a uomini e donne di farsi maggiormente carico della condivisione lavoro-famiglia, perché deve spettare a entrambi, uomini e donne, motivo per cui noi insistiamo sul congedo paritario. Lo stesso vale sull'Ucraina: in maniera sintetica, noi siamo per continuare con ogni mezzo necessario il sostegno all'Ucraina finché sarà necessario, per arrivare a una pace duratura e stabile. A volte uno dice: perché questo Governo rischia di rimanere isolato in Europa? Basterebbe sentire gli interventi del collega Borghi e del collega Romeo sui fondamentali della politica estera, della costruzione e della risposta alle sfide comuni, La risposta non è uscire dall'Europa. La risposta non è andare per conto proprio, ma investire maggiormente nella dimensione europea. Questo vale per il lavoro che è stato fatto. Io do atto anche di un lavoro diplomatico importante fatto all'interno del G7 per allargare anche a Paesi fuori fuori dalla sfera occidentale. Non si arriva a una pace duratura pensando di aprire un canale direttamente con Putin; lo si fa ampliando la sfera dei contatti e delle relazioni diplomatiche, andando oltre quel rischio che c'è, ossia «*the West against the rest*». Bene che a Bürgenstock, dove ha partecipato la Presidenza del Consiglio, siano state invitate anche le espressioni delle democrazie e anche di quei regimi più forti del Sud del mondo, perché noi non possiamo pensare di giocare la partita Occidente contro Oriente. Questo è il salto di qualità che bisogna fare: non aprire un canale preferenziale con Putin, che dà l'idea che noi indeboliamo il fronte delle democrazie liberali, che invece è stato un *plus* da questo punto di vista. Accanto agli Stati Uniti, investendo nell'autonomia strategica europea, pilastro europeo, abbiamo il dovere, anche in questo senso, di stare accanto agli americani nel sostenere con forza e determinazione il piano Biden per Gaza, con una forte pressione. Io penso che il Governo italiano abbia un ruolo importante in Europa per costruire una posizione comune, sia per chiedere che ci sia con forza una determinazione europea per evitare l'escalation nel Libano (siamo molto preoccupati per la violazione della risoluzione 1701/2006 Da questo punto di vista, l'Europa può e deve prendere una soluzione. Anche qui Orbán va convinto, perché io capisco che non può diventare il capro espiatorio di tutti i mali in Europa, ma di certo è un problema in alcuni passaggi. Lo abbiamo visto sui 50 miliardi per l'Ucraina, l'abbiamo visto su alcuni passaggi del PNRR e l'abbiamo visto sulle posizioni europee nel sostegno all'Ucraina. Signora Presidente del Consiglio, quando lei era assente ho detto che dobbiamo decidere da che parte stare. Le ambiguità ce le abbiamo tutti, le abbiamo tutti, le abbiamo anche noi e sappiamo che le dobbiamo risolvere, se vogliamo tornare al Governo del Paese. Adesso però è lei al Governo del Paese e a queste ambiguità deve rispondere: sta dalla parte di chi chiede più Europa o dalla parte di chi chiede meno Europa? Questa è la sfida principale e ci deve dare una risposta, da questo punto di vista. Vale sul Medio Oriente: penso che dobbiamo stare accanto agli Stati Uniti e dobbiamo fare un passo in più. Della prospettiva di due popoli, due Stati ci siamo riempiti tutti la bocca. Non basta più: abbiamo bisogno di dare un segnale più forte. Per fare questo, noi, perché siamo amici del popolo israeliano, sappiamo che Netanyahu sta diventando un problema per il popolo israeliano. Allora, per dare seriamente solidità a quella prospettiva, pensiamo che a livello europeo una posizione importante e comune per il riconoscimento dello Stato palestinese aiuti a dare un segnale molto forte nel senso che noi siamo amici del popolo israeliano e proprio per questo andiamo a stigmatizzare i comportamenti peggiori di Netanyahu che allontanano la pace e una soluzione. Invece noi, insieme all'alleato americano e ai Paesi europei, possiamo esercitare un ruolo. Per fare questo, serve un salto di qualità. Ha ragione a dire che a volte è un gigante burocratico quest'Europa; deve diventare un gigante politico-economico. Dobbiamo affrontare il tema delle riforme. Dicevo poco fa al ministro Fitto poi dobbiamo prendere posizione su una convenzione o su una conferenza intergovernativa, perché è vero, l'Europa va cambiata e serve più Europa, da questo punto di vista. Diritto di iniziativa legislativa del Parlamento europeo: siete d'accordo o non siete d'accordo? La facciamo insieme questa battaglia? A proposito di democrazia, prima ci ha fatto una bella lezioncina di democrazia europea. Forse la stessa enfasi enfasi e la stessa passione ce l'aspettiamo nei confronti di autorevoli rappresentanti della maggioranza, quando gli ricorderà che, quando si perdono le elezioni amministrative, si può ammettere di aver perso e non si cambiano le regole del gioco Da ultimo: equilibri generali. Io seguo il suo ragionamento e, se fosse quello il ragionamento sui risultati delle elezioni del Parlamento europeo e lo applichiamo alla politica italiana, noi siamo la seconda forza. Allora dovremmo essere al Governo con voi? No, è evidente che a livello a livello europeo si costruiscono delle condizioni e si costruiscono degli accordi sulla base della condivisione di un'idea d'Europa. *(Applausi)*. Socialisti, liberali e Partito popolare europeo hanno investito sulla costruzione europea non da adesso, ma da tanti anni. Voglio ricordare quell'immagine bellissima del settembre del 1984, quando Helmut Kohl e François Mitterrand, insieme, mano nella mano, davanti al memoriale di Verdun, dissero: mai più barbarie della guerra, perché in Europa non ci potrà essere più. *(Applausi)*. Ed erano della famiglia del Partito popolare europeo e dei socialisti. Dentro quella tradizione politica contro il nazifascismo è nata quella coalizione; certo, anche per la gestione di equilibri di potere, ma è nata lì e dentro quel perimetro. Ve l'ha ricordato prima di tutti Tusk. Cosa diversa invece - e vado a concludere è il lavoro che lei dovrà fare e che ci auguriamo abbia successo. Noi tifiamo per l'Italia e tifiamo per lei, perché l'Italia possa avere il migliore dei commissari europei possibili, con una delega pesante, come è stato negli anni passati. Antonio Tajani, che è stato Presidente del Parlamento europeo. E vorrei ringraziare, a nome delle senatrici e dei senatori del Partito Democratico, il lavoro importante e straordinario fatto da Paolo Gentiloni in questi cinque anni *(Applausi)*, per investire nel debito comune, per permettere a lei e al suo Governo di investire sul futuro dell'Europa in maniera diversa. Chiudo con le parole, se mi permette, Presidente, e vado a chiudere, a proposito di questo... a ricordare, da questo punto di vista, un altro grande italiano, che nel 2019 aprì la Presidenza del Parlamento europeo, ricordando come il sogno europeo, oltre ai nazionalismi, abbia portato alla costruzione dell'Europa. Voglio ricordare qui David Sassoli e queste persone che, con passione e con orgoglio, si sono mosse per il sogno europeo. *(Applausi)*. Io auguro a lei, Presidente del Consiglio, di stare nel solco delle capacità, della qualità umana e delle competenze di queste persone, per individuare il nuovo commissario. Noi faremo il tifo per l'Italia.

siamo orgogliosi, come senatori di Fratelli d'Italia, per il modo in cui lei, signor Presidente del Consiglio, rappresenta l'Italia nelle sedi europee e internazionali, non soltanto per le sue capacità e il suo impegno personale, ma per il risultato elettorale che fa dell'Italia un'eccezione a livello dei grandi Stati europei, perché è l'unico

governiamo in più città di quante ne governassimo prima. Per cui, insomma, parlare di *débâcle* mi sembra francamente arrischiato ovvero falso. Il nostro Presidente del Consiglio arriva in sede europea con il prestigio dovuto a questo risultato elettorale e ai risultati ottenuti dal Governo: i *record* di occupazione che si susseguono mese dopo mese, il *record* dell'occupazione femminile, i *record* sugli obiettivi colti con il PNRR. Vedo qui il ministro Fitto, che ha fatto un enorme lavoro su questo tema.

Quando il Governo Meloni ha iniziato il suo lavoro era lo Stato europeo con l'inflazione più alta. Di passaggio dico che era all'11,8 per cento, mentre oggi è sotto l'uno per cento: c'è stata una tendenza generale alla discesa dell'inflazione, ma dai massimi ai minimi, quindi evidentemente il Governo anche qui ha lavorato bene. Lo *spread* è al di sotto del livello di tutti gli ultimi Governi precedenti. L'Italia con il Piano Mattei ha dato una svolta in politica internazionale; dopo decenni in cui l'Africa veniva ignorata, ora, non soltanto per l'Italia ma per l'Europa e a livello internazionale, c'è nuovamente questa attenzione. Forse esageriamo nell'essere sobri parlando delle cose fatte, ma pochi mesi fa in quest'Aula c'erano decine di Capi di Governo e Capi di Stato africani invitati dal nostro Governo *(Applausi)* che hanno segnato una svolta, un momento storico di di cui tendiamo a non parlare tanto perché pensiamo sempre a quello che c'è da fare da oggi in poi. Intanto questo è stato fatto ed è stata segnata una svolta. in vista di questo vertice, ci sono già fin d'ora diversi successi da segnalare, ad esempio il fatto di avere inserito nel preambolo dell'agenda di questo vertice il principio di sussidiarietà, troppo spesso dimenticato da chi vorrebbe un'Europa che decide tutto, come è stato detto, ossia da come dobbiamo mangiare all'auto che dobbiamo guidare.

Sull'immigrazione in generale si è cambiato finalmente il parametro. Ora finalmente si è tornati al principio fondamentale, e cioè che in Europa - e noi diciamo soprattutto in Italia - si entra legalmente e non attraverso il traffico dei trafficanti di esseri umani, che sono dei criminali ed anche fiancheggiatori del terrorismo. Questi sono aspetti estremamente importanti che vanno ben al di là delle nomine che potranno avvenire in questi giorni.

per intervenire su percentuali bassissime del nostro patrimonio edilizio. *(Applausi)*. Quello sì che ha creato del debito, non certo le politiche per lo sviluppo che hanno fatto sì che l'Italia abbia numeri migliori della media dell'Europa. Un altro punto è stato

una parte di quegli elettori non sono andati a votare per nulla, un'altra parte evidentemente ha votato per Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra, che hanno migliorato le loro posizioni.

Ricordo anche la necessità della deregolamentazione, citando il famoso detto secondo cui l'America innova, la Cina copia, copia, e l'Europa regolamenta e dunque spesso mette degli ostacoli enormi a chi vuole produrre o anche ai comuni cittadini che vogliono semplicemente vivere, avere una casa, magari un'automobile. Ebbene questa iper-regolamentazione va certamente combattuta, il presidente Meloni ha proposto ha proposto l'idea che ci sia addirittura una delega specifica sulla deregolamentazione. Sono cose estremamente importanti, perché non può essere un caso che l'Europa da troppo tempo sia l'area del mondo che meno cresce dal punto di vista economico rispetto a tutte le altre. Evidentemente bisogna cambiare, invertire la tendenza e andare avanti su una posizione che veda l'Italia protagonista, un'Italia che non sta col cappello in mano a correre dietro al famoso duo Francia-Germania, il quale è in è in grave difficoltà perché, a differenza di quanto è avvenuto da noi, gli elettori hanno bocciato in modo molto severo le maggioranze di governo. I due partiti principali di governo di Francia e Germania insieme raggiungono la sola percentuale di voto di Fratelli d'Italia, e in più noi abbiamo degli degli alleati che ci fanno andare evidentemente molto più in alto. Noi siamo con lei, presidente Meloni, nel suo impegno per un'Europa che, come volevano i padri fondatori De Gasperi, Schuman e Adenauer, faccia ciò che conviene fare insieme e lo faccia bene e non tolga agli Stati la loro autonomia e la loro identità. I senatori di Fratelli d'Italia sono con lei, presidente Meloni, per far valere le ragioni di chi alle elezioni, non soltanto in Italia, ha votato per un cambiamento in Europa, per far valere l'interesse nazionale e di tutti gli italiani di fronte a chi a Bruxelles sembra ragionare sembra ragionare in termini di potere di partito e non per il bene comune dei cittadini. Siamo con lei con orgoglio e determinazione, mi permetto di dire con ammirazione per la dedizione totale con con la quale sta interpretando il suo ruolo di rappresentare al meglio l'Italia in Europa e nel mondo.

Non tolgo la seduta perché vi sono gli immancabili interventi di fine seduta, che la vice presidente Ronzulli è ben lieta di seguire.

nel cielo e nel mare di Ustica quella sera del 27 giugno 1980. Il mio pensiero innanzitutto va alle vittime, ai loro familiari e a coloro che, come Daria Bonfietti, anche da questi banchi, insieme alla sua associazione, si è sempre battuta e si batte per mettere finalmente la parola fine a menzogne e depistaggi, per affermare finalmente quella che ormai riconosciuta da tutti (o quasi tutti) come la verità. Quella sera ci fu una vera e propria azione di guerra sotto copertura e poi sotto occultamento di prove, di tracciati radar, di testimonianze e perfino di morti e suicidi sospetti, di persone che sapevano e non dovevano parlare; un'azione di guerra che vide protagonisti aerei di Paesi alleati. Si pensava che dentro quel Mig libico, che per proteggersi volava sotto la traiettoria dell'aereo DC Itavia, partito alle ore 20,59 da Bologna per Palermo, ci fosse il presidente Gheddafi, che doveva essere colpito. L'azione di fuoco fu documentata da inchieste, sentenze e ordinanze, come quella del giudice Priore, da sentenze in sedi civili, che hanno condannato lo Stato con la motivazione che non ha saputo proteggere la sicurezza dei voli, da esami di tracciati NATO, azione ammessa o indicata anche da ex Presidenti della Repubblica, come Cossiga, o indicata da statisti come l'ex presidente del Consiglio Amato. Quell'azione di fuoco fu esercitata da quegli aerei alleati, francesi, belgi e americani, comunque NATO; ad essere colpito fu il DC Itavia, a morire furono 81 persone. Fu un'inchiesta giornalistica, quella condotta da Andrea Purgatori, che manca a questo Paese e che ricordiamo con stima e gratitudine anche per questo, a indicare da subito la verità, occultata e depistata per troppi anni. Anche ieri sera - mi avvio a concludere - c'è stata una nuova inchiesta, condotta dal giornalista Giletti, a fornire ulteriori testimonianze, tra cui quella dell'ex addetto militare dell'ambasciata di Francia a Roma. Cos'altro impedisce la verità allora? C'è solo da mettere finalmente la firma di quella strage. È la Francia, innanzitutto, che deve ammettere cosa accadde quella sera ed è il Governo italiano, anche alla luce dei nuovi elementi, che dovrebbe subito, con determinazione, chiedere pretendere dal Governo francese una cosa semplice e importante: l'ammissione della verità. Abbiamo presentato come Gruppo PD un'interrogazione in questo senso. Chiediamo questa iniziativa immediata del Governo e chiediamo che il ministro Tajani venga a riferire. PRESIDENTE. Abbiamo chiesto di muoversi. Domani mattina - e ho finito, Presidente - saremo, come altre volte, a Bologna, alla cerimonia di commemorazione di quella strage. Anche lì risuonerà…*(Il mi faccia concludere. Anche lì risuonerà questa richiesta: basta con i depistaggi. Allora, Presidente, si provi a ricucire quella ferita di familiari e del Paese nell'unico modo possibile: il rispetto del dolore, della dignità e della verità.

una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1997 per riflettere sulle sofferenze indicibili che troppe persone nel mondo continuano a subire a causa di regimi repressivi e fintamente democratici. Oggi è anche un momento per riaffermare con forza il nostro sostegno ad ogni azione politica, istituzionale e sociale che vada verso l'eradicazione totale di questa pratica disumana e inaccettabile. La tortura è una violazione dei diritti umani fondamentali e un attacco alla dignità umana che non possiamo tollerare in nessun contesto. È importante ricordare che nel 2017 l'Italia ha introdotto nel proprio ordinamento il reato di tortura, segnando un passo cruciale nella nostra legislazione. Oltre confine, 173 Nazioni hanno ratificato la Convenzione contro la tortura e 108 sono quelle che hanno adottato leggi specifiche. Tuttavia, dobbiamo riconoscere che c'è ancora molto da fare, in questo come in molti altri Paesi, in alcuni casi, le leggi esistenti non rispecchiano pienamente la definizione fornita dalla Convenzione. Ora, in tre minuti, non posso affrontare bene questo argomento. Conosciamo fin troppo bene tante violazioni dei diritti umani perpetrate nel mondo, dall'Iran a Cuba. Ma oggi voglio soffermarmi su una specificatamente, della quale si parla sempre troppo poco: la drammatica situazione dei praticanti del Falun Gong in Cina. Il Falun Gong è uno stile di vita basato su princìpi di verità, compassione e tolleranza, quindi una filosofia dell'esistenza pacata e tranquilla; una religione diffusasi a partire dal 1992, che in breve ha coinvolto tra i 70 e i 100 milioni di praticanti cinesi. Tuttavia, nonostante la sua natura pacifica e meditativa, le autorità cinesi hanno avviato una campagna di repressione disumana e sistematica contro i suoi aderenti. Più di 100.000 persone sono state inviate in campi di rieducazione, 5.000 imprigionate e condannate a pene detentive superiori a diciotto anni. Soprattutto, oltre agli arresti immotivati, alle umiliazioni indescrivibili e agli abusi sessuali, i cinesi praticanti del Falun Gong subiscono pratiche crudeli come l'espianto coercitivo di organi, tolti a persone vive senza anestesia. Il nostro impegno contro la tortura deve essere incondizionato e continuo e deve riguardare i i praticanti del Falun Gong come le altre minoranze in Cina (gli uiguri, i tibetani e i cristiani). Dobbiamo sostenere tutte le iniziative volte a garantire la democrazia, la libertà religiosa e la libertà di espressione, ribadendo la nostra ferma condanna della violazione dei diritti umani in Cina. Concludo dicendo che in questa giornata rinforziamo il nostro sostegno alle vittime, promettendo di lavorare instancabilmente, come istituzione, per un mondo libero dalla tortura e da ogni atto violento e atroce che umilia la persona e la sua dignità.

abitanti. Questa comunità è stufa di rimanere vittima di un degrado ambientale che da anni mette a rischio la salute di migliaia di cittadini e la salubrità dei luoghi. Ricordo che il MoVimento 5 Stelle da oltre dieci anni conduce battaglie ambientaliste per ottenere la bonifica dei luoghi e delle discariche contaminate presso l'ottava municipalità di Napoli, organizzando diversi sopralluoghi che hanno coinvolto anche i parlamentari, oltre a numerosi cittadini partenopei. Tuttavia ancora oggi, dopo anni di lotte, mi giungono notizie che non avrei mai voluto sentire e che vedono coinvolte la seconda, la settima e l'ottava municipalità di Napoli. Infatti, nelle ultime settimane, sotto la lente di ingrandimento della procura della Repubblica di Napoli è finita anche Cava Suarez, invaso un tempo usato per estrarre tufo e successivamente, stando agli inquirenti, utilizzato come enorme discarica abusiva. Al suo interno, secondo le indagini, sarebbero stati rinvenuti amianto e metalli pesanti, per una mole di rifiuti pericolosi pari a circa 270.000 tonnellate. L'aspetto più grave è che i rifiuti, per effetto delle piogge, si sarebbero sicuramente poi dispersi anche in altre zone, scivolando a valle verso il vallone di San Rocco, tra i quartieri di Miano e Capodimonte, zone densamente popolate di Napoli (settima e seconda municipalità). Mi chiedo e vi chiedo: noi istituzioni come possiamo tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini, se, pur sapendo di questo disastro ambientale, ci si gira dall'altra parte? C'è un unico modo, secondo me: intervenire immediatamente stanziando delle risorse per una bonifica immediata. Per questo motivo, non posso che fare mie le parole di Nicola Nardella, presidente dell'ottava municipalità di Napoli, secondo cui a farsene carico deve essere necessariamente il Governo, perché nessuna delle istituzioni locali potrà da sola garantire la messa in sicurezza e la bonifica di un'area che che nel 2008 ha già maturato un credito ambientale enorme nei confronti dello Stato italiano, ospitando una discarica per l'emergenza dei rifiuti. Presidente, onorevoli colleghi, i cittadini napoletani meritano rispetto. Per questo motivo depositerò un'interrogazione parlamentare in cui chiedo al Ministro dell'ambiente e della sicurezza di risolvere immediatamente queste criticità, così da tutelare l'ambiente e la salute umana, invitando il Governo ad utilizzare ogni risorsa a disposizione, dai fondi del PNRR alla dotazione previsti per i siti orfani, così da bonificare cava Suarez e gli altri siti inquinati di Chiaiano. Inoltre, ho chiesto al Ministero di avviare un'attività ispettiva al fine di accertare le responsabilità connesse all'inquinamento di cava Suarez e se il Ministero intende costituirsi parte civile. Auspico di avere delle risposte esaurienti e in tempi celeri, nell'interesse di migliaia di campani e delle future generazioni, che non chiedono privilegi, bensì il rispetto dei propri diritti inalienabili. Come recita nei primi due capoversi l'articolo 32 della Costituzione: «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività».

si sono battuti tantissimo su tutto il territorio a livello nazionale. È con immensa gioia e profonda soddisfazione che oggi abbiamo avuto la notizia che, dopo anni di ingiustizie e dura prigionia nelle carceri britanniche, il fondatore di Wikileaks Julian Assange è finalmente tornato in libertà. La fine di un vergognoso calvario è considerata una vittoria per la libertà dell'informazione e in generale per i diritti umani e civili, e in parte lo è. è. Soprattutto è la vittoria di chi si è opposto a una brutale ingiustizia e di tutti coloro che hanno impedito che questa vicenda passasse sotto silenzio, proprio qui nel cuore della democrazia occidentale, per colpa di politici pavidi e di tutta un'informazione asservita e sottomessa. È una battaglia che il MoVimento 5 Stelle ha sostenuto sin dall'inizio con determinazione ed estrema convinzione, consapevoli dell'importanza di difendere i princìpi fondamentali su cui si basa una società giusta e trasparente. La vicenda di Assange ha sollevato questioni cruciali sul diritto alla verità e sulla protezione delle fonti giornalistiche. La sua è una lotta per la trasparenza che ha ispirato molti e che ha evidenziato la necessità di un giornalismo di un giornalismo libero e indipendente, capace di svelare le verità scomode e di mettere i potenti sotto controllo. La libertà di Assange è anche un segnale forte a tutti coloro che si battono per la giustizia e la verità. Desidero ringraziare soprattutto tutte le persone che, a livello mondiale e globale, si sono prodigate con passione e determinazione per questa nobile causa. Senza il loro impegno e senza la loro perseveranza Assange non avrebbe mai potuto riabbracciare i propri cari. A livello internazionale, la solidarietà e la mobilitazione hanno dimostrato che l'unione delle forze può portare grandi risultati e che la voce della giustizia non può essere soffocata. Alla moglie di Assange, Stella, e ai suoi figli esprimiamo tutta la nostra vicinanza e il nostro affetto. Ci uniamo a loro in questo momento di gioia. Sono passati oltre dieci anni e la loro forza e il loro coraggio sono stati un esempio e un faro per tantissime persone. La loro sofferenza ci ricorda quanto sia preziosa e importante la libertà e quanto sia fondamentale lottare per questo.

ricordando sempre che la verità e la giustizia devono prevalere su ogni forma di repressione. Viva la libertà.